la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta

nell'intervento di oggi intendo affrontare i temi in discussione nel Consiglio europeo di questa settimana. Si tratta di pandemia e vaccini, transizione digitale, costo dell'energia, migrazioni, commercio estero, impegni internazionali e, in particolare, la COP 26. Dopo un avvio stentato, la campagna di vaccinazione europea ha raggiunto risultati molto soddisfacenti. Nell'Unione europea quasi quattro adulti su cinque hanno ricevuto almeno una dose, per un totale di 307 milioni di persone. In Europa abbiamo somministrato 130 dosi di vaccino per 100 abitanti, a fronte delle 121 negli Stati Uniti. In Italia la campagna procede più spedita della media europea: ad oggi l'86 per cento della popolazione sopra i dodici anni ha ricevuto almeno una dose e l'81 per cento è completamente vaccinata. Voglio ricordare che prima dell'ultimo Consiglio europeo, a fine giugno, meno di un terzo della platea aveva completato il ciclo vaccinale. Oggi, come ho detto, l'81 per cento è completamente vaccinato. Negli ultimi tre mesi e mezzo l'Italia ha dunque vaccinato metà della popolazione con più di dodici anni; uno sforzo straordinario per cui dobbiamo essere grati al nostro sistema sanitario, a partire da medici e infermieri

a partire da medici e infermieri *(Applausi)*, e all'immane opera logistica che è stata compiuta sin dall'inizio di questo Governo. Voglio inoltre ringraziare, ancora una volta, tutti i cittadini che hanno scelto di vaccinarsi, in particolare i giovani e i giovanissimi e anche chi ha deciso di farlo nelle scorse settimane, dopo aver superato le proprie esitazioni. La curva epidemiologica è oggi sotto controllo, grazie al senso di responsabilità dei cittadini. Questo ci permette di tenere aperte le scuole, le attività economiche e i luoghi della nostra società. Il Consiglio europeo riaffermerà il proprio impegno a contribuire alla solidarietà internazionale in materia di vaccini. Dobbiamo incrementare la fornitura di dosi ai Paesi più fragili, perché possano proteggere i loro cittadini e per impedire l'insorgenza e la diffusione di nuove e pericolose varianti. Solo il 2,8 per cento di chi vive in un Paese a basso reddito ha ricevuto almeno una dose di vaccino, a fronte di quasi il 50 per cento della popolazione mondiale. L'Italia ha recentemente triplicato le donazioni di vaccino, da 15 a 45 milioni di dosi, da distribuire principalmente attraverso il meccanismo Covax. Ad oggi abbiamo assegnato più di 11 milioni circa 3 milioni ciascuno a Vietnam e Indonesia, un milione e mezzo all'Iran, 700.000 dosi a Libano, Yemen e Iraq. Poi segue un lungo elenco di Stati: l'Albania con 188.000 dosi, l'Uganda con 488.000, la Libia con 261.000, poi la Macedonia, la Costa d'Avorio, l'Algeria. Al Consiglio d'Europa discuteremo inoltre dell'approccio europeo per affrontare e superare eventuali future pandemie. Al Global Health Summit dello scorso maggio abbiamo firmato la Dichiarazione di Roma, che ci impegna a migliorare la condivisione di dati e conoscenze a livello globale. Dobbiamo investire nella scienza e nella ricerca, che ci hanno permesso di avere vaccini efficaci e sicuri in pochi mesi. A settembre la Commissione europea ha inaugurato l'HERA, l'Autorità europea per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie. Il suo scopo è migliorare il coordinamento interno all'Unione, sia nella preparazione che nella gestione di crisi future. Si occuperà, ad esempio, dell'attivazione di misure di emergenza per lo sviluppo, l'approvvigionamento e la distribuzione di prodotti medici e sanitari. Dobbiamo evitare il ripetersi dei pericolosi episodi di protezionismo sanitario a cui abbiamo assistito nei primi mesi della pandemia. Continueremo a lavorare per migliorare la risposta globale a future crisi sanitarie e in tutte le sedi multilaterali appropriate. Per quanto riguarda l'Agenda digitale, il Consiglio intende definire la tabella di marcia per gli obiettivi del 2030, anche con l'indicazione di scadenze e di un sistema di monitoraggio. Gli obiettivi europei per il 2030 riguardano quattro aree prioritarie: infrastrutture digitali sicure, efficienti e sostenibili, trasformazione digitale delle imprese, digitalizzazione dei servizi pubblici e la formazione di competenze digitali. L'Italia ha fatto propri questi obiettivi e ne ha anticipato il raggiungimento al 2026, anche grazie alle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Noi siamo ancora indietro in questo campo, molto indietro, ma intendiamo colmare rapidamente il divario che ci separa dal resto d'Europa e, in alcuni settori, arrivare a guidare la transizione digitale europea. Per farlo abbiamo stanziato 50 miliardi di euro, oltre un quarto della dotazione complessiva del Piano. La Presidenza del Consiglio e i Ministri coinvolti hanno già predisposto meccanismi di verifica sui progressi compiuti. Questi meccanismi

Allo stesso tempo, dobbiamo migliorare la collaborazione tra gli Stati membri dell'Unione europea nel digitale. Vogliamo trovare soluzioni condivise su quattro versanti: la sicurezza cibernetica, la concorrenza, i servizi digitali e l'intelligenza artificiale. Sul fronte della cybersicurezza, il nostro obiettivo è garantire un quadro normativo chiaro e identificare risposte rapide e coordinate. L'Italia, come sapete, si è dotata recentemente di un'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, che promuove lo sviluppo di capacità di prevenzione, monitoraggio, rilevamento e mitigazione. È un tema prioritario per l'Europa, che metterà in campo degli strumenti legislativi appositi. Sulla concorrenza lavoriamo sulle proposte di regolamentazione europea per il mercato e i servizi digitali. L'Italia sostiene la proposta di regolamento sui mercati digitali e ne auspica la pronta adozione. Intendiamo poi fissare adeguate garanzie per la libertà di impresa e di espressione. Occorre assicurare, al contempo, la non discriminazione e la corretta attribuzione delle responsabilità sulla distribuzione e pubblicazione di contenuti e prodotti *online*. L'Italia sostiene il regolamento dell'Unione europea sui servizi digitali, anche per proteggere efficacemente prodotti e contenuti realizzati in Italia. La nostra convinzione è che quello che è illecito *offline* debba essere illecito anche *online*. Infine, sull'intelligenza artificiale il nostro obiettivo è promuoverne la sperimentazione e, soprattutto, renderne l'utilizzo più sicuro e trasparente. Allo stesso tempo, dobbiamo alimentare la fiducia dei cittadini per queste nuove soluzioni tecnologiche. La strategia nazionale sull'intelligenza artificiale, adottata dal Comitato interministeriale per la transizione digitale, costituisce il quadro per migliorare il posizionamento competitivo del nostro Paese. Una sfida decisiva per l'Europa è raggiungere l'autonomia tecnologica nei semiconduttori e nelle tecnologie quantistiche.

ad appena il 9 per cento nel 2021. Dipendiamo sempre di più dalle forniture extraeuropee quando queste ritardano o si bloccano, come è accaduto in questi mesi di ripartenza economica, le aziende possono vedersi costrette a fermare o rallentare di molto la loro produzione. L'Unione europea intende produrre il 20 per cento della produzione mondiale dei semiconduttori entro il 2030; per farlo, dobbiamo intervenire subito e con decisione. La Cina e gli Stati Uniti lo stanno già facendo, investendo decine di miliardi ciascuno in questo settore. Per darvi un'idea, i sussidi statali della Cina e degli Stati Uniti vanno dal 30 al 60 per cento del costo di un impianto di semiconduttori. Questo fa venire alla mente un punto più generale: per fare la transizione ecologica e la transizione digitale non ci sono alternative all'intervento dello Stato; lo Stato non può che essere pienamente impegnato; altrimenti, se non c'è lo Stato, queste due transizioni non avverranno. Questo vale anche nei nostri rapporti con gli altri Paesi dell'Unione europea per quanto riguarda le molte regole che sono state sospese in questo momento.

ho voluto illustrare alcuni punti, forse il punto fondamentale, che bisogna affrontare nella discussione sulla ricostruzione di queste regole. L'Unione europea deve mettere insieme le capacità di ricerca, progettazione, sperimentazione e produzione di tutti i Paesi europei, per creare ad esempio un ecosistema europeo di *microchip* all'avanguardia. Sosteniamo con convinzione la proposta della Commissione dell'Unione europea di adottare uno *European Chips Act* (che è esattamente quello che hanno già fatto gli Stati Uniti con il *Chips Act*) per coordinare investimenti e produzione europei di *microchip* e circuiti integrati. Dobbiamo inoltre agire con la massima urgenza per rafforzare la cooperazione tra pubblico e privato e attrarre investimenti alla frontiera tecnologica. Un altro tema che tratteremo questa settimana è quello del costo dell'energia. Negli ultimi mesi abbiamo assistito a un forte aumento del costo del gas e dell'elettricità. Questi rincari sono dovuti principalmente ai movimenti dei prezzi sui mercati internazionali. La domanda di energia da parte di famiglie e imprese è aumentata a livello europeo e sui mercati asiatici e ha contribuito a ridurre le scorte e le forniture disponibili. Il Governo si è impegnato a contenere il rincaro delle bollette. Lo scorso giugno avevamo già stanziato 1,2 miliardi di euro per ridurre gli oneri di sistema. Poche settimane fa siamo intervenuti ulteriormente con più di 3 miliardi di euro per calmierare i prezzi dell'ultimo trimestre dell'anno soprattutto per le fasce più deboli della popolazione.

quanto entrambe comporteranno dei costi che vanno distribuiti avendo in mente l'eguaglianza. Si tratta di misure immediate a cui dovranno necessariamente seguirne altre di lungo periodo, per migliorare la sicurezza degli approvvigionamenti e prevenire un'eccessiva volatilità dei prezzi. Il 13 ottobre scorso la Commissione ha pubblicato una comunicazione sul tema dell'aumento del costo dell'energia. Il documento descrive gli interventi emergenziali possibili per gestire la situazione attuale e ipotizza soluzioni per rendere le forniture più sicure e affidabili in futuro. Il Governo italiano ha sollecitato la Commissione a esplorare rapidamente l'opzione di acquisti e stoccaggi congiunti di gas naturale su base volontaria con misure di medio periodo. Questa strategia può essere utile per resistere meglio agli *shock* e sviluppare le capacità industriali di deposito. La Commissione presenterà una proposta di revisione del quadro normativo entro dicembre. Il nostro obiettivo di medio termine resta quello di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e aumentare sostanzialmente l'utilizzo di fonti rinnovabili. Vogliamo procedere con la transizione ambientale e rispettare gli obiettivi di decarbonizzazione che ci siamo posti per il 2030 e il 2050. come dicevo prima, lo Stato deve tutelare le fasce più deboli della popolazione dai costi della trasformazione energetica e assicurarsi che i tempi della transizione siano compatibili con le capacità di adattamento delle aziende. Affinché la riconversione del nostro sistema economico abbia successo, è necessario il sostegno di tutti: Istituzioni, imprese e cittadini. Dobbiamo portare avanti un'agenda climatica ambiziosa, facendo in modo che le nostre scelte siano accettate e condivise in maniera ampia dalla popolazione e dimostrando quel che abbiamo detto e che dicono un po' tutti, ossia che la transizione ecologica comporta non necessariamente una distruzione di posti di lavoro, ma - semmai - un ampliamento dell'occupazione. Ci sono alcuni dati che cominciano ad emergere in Paesi che hanno affrontato più rapidamente alcuni passi della transizione e che dal punto di vista dell'occupazione per il momento sono incoraggianti; questo è un punto da tenere presente nella velocità di attuazione di questa agenda climatica. Per quanto riguarda le migrazioni, l'Italia aveva promosso una discussione sul tema nel Consiglio europeo di giugno, con l'obiettivo di incoraggiare una gestione davvero europea dei flussi. Anche i Paesi preoccupati dai cosiddetti movimenti secondari hanno preso atto dell'importanza di prevenire e contenere i flussi irregolari e di incentivare i canali di migrazione legali. Su quest'ultimo aspetto l'Europa dovrebbe impegnarsi di più, seguendo ad esempio il modello dei cosiddetti corridoi umanitari. Il Consiglio di giugno si è impegnato a lavorare con i Paesi di origine e di transito, in collaborazione con l'Alto commissario dell'ONU per i rifugiati e l'Organizzazione internazionale per la migrazione. Questa prospettiva concordata ora necessita di una attuazione puntuale. Due degli impegni previsti hanno scadenza questo autunno: il primo è la presentazione da parte della Commissione e dell'alto rappresentante Borrell, in collaborazione con gli Stati membri, di piani di azione per i Paesi di origine e transito prioritari. Questi piani devono includere obiettivi, misure di sostegno, tempistiche precise. Il secondo è la presentazione di un rapporto al Consiglio sul miglior utilizzo possibile di almeno il 10 per cento dei fondi dello strumento di vicinato, sviluppo e cooperazione internazionale. Quest'estate l'Italia ha continuato a far fronte agli obblighi internazionali di salvataggio in mare e di garanzia di protezione internazionale agli aventi diritto. Lo abbiamo fatto con umanità, per difendere i valori europei della solidarietà e dell'accoglienza. però essenziale che a questo Consiglio la Commissione presenti piani di azione chiari, adeguatamente finanziati e rivolti con pari priorità con pari priorità a tutte le rotte del Mediterraneo, compresa quella meridionale. A questi piani poi andrà data una rapida attuazione. L'Unione europea deve inoltre prestare attenzione alla specificità delle frontiere marittime e all'effettiva stabilità politica della Libia e della Tunisia. Intendo proporre che la Commissione europea aggiorni i Capi di Stato e di Governo in ciascun Consiglio europeo sul grado di attuazione e di avanzamento degli impegni assunti. Solo in questo modo potremo rendere conto ai nostri Parlamenti e soprattutto ai nostri cittadini dei progressi compiuti a livello europeo e di quello che ancora resta da fare. Il Consiglio europeo discuterà anche di commercio internazionale. Dall'inizio di quest'anno abbiamo assistito a una ripresa robusta degli scambi tra Paesi. È un'ottima notizia, visto che il peso delle esportazioni nell'economia italiana è aumentato. Il valore totale dei beni esportati nel secondo trimestre di quest'anno era del 5 per cento che nello stesso periodo di due anni fa, prima della pandemia, quindi in sostanza la crescita delle esportazioni ha ora superato la crescita che avveniva prima della pandemia.

da interruzioni nelle catene di fornitura. La difficoltà nel reperire materie prime e componenti, unita a rallentamenti nei processi di trasporto e consegna, hanno contribuito ovunque ad un aumento del tasso di inflazione. Un tema fondamentale per la politica commerciale europea è quello del contrasto al protezionismo: dobbiamo migliorare i meccanismi multilaterali esistenti basati sulle regole e incoraggiarne l'utilizzo ampio e condiviso. Per quanto riguarda la riforma dell'Organizzazione mondiale del commercio, ci auguriamo che la dodicesima conferenza ministeriale di fine novembre abbia successo che si superino le criticità nei negoziati sui sussidi alla pesca e sulla politica commerciale sanitaria *post* Covid-19. Infine, il Consiglio europeo discuterà di relazioni esterne. Il 30 e 31 ottobre si terrà a Roma il vertice del G20 che concluderà l'anno della Presidenza italiana. La scorsa settimana abbiamo tenuto una riunione straordinaria del G20 sull'Afghanistan, in cui ci siamo concentrati sugli aiuti umanitari, sulla lotta al terrorismo e sulla mobilità. A Roma ci occuperemo principalmente dei temi della Presidenza italiana, dalla lotta al cambiamento climatico, alla pandemia, al sostegno della ripresa globale. In particolare, anticiperemo alcune delle negoziazioni che si terranno durante la COP26 di Glasgow, per la quale l'Italia è in partenariato con il Regno Unito. Come sapete, infatti, l'Italia e il Regno Unito copresiedono la Conferenza di Glasgow. L'Unione europea si è posta obiettivi ambiziosi, che includono la riduzione delle emissioni di gas climalteranti del 55 per cento rispetto ai livelli del 1990

Come sapete, l'Unione europea è responsabile di appena l'8 per cento delle emissioni globali, pertanto senza il coinvolgimento delle maggiori economie mondiali non potremo rispettare gli accordi di Parigi e contenere il riscaldamento globale entro un grado e mezzo. I Paesi del G20 nel loro complesso producono circa tre quarti del totale mondiale delle emissioni; la crisi climatica può dunque essere gestita solo se tutti i principali attori globali decidono di agire in modo incisivo, coordinato e simultaneo. In tutti questi ambiti l'Italia intende muoversi con convinzione per tutelare l'interesse dei cittadini italiani e di quelli europei. L'appoggio del Parlamento - il vostro appoggio - è decisivo perché la nostra azione possa essere davvero efficace. Vi ringrazio per le osservazioni che farete e per la pazienza con cui mi avete ascoltato.

Mi permetterà allora di allargare il ragionamento che lei ha svolto sui contenuti oggetto del dibattito dei prossimi giorni con alcune considerazioni più ampie e più politiche, meno legate ai singoli temi,

Lo farà in una cornice geopolitica profondamente diversa da quella di solo qualche mese fa, ma anche in una cornice europea profondamente diversa. lei sa meglio di me che il cambiamento di Governo in Germania è un altro fatto rilevante, un altro tornante della storia; dopo sedici anni di governo Merkel, si apre la formula del Governo Scholz con il cosiddetto semaforo, questa inedita alleanza che per la prima volta governerà Berlino. La Francia è dentro una campagna elettorale come sempre complicata. La Francia infatti talvolta ci prende in giro per l'imprevedibilità della nostra politica, ma non dimentichiamo che esattamente cinque anni fa, nell'ottobre del 2016, quando mancavano gli stessi mesi che mancano oggi alle elezioni presidenziali francesi del 2017, tutti davano per scontato un confronto tra Hollande e Sarkozy. A dicembre tutti davano scontato un confronto tra Valls e Fillon; è finita con Macron contro Le Pen. Vedremo che cosa accadrà adesso. E poi, signor Presidente, glielo dico in modo poco diplomatico; lei che è maestro di buona politica e diplomazia saprà prenderlo in positivo. Ai colleghi polacchi, ungheresi e sloveni farei capire una cosa molto semplice, se è possibile: va bene lamentarsi dell'Europa, ma se si sentono così a disagio con i valori europei, rinuncino ai soldi europei con i quali hanno salvato le loro barcollanti economie. Sentirsi infatti prendere in giro da Paesi come la Polonia, l'Ungheria e la Slovenia, o meglio dalle *leadership* di questi Paesi, fa venire un dubbio. Diciamolo con chiarezza ai polacchi: se vogliono stare in Europa, grazie alla quale sono tornati a crescere, inizino a rispettare i valori fondamentali perché l'Unione europea non è un bancomat. Sulle considerazioni che invece lei, signor Presidente, ha esposto, non soltanto le confermo l'appoggio e il sostegno di Italia Viva, ma le dico che siamo profondamente orgogliosi del lavoro che il Governo ha fatto, ad esempio, sulla vaccinazione. Aver cambiato linea, stile e passo tra Arcuri e Figliuolo, permette oggi a lei, al suo Governo e al nostro Paese di essere il modello non solo in Europa, come Anthony Fauci ha recentemente ricordato. Contemporaneamente dobbiamo dire che il nostro Governo sta svolgendo una funzione significativa anche nell'affrontare il tema del *climate change* e della sostenibilità, come lei ha ricordato, in una dimensione meno ideologica di quella che altri Paesi vorrebbero, anche perché poi, come sappiamo, in Europa sono tutti bravi a fare i documenti e poi sono i primi a mantenere gli interessi nazionali senza una visione unitaria e forte. prima di arrivare alle considerazioni che riguardano più specificamente la transizione digitale, un passaggio sull'immigrazione. Parlo senza alcuna polemica nei confronti dei colleghi del primo partito di opposizione di questa Assemblea, vale a dire Fratelli d'Italia; anzi essendo una maggioranza molto ampia, va garantito e e rispettato profondamente il lavoro delle opposizioni e della principale forza di opposizione. Sul tema dell'immigrazione, come il Presidente del Consiglio ha chiarito bene, c'è un punto fondamentale: o si cambia l'Accordo di Dublino o non si cambia tale Accordo, o o ci si fa carico in un momento come questo di cambiare quelle regole che dal 2003 permettono ai singoli Paesi di disinteressarsi della questione migratoria o non si va da nessuna parte. Mi rivolgo a Fratelli d'Italia perché sono guidati da una importante e significativa *leader* politica nazionale che guida anche il partito europeo nel quale è più forte l'avversione a tutti i tentativi di cambiare l'accordo di Dublino. Dunque se vogliamo fare l'interesse del nostro Paese, forse dobbiamo guardare un pochino di più a Lampedusa e un po' meno a Visegrad. Detto questo, signora Presidente, purtroppo l'Europa vive questa stagione nel momento più difficile. Javier Cercas, un grandissimo scrittore catalano e, come dice lui, un grandissimo scrittore europeo, ha detto parole meravigliose affermando che il problema in Italia e in Europa oggi non è il fascismo. il problema in Italia e in Europa oggi non è il fascismo. Il problema in Italia e in Europa è il nazional-populismo e l'Europa è l'unica forza politica e geopolitica che può affrontare certe sfide. Pensate soltanto alle sfide fondamentali di cui parlava il Presidente del Consiglio sulla transizione digitale. Ci rendiamo conto che siamo un gigante dai piedi d'argilla senza una strategia europea e ben vengano gli sforzi, molto apprezzati, del ministro Colao in questa direzione. Non dimentichiamo però che la partita oggi la stanno giocando gli americani contro i cinesi in Champions league e noi siamo in Lega pro. Questa sfida porta alcune intelligenze italiane, ad esempio, a condurre il loro valore fuori dai confini del nostro Paese. Lo dico in particolar modo guardando due autorevoli esponenti del mondo accademico, come la ministra Messa e la ministra Bonetti. C'è una ragazza italiana di quarantuno del Sud, siciliana, che si chiama Anna Grassellino, che sta guidando il laboratorio per la svolta quantistica sul computer quantistico nel Fermilab di Chicago. Si chiama Fermilab e io ho avuto l'onore di visitarlo accompagnato dal collega senatore, professore e premio Nobel Rubbia. Questa ragazza è costretta a vincere la sfida contro i cinesi, ma in quel laboratorio non vedono lo sforzo europeo, perché l'Europa, come ha detto il Presidente del Consiglio (e noi siamo convintamente dalla sua parte), non sta giocando la partita che potrebbe giocare. Molto di quel talento, formato nelle università italiane, molto di quel talento, che è fondamentale nella scommessa sulla sfida del futuro, oggi è lontano da noi. Signor Presidente, lei ha un compito straordinario. Lei ha salvato l'euro; tutti dicono che le è bastata una parola, ma lei sa e noi sappiamo che non le è bastata una parola. Ha fatto un grande lavoro per salvare l'euro. In questi mesi, piaccia o non piaccia ai polemici, ha dato una grande mano a far ripartire il Paese e a salvare l'Italia. Oggi lei ha un compito in più, perché nel 2022 si inizia a discutere di Patto di stabilità e persino i nostri amici tedeschi sembrano mettere già i puntini sulle "i", perché nel 2022 prima o poi qualcuno dovrà pur affrontare il grande tema della crisi democratica, che non riguarda noi.

per i populisti e nell'autoritarismo illiberale di alcune che non sono più democrazie (o non lo sono mai state), si sta affermando in tutti i Paesi un modello di sviluppo molto più agevole da governare, ma profondamente contrario ai nostri valori. O l'Europa riesce a recuperare i propri valori e quindi a dare una visione, come Javier Cercas ha cercato di dire in quella straordinaria intervista a "La Stampa", o non va da nessuna parte ed è costretta a essere distrutta dallo scontro tra America e Cina. Il presidente del Consiglio Draghi si trova in una fase in cui, per la sua forza, per la sua autorevolezza e per la sua esperienza, è, forse suo malgrado, il punto di riferimento di un'Unione europea che non ha più il *leader* degli ultimi sedici anni. Henry Kissinger diceva: qual è il numero di telefono dell'Europa? Negli ultimi sedici anni il numero di telefono dell'Europa è stato il cellulare di Angela Merkel; nei prossimi mesi il numero di telefono dell'Europa ha un prefisso italiano. Io penso che dovremmo fare tutti uno sforzo per elevarci rispetto alle politicucce, anche perché sennò, caro Presidente, va a finire come quella vicenda degli ultimi mesi, secondo me la più divertente e la più tragicomica letta sui giornali (non so se l'avete vista). A un certo punto, in una campagna turca, un signore cinquantenne cinquantenne è stato smarrito e non lo si trovava più; pare che fosse totalmente ubriaco. Tutti gli amici si sono messi a cercarlo e tutti intorno hanno iniziato a cercarlo; si sono messi a cercare questo ubriaco che si era perso e a questo gruppo che lo stava cercando si è unito anche lo stesso ubriaco, che se n'è accorto soltanto quando hanno chiamato il suo nome. Ecco, l'Europa rischia di finire così; è ciò di cui abbiamo bisogno, ma talvolta dimentichiamo che siamo noi quelli che stiamo cercando. Buon lavoro, signor Presidente.

Presidente, la gestione Europea dei flussi, che lei stesso ha definito direi quasi fallimentare, dicendo poco fa che l'Europa deve impegnarsi di più,

del presidente Renzi, ribadita anche con qualche spunto di critica nei confronti per esempio della Polonia. Vorrei dire due cose sulla Polonia, perfettamente integrata nella nostra idea di Europa, dove convivono popoli diversi e culture lontane, storie e tragedie, confronti che ci rendono parte di uno stesso destino di unità. Non posso ad esempio non pensare all'inno polacco, senatore Renzi, dove si parla di libertà, di indipendenza e anche esplicitamente di Italia. Fu scritto, senatore Renzi, proprio in Italia e proprio a Reggio Emilia, dove pochi mesi prima era stato ideato il nostro tricolore. Le parole dell'inno polacco - fareste bene a saperlo, colleghi, perché può essere utile - non sono troppo diverse da quelle del nostro inno, che infatti ricambia la cortesia citando il sangue polacco, come sangue di un popolo all'epoca, come noi, era schiacciato dalla stessa oppressione e dalla stessa tirannide. Non siamo quindi popoli uguali, ma popoli fratelli e per ogni Nazione europea potremmo raccontare dei legami che ci uniscono e che non sono legami

Signor presidente Draghi, 12 Nazioni hanno chiesto la possibilità e l'aiuto per costruire un muro, per impedire l'arrivo di migranti irregolari (semplicemente per questo), affermando che le barriere fisiche sembrano essere un'efficace misura di protezione, che serve gli interessi dell'intera Unione europea e non solo dei Paesi membri. La lettera è firmata da 12 Nazioni dell'Est Europa, che conoscono bene cosa voglia dire avere un muro in casa, che impedisce la circolazione e la libertà. Sono Nazioni che ricordano bene che, fino a trenta anni fa, esisteva un muro a Berlino, un muro fisico e terribile per i tedeschi, ma per tutti gli europei dell'Est un simbolo oppressivo e letale dell'oppressione comunista, subita dalla fine della Seconda guerra mondiale fino a trent'anni fa. fa. Questa esigenza di sicurezza non può essere considerata egoismo o crudeltà, ma è la richiesta di aiuto, in risposta ad un'esigenza reale un'emergenza che riguarda tutta l'Europa. Lo diciamo da tempo: un problema comune ha bisogno di soluzioni comuni. Ci fa piacere che qualcuno abbia apprezzato la richiesta di aiuto proveniente dall'Est: la socialdemocratica Johansson, commissaria agli affari interni, ha affermato che questi Paesi hanno il diritto e la responsabilità di tutelare i loro confini. È una sinistra che ha dimostrato di essere «Se uno Stato ritiene che sia necessario costruire una recinzione, lo può fare e non ho nulla da obiettare» ha affermato il politico della sinistra europea. europea. È chiaro che questo non basta e l'Unione europea deve aiutare e contribuire alla difesa dei nostri confini: non basta riempire di soldi Erdoğan, ci vuole molto di più: deve esserci uno sforzo condiviso. Siamo o non siamo un'unione? Per risolvere i problemi, la prima cosa da fare è riconoscerli e non far finta che non esistano, perché l'immigrazione irregolare e incontrollata non arriva solo nell'Est europeo. In Italia, dal 1o gennaio al 15 ottobre 2021, sono sbarcati 49.235 migranti irregolari, praticamente il doppio rispetto allo stesso periodo del 2020 e sono sestuplicati rispetto al 2019, senza contare naturalmente quelli che attraversano la rotta balcanica, con gli sbarchi fantasma. Ovviamente non possiamo costruire un muro con la Libia, ma dobbiamo ragionare su un nuovo modo, finalmente efficace, di difendere i confini dell'Unione europea, terrestri o marittimi che siano, finanziando, come già proposto da Fratelli d'Italia, gli Stati da cui partono i migranti irregolari solo se bloccano realmente le partenze e non riempiendo di soldi chi lo promette soltanto. Oggi abbiamo l'occasione di costruire un'Europa che non sia solo regole burocratiche e un nome scritto in piccolo su una cartina geografica o su un cartello per i turisti ma unione reale tra popoli tra popoli diversi ma fratelli per storia e cultura. Non è facile e

C'è sempre stata la contestazione sui tempi. *(Commenti).* Ha dato un minuto in più all'altro. Mi rifiuto di fare il Presidente dell'orologio.

Signor Presidente del Consiglio, Governo tutto, care colleghe e cari colleghi, è stato un intervento ricco di spunti e di grandi sfide che lei, signor Presidente del Consiglio, del Consiglio, ha posto alla nostra attenzione. Ci ha parlato di un'Europa che deve essere unita più che mai e che sicuramente da un anno e mezzo a questa parte - ormai anche qualcosa di più si è riscoperta unita. Un'Europa che deve essere capace di collaborare, cooperare e soprattutto costruire delle strategie comuni e condivise per essere sempre più forte.

ma abbiamo dimostrato, sia nell'occasione della comparsa del coronavirus nel nostro Paese e poi via via affrontando tutte le fasi in maniera

tuttavia, a volte la memoria è corta e, quindi, fa piacere anche ciò che lei, Presidente, ha ricordato. Mi riferisco all'impegno di tutto il sistema sanitario, al quale anche il Partito Democratico rivolge tutti i ringraziamenti del caso, sia per la prima parte della gestione della pandemia, sia per la seconda parte relativa alla gestione della vaccinazione, che ci vede adesso non soltanto in Europa, ma nel mondo. Anche noi ringraziamo tutto il sistema sanitario e diciamo che, grazie a tutto questo lavoro, come già lei ha ricordato, rispetto all'anno scorso in cui temevamo, come poi è stato, di non poter fare un Natale in sicurezza e in tranquillità, adesso invece viviamo un'altra situazione di apertura. Viviamo una situazione in cui le nostre scuole stanno funzionando, i nostri studenti sono in presenza; riaprono le attività; hanno riaperto hanno riaperto i luoghi della cultura e, come ha detto lei, i luoghi della società, ma direi della socialità. Credo che ciò sia un obiettivo che il Paese si era posto e che è stato raggiunto e di questo dobbiamo essere assolutamente orgogliosi. In Europa abbiamo dato un grande esempio di come l'Italia può lavorare. La ringrazio per aver fatto riferimento a

come Partito Democratico che il Governo batta sempre su quel punto e lo faccia non soltanto in Italia ricordando a tutti che questa è la strada, ma anche in Europa. È indubbio che si debba intervenire investendo in ricerca e scienza. Sappiamo quanto, purtroppo, gli investimenti in questi campi non sempre siano stati all'altezza dei nomi, dei cervelli che abbiamo in questo Paese. Tuttavia, questo anno e mezzo ci ha insegnato che proprio lì dobbiamo investire perché altrimenti non avremo risorse importanti come il vaccino e tante altre che ci hanno aiutato e stanno aiutando a uscire da questa gravissima

climatica sono tra le più importanti. Noi siamo con lei, siamo con il Governo nel dare tutto l'appoggio possibile al Paese attraverso le risorse che anche dall'Europa arriveranno, perché anche in questa pandemia ci siamo accorti di quanto sia primaria e fondamentale la digitalizzazione completa del sistema Paese, che è un circolo adesso forse vizioso, ma che speriamo di trasformare in virtuoso in modo tale che davvero tutta l'Italia possa crescere: dalla pubblica amministrazione alle aziende,

Tutti i costi da sostenere per accompagnare la transizione devono avere in mente l'uguaglianza, e questo è un aspetto che al Partito Democratico sta particolarmente a cuore.

*(Misto-+Eu-Az)*. Signor Presidente del Consiglio, non ripeterò quello che lei ha già detto, che in buona sostanza condivido.

a forza di tirare in lungo e in largo, non solo non facciamo passi in avanti, ma consentiamo a questi Paesi di fare passi indietro.

dell'Unione europea in quanto tale. Quindi, altro che andare avanti! Stiamo cercando o, almeno, alcuni tentano di avere e imporre un'altra visione d'Europa.

per il semplice motivo che, tra gli otto temi sottoposti al dibattito, manca quello per me più importante, cioè quello della questione istituzionale. Io resto convinta che, se non riusciamo a mettere nel cassetto il voto all'unanimità nel Consiglio dei Capi di Stato e di Governo, non andremo da nessuna parte, né sui migranti né, con buona pace di Macron, su l'*Europe de la santé*. L'*Europe de la santé*, con i trattati attuali, non si può fare. Non si fa, è semplice. Quindi, il punto essenziale di tutto questo circo che dura da più di un anno, in cui parlano i cittadini e chiacchierano di tutto e di più, alla fine è la modifica dei trattati, il superamento del voto all'unanimità del Consiglio e la capacità propositiva del Parlamento europeo. Queste sono, secondo me, le questioni essenziali. Ovviamente discuterete di molte questioni. Una delle cose che dico da quando ero ragazza è che non conosco organizzazioni più opache dei vertici europei. Non c'è mai neanche, salvo per qualche spiffero di stampa, l'ordine del giorno dei lavori. Non c'è, però lo direte dopo, ognuno in conferenza stampa e avendo ognuno vinto chissà quale battaglia straordinaria. Quindi, io le volevo dare alcuni suggerimenti. Punto uno: Polonia, Ungheria e Slovenia, perché questo virus o si stoppa subito oppure rischia di dilagare. Tanto l'Europa c'è e, quindi, possiamo anche permetterci di violarne i trattati. Tanto l'Europa sta lì; quando ci serve la usiamo, quando non ci serve non la usiamo. L'altro punto, che nei corridoi, ma io spero persino in plenaria, vorrei ricordare, prima che passi nel dimenticatoio della nostra memoria breve, è l'Afghanistan.

una mappa per capire benissimo gli interessi, cinesi in particolare, sul territorio dell'Afghanistan.

Non si sa) e i talebani, di cui si sa meno ancora: certo, c'era Baradar, lo abbiamo visto, ma chi altro sedeva dall'altra parte del tavolo? E il documento finale striminzito, di quattro pagine, non solo non accenna per niente alla questione dei diritti umani, ma ma si focalizza sulla lotta al terrorismo. Ora, è ben strano che i Servizi di *intelligence* della NATO, degli Stati Uniti o di quello che volete e la nostra presenza sul terreno non abbiano visto crescere, radicarsi ed essere operativo il cosiddetto ISIS-K. ISIS-K. È veramente strano, eppure, evidentemente, era così ben radicato e così ben organizzato che, a due giorni dalla presa dell'aeroporto di Kabul,

Tanto è vero che persino gli americani sono stati costretti a dire che i talebani, chiunque essi siano, non stanno rispettando i patti; non solo non li rispettano, ma i più grandi signori della guerra sulle liste nere dell'FBI o delle Nazioni Unite sono al Governo,

che ha senso per ora a livello internazionale: l'istituzione di un *rapporteur* speciale sull'Afghanistan, che ci aiuti a non spegnere proprio tutte le luci

Guardate, è l'unica iniziativa che è stata assunta - e mi piace esserne stata parte fin dall'inizio - per non spegnere le luci, che già si sono spente, a parte qualche giornalista coraggioso che *in loco*, finché potrà

«abbiamo bisogno di un'Unione europea forte ed efficace, un'Unione europea che sia *leader* globale nella transizione verso uno sviluppo sostenibile, climaticamente neutrale e trainato dal digitale. Occorre un'Unione europea nella quale ci possiamo tutti identificare, certi di aver fatto tutto il possibile a beneficio delle generazioni future. Insieme possiamo raggiungere quest'obiettivo». Non sono parole mie, presidente Draghi, ma del presidente Sergio Mattarella, che le indirizzava ai cittadini dell'Unione in occasione della Giornata dell'Europa, il 9 maggio scorso, facendoci riscoprire l'importanza e la forza di un'Europa unita e solidale; quella che sospende il Patto di stabilità, che rivede le regole per fronteggiare unita il flagello della pandemia, che decide di governare insieme le conseguenze economiche, con un programma di investimenti finanziato per la prima volta con un debito comune. Vorrei soffermarmi su un punto, che ritengo fondamentale e che abbraccia ogni argomento, dall'immigrazione, all'energia, alla digitalizzazione, al tema del Covid-19: il ruolo centrale della valorizzazione della nostra materia prima imprescindibile, il capitale umano. *(Applausi)*. Il capitale umano svolgerà un ruolo fondamentale per uscire dal tunnel. Tutto ciò che è cultura, formazione, creatività e ricerca sarà elemento imprescindibile per il rilancio. Che bello, presidente Draghi, sentirle dire della necessità e della volontà di investire in scienza e ricerca. Ecco il ruolo delle istituzioni, che devono diventare il pilastro a sostegno del nostro sviluppo e della nostra crescita. E che bello, presidente Draghi, sentirle dire che senza Stato le transizioni non avverranno. Ogni punto sottolineato da lei oggi è da noi condiviso e troverà in questo Parlamento lavoro per migliorare e creare le condizioni di condivisione con i cittadini da lei auspicate. Ci sono le famose risorse del Next generation EU, affidate per fortuna alla competenza e alla sua riconosciuta autorevolezza, presidente Draghi, perché sarà lei a doverle investire, come l'Europa ci chiede, per farne il motore della ripresa e dello sviluppo del Paese. E noi saremo al suo fianco, al lavoro, per per portarle istanze e necessità, per favorire, attraverso corretta informazione e condivisione, quell'opera di riconversione e quella transizione necessaria per portare l'Italia al centro dell'Europa e - perché no?- al centro del mondo. Che bello sentirle dire, presidente Draghi, che la transizione non deve spaventare, ma deve diventare l'opportunità per creare e aumentare posti di lavoro; qua ritorna la necessità di investire enormemente sulla formazione per governare l'innovazione. Sul tema dell'energia, premesso che condividiamo totalmente le scelte e gli obiettivi dell'Unione europea sul pacchetto Fit for 55 e le emissioni zero, questo però non deve avvenire violentando il nostro sistema produttivo, con conseguenze sociali di difficile valutazione. Su questo ci siamo confrontati col vice ministro Picchetto Fratin proprio l'altra sera. I costi della transizione non devono ricadere sui cittadini e sappiamo che il Governo sta lavorando per questo, intervenendo per rafforzare i dati economici in miglioramento e recuperare i ritardi senza gravare su imprese e famiglie, perché gli investimenti pubblici siano veramente funzionali al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibili individuati dall'Agenda 2030. Mi raccomando, Presidente, e mi perdoni la divagazione sul tema, ma stamattina c'era molto fermento per la notizia della proroga del superbonus al 110 per cento alle sole unità condominiali: gli ecobonus vanno mantenuti, prorogati ed estesi. Ci sono ben altri provvedimenti che potranno essere tagliati. Dobbiamo perseguire la sostenibilità a tutto tondo, dobbiamo saper coniugare sostenibilità ambientale, sostenibilità economica e sostenibilità sociale, pena l'impoverimento e il blocco del sistema Paese. Per creare le condizioni di equilibrio tra tutela ambientale e mantenimento del benessere sociale è necessario puntare sull'innovazione tecnologica. Quindi, basta alla paura degli impianti nuovi, basta alla paura dell'innovazione; solo attraverso l'innovazione e il governo dell'innovazione attraverso la formazione noi potremo fare un salto grandissimo. E che bello, presidente Draghi, sentirla parlare di alleanza pubblico-privato per accompagnare le riconversioni, le *reskill* aziendali e culturali che vanno assistite e sostenute, attraverso riforme efficaci, come questo Governo sta facendo, di semplificazione, con il ministro Brunetta, e di digitalizzazione della pubblica amministrazione. il Paese che ha fatto dell'ingegno la propria materia prima. È un Paese la cui ossatura è formata dalle piccole e medie industrie, dal manifatturiero e dalle attività produttive. È un Paese dove la libera iniziativa produce capolavori, ma è anche un Paese dove la capacità di creare prodotto e lavoro viene frenata, messa in difficoltà e osteggiata da un sistema burocratico complesso, ingiustificato e ormai pletorico per un Paese che non solo deve dimostrare resilienza - questo l'ha detto lei, presidente Draghi,

infatti accelerare il processo di installazione delle rinnovabili per sganciarsi quanto prima dal costo del gas. Per fare questo processo - ritorno a bomba - servono semplificazioni, certezze normative e regole per garantire l'efficienza della pubblica amministrazione. Mi sembra che siamo sulla strada giusta. Forza Italia è a favore delle nuove tecnologie sostenibili che ci possono rendere autosufficienti sul versante dell'approvvigionamento energetico. E respinge in modo netto qualsiasi posizione ideologica che nasce da una totale mancanza di informazione e fa solo danni. Anche sul nucleare pulito, informiamoci sulla differenza tra

I pesanti aumenti colpiscono le nostre attività economiche, che vedono ulteriormente indebolita la propria competitività sui mercati europei e internazionali, che da anni beneficiano di prezzi delle energie inferiori, e colpiscono le famiglie, sia direttamente in bolletta sia per gli inevitabili aumenti dei prezzi dei beni di consumo per effetto degli aumenti dei costi di produzione. Il rischio che parta l'inflazione è altissimo. Le cause: per il 20 per cento l'aumento dei prezzi della CO₂ e, dunque, l'effetto diretto degli obiettivi della decarbonizzazione spinta; il restante 80 per cento dipende dall'aumento dei costi del gas naturale. Qui le regole del mercato e una tempesta perfetta sono stati deflagranti. Vi è l'impennata della domanda mondiale di energia a seguito della ripresa economica *post* Covid; vi sono le strozzature nell'offerta delle forniture di gas a partire dalla Russia; vi è stata la bonaccia nel Mare del Nord, che ha lasciato in panne gli impianti eolici. E così nell'ultimo anno per il gas abbiamo registrato aumenti del 600 per cento. Molti, superficialmente, hanno individuato proprio nel gas il colpevole del caro energie e, dunque, giù a demonizzarlo per escluderlo. Io invece ritengo che l'impennata della sua domanda è anch'essa legata alla transizione, per le conversioni delle centrali a carbone, e questo avviene anche in Cina; per la decarbonizzazione delle acciaierie; per la maggior produzione di alluminio che guarda avanti, dalla bauxite sta producendo molto più alluminio, che serve a loro e a noi per la transizione ecologica. Pechino sta facendo incetta di materia prima e di prodotti energetici anche lo *shale* *gas* USA ormai va in Cina - mentre l'Italia e l'Europa rischiano di rimanere a secco. Di più: Pechino, proprio perché ora vuole smarcarsi dal caro gas, continua a costruire nuove centrali a carbone e massimizza la produzione di questo prodotto presso le proprie miniere. A loro interessa non inquinare, ma produrre a bassi costi. *(Applausi)*. Insomma, il gas naturale, da molti ripudiato, prepotentemente sta esercitando il suo ruolo strategico di fonte energetica di accompagnamento alla transizione ecologica. Siamo a una situazione allarmante: ormai il costo dell'energia è fuori controllo e non è più compatibile con le attività delle imprese *gas intensive*, tanto da determinare la sospensione delle attività e delle produzioni.

Come darle torto? Il prezzo unico nazionale è da giorni sopra i 220-230 euro a megawattora, un livello molto superiore a quelli che hanno determinato l'aumento di fine settembre. Vengo alle ricette europee sul caro energia. le misure immediate *ad hoc* per la tutela di consumatori e imprese vulnerabili. Ma sulle misure a medio termine, *premier* Draghi, siamo sicuri che, come si vuol procedere, la transizione verde all'energia pulita deve essere accelerata perché considerata il modo migliore per uscire da questo dramma e per scongiurare altri *shock* in futuro? Siamo sicuri che un sistema energetico caratterizzato da tante rinnovabili sia l'unica soluzione e si traduca in prezzi dell'energia all'ingrosso più convenienti? Siamo sicuri di fermare gli investimenti per il gas e dirottarli esclusivamente sulle rinnovabili pensando, magari senza il nucleare, che queste possano rispondere alla domanda di energia globale, crescente nonostante i sacrosanti interventi di efficientamento energetico? Non scherziamo, con il solo fotovoltaico e l'eolico non andiamo da nessuna parte. *(Applausi)*. Non si tratta solo di tutelare il paesaggio e le aree agricole coltivabili. Il grande problema è che queste fonti rinnovabili ammesso e non concesso che riusciremo a recuperare i forti ritardi in nuova capacità installativa - non sono programmabili e producono solo quando ci sono vento e sole. È molto semplice e persino banale. I sistemi di accumulo sono lungi dall'essere tecnologicamente pronti, sviluppati e distribuiti sul territorio. Inoltre, occorre considerare il necessario e costoso sviluppo delle reti di trasmissione, di distribuzione e delle infrastrutture di ricarica elettrica. Le ricette dell'Europa francamente non mi convincono. Presidente Draghi, secondo la Lega la transizione ecologica deve essere graduale e pragmatica, senza spinte ideologiche alla decarbonizzazione che rischiano di mettere in ginocchio le nostre imprese. Attenzione ai facili entusiasmi - vere e proprie ubriacature per il solo rinnovabili - per il no immediato ai fossili (stile Greta Thunberg) per il solo idrogeno verde, per il solo mobilità elettrica e per l'assurdo *plastic free.* La transizione ecologica deve essere soprattutto condivisa, come lei ha detto poc'anzi, presidente Draghi. Non esiste che l'Europa, responsabile del solo 8-9 per cento di emissioni di CO2, faccia la prima della classe ed essere *carbon neutral* al 2050 e che altri Paesi (a partire dalla Cina che, con il 28 per cento di CO2 è il più grande inquinatore del pianeta) non si assumano i medesimi impegni. La transizione ecologica deve assicurare il sacrosanto principio della neutralità tecnologica, perché tutte le tecnologie che contribuiscono a decarbonizzare devono essere impiegate e - piaccia o no - il gas naturale non è morto. Occorre avere l'umiltà di ammettere che le fonti energetiche per decarbonizzare durante la transizione ecologica sono il gas naturale a bassa emissione di carbonio e il nucleare a zero emissioni. all'energia atomica pulita di quarta generazione, ricordo che la Francia ha 56 centrali nucleari e che il Governo britannico, che ha al centro della propria strategia la transizione energetica, punta a inserire l'energia atomica per decarbonizzare al 2050. Occorre dunque fare investimenti per rispondere adeguatamente alla domanda del gas, che resterà alta nel tempo e serve per decarbonizzare. Presidente Draghi, lei che è un *premier* autorevole, quando, domani e venerdì, discuterà con gli altri Capi di Stato e di Governo, faccia valere in Europa il pragmatismo. Occorre ridurre la dipendenza energetica dell'Europa e la nostra italiana (per il 95 rispetto al gas, anche impiegando maggiormente le proprie risorse naturali e investire per diversificare le fonti di approvvigionamento per garantire la sicurezza del sistema energetico. Occorre negoziare con la Russia che fornisce il 50 per cento del gas all'Europa, anche per evitare amare sorprese nell'inverno che potrebbe essere rigido. Occorre definire regole comuni per la gestione della sicurezza degli approvvigionamenti del gas e per la regolamentazione degli stoccaggi e delle scorte. Nel pacchetto sulla finanza sostenibile, tra i criteri della tassonomia degli investimenti verdi, siamo d'accordo a eliminare petrolio e carbone. Ma occorre riconsiderare il ruolo di accompagnamento strategico del gas naturale nella transizione ecologica ed energetica, sia ai fini del contenimento dei costi dell'energia, sia per garantire stabilità, sicurezza e resilienza del sistema energetico. Ricordo che la Germania,

pensiamo seriamente a un riordino della disciplina degli oneri di sistema e delle altre voci in bolletta, come i costi di trasporto; nonché a valutare la possibilità di effettuare una misura di equità, come un prelievo temporaneo sugli *extra* profitti e sulle rendite inframarginali di cui diversi beneficiano in questa situazione. Mi permetto una riflessione sul Fit For 55. Il pacchetto formalizzato a luglio scorso dalla Commissione ha molte criticità. L'estensione del sistema EU ETS ad altri settori quali il trasporto marittimo su strada e l'edilizio - il che significa altre tasse - e, soprattutto, il bando dal 2035 delle auto a combustione interna con il solo modello elettrico scelto dall'industria automobilistica tedesca sono una follia. Questa previsione è un assurdo. *(Applausi)*. È una follia entrare a gamba tesa e cancellare le auto Euro 6 e 7 di ultima generazione, quelle alimentate con carburanti *low carbon*, quella a biometano, quelle ibride, capaci anch'esse di ridurre le emissioni della CO2, a vantaggio delle sole auto elettriche classificate falsamente come veicoli a emissioni zero. È un'ipocrisia misurare ancora le emissioni al tubo di scarico: l'elettrico inquina anch'esso nel suo ciclo di vita. Questo bando mina il principio della neutralità tecnologica; distrugge il comparto della meccanica italiana, la filiera dell'*automotive* e quella della raffinazione e inganna sulla tutela dell'ambiente. A proposito di impatto sociale, ricordo che Volkswagen,

*(M5S)*. Presidente Draghi, il Consiglio europeo a cui parteciperà è un'occasione importante per il nostro Paese perché, oltre che delle politiche di contrasto al Covid, si parlerà anche di trasformazione digitale e di prezzi dell'energia, tematiche prioritarie per il MoVimento 5 Stelle e per tutti gli italiani. Sappiamo tutti - Presidente - che, per colpa di scelte politiche miopi portate avanti negli ultimi venti-trent'anni, in Italia sono ancora pochi coloro che hanno una connessione Internet decente ed è ancora troppo bassa la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, così da abbattere i costi sia in bolletta, sia ambientali. Dove va ad agire il Piano nazionale di ripresa italiano? Principalmente nei seguenti ambiti: transizione digitale A differenza del passato, oggi oltre alla spinta ecologica del MoVimento 5 Stelle c'è un fattore in più: abbiamo i soldi per una rivoluzione verde e digitale, un'opportunità unica e straordinaria ottenuta dal suo predecessore Giuseppe Conte e che ora lei deve concretizzare, trasformando i soldi in cantieri e in opere completate entro la fine del 2026. Come le dissi il giorno del suo insediamento, signor Presidente, in questa innaturale maggioranza di Governo la fiducia sarà non incondizionata, ma ponderata sulle azioni che sta intraprendendo giorno per giorno e, per quanto ci dicano che va sempre tutto a gonfie vele, la realtà appare più nebulosa, soprattutto sul *recovery* italiano. Le informazioni che arrivano a questo Parlamento, Presidente, dal Governo sono ad oggi poche e frammentate. È sufficiente entrare nel sito Internet governativo dedicato al Piano di ripresa italiadomani.gov.it - per capire che c'è ancora poco, non si sa ancora bene chi fa cosa, come lo fa e quando lo fa; come non si conosce con certezza la distribuzione territoriale dei fondi. Eppure, Presidente, la legge di bilancio 2021 era stata chiara e prevedeva l'obbligo per il Governo entro il 30 giugno di ogni anno, a partire da quest'anno, il 2021, di approvare e trasmettere alle Camere una relazione indicante lo stato dell'arte sull'impiego dei fondi del Piano nazionale.

il Governo per molto meno: era sufficiente una conferenza stampa del suo predecessore fatta in piena pandemia per rassicurare gli italiani e spiegare loro le nuove norme anti-Covid per far urlare alla dittatura del DPCM e allo svilimento del Parlamento. Lo ricorderanno tutti in quest'Aula. con un Governo con un certo ritardo di qualche mese nell'informare il Parlamento su un tema importante come il *recovery* italiano, tutto tace. Capisco che il suo grande *curriculum* e la sua esperienza internazionale le abbiano consentito di avere uno scudo protettivo politico e mediatico, ma qui le chiediamo solo di rispettare gli impegni. quindi un paio di domande specifiche: le chiedo quando il Parlamento avrà tutte le doverose informazioni a disposizione e quando gli italiani potranno sapere quali e quanti soldi saranno impegnati sui loro territori e soprattutto chi li dovrà gestire, così almeno sapremo chi dovrà assumersi le dovute responsabilità in caso andasse male la gestione. Se da una parte sappiamo, Presidente, che il blasone del suo nome aiuta e può aiutare l'Italia nei decisivi tavoli europei; dall'altra parte, dobbiamo rammentarle che questo non può bastare, perché alla fine sono i risultati concreti che contano e che interessano ai cittadini. Ad oggi, signor l'unica cosa certa è che ci stiamo giocando il futuro delle prossime generazioni e non possiamo sbagliare. Siamo con lei, signor Presidente del Consiglio, e la sosteniamo quando si oppone a coloro che attaccano i poveri cercando di eliminare il reddito di cittadinanza. bene a non cedere alla loro opportunistica cattiveria di cancellarlo. Sappiamo che togliere fondi alla parte più debole della società e dirottarli alle tante collaborazioni esistenti fa guadagnare soldi e potere ai politici che lo fanno. modo siamo con lei, signor Presidente del Consiglio, e la sosteniamo quando tira dritto con quei soggetti che dovrebbero solo vergognarsi quando attaccano la gestione dell'ordine pubblico da parte della ministra Lamorgese. Non sto difendendo l'operato della sua Ministra, conscio degli errori commessi, ma sto parlando del contorsionismo di Giorgia Meloni e di Fratelli d'Italia, che urlano contro una Ministra per non avere subito arrestato un delinquente che, alla prova dei fatti, politicamente è sempre andato a braccetto con loro, in un capovolgimento della realtà che farebbe ridere se non ci fosse di mezzo alla violenza. Siamo con lei, signor Presidente del Consiglio, quando difende il superbonus al 110 per cento prorogandolo al 2023 per i condomini. Non siamo con lei quando da questa proroga rimangono escluse le abitazioni unifamiliari, come sta accadendo. *(Applausi)*. Vogliamo capire che l'importante ripresa economica in atto è dovuta soprattutto al *boom* del settore delle costruzioni conseguente conseguente al superbonus? Si tratta della misura più importante e impattante per una crescita felice attraverso la transizione a un'economia ecologica: limitarla è un grosso errore a cui cercheremo di porre rimedio.

il costo delle bollette tanto aumentato. Questo è un altro tema che lei andrà ad affrontare in Europa e che dovrebbe forse anche affrontare con il ministro Cingolani, che - ci dispiace dirlo - a volte ci appare più innamorato

gli applausi di Confindustria. Cerchi gli applausi della gente normale; spieghi loro ciò che sta facendo oggi e che ha intenzione di fare domani. Parta dai dubbi e non dalle certezze. Si domandi come mai oggi ci sono più tensioni sociali rispetto al passato, quando non c'erano i vaccini e oggi c'è il crollo dei contagi.

che ha rinunciato all'intervento. Una volta tanto abbiamo qualche minuto in più per parlare noi europeisti, visto che in questo Paese sembra che i *media* in particolare vogliano dedicare più spazio a chi è contro l'Europa rispetto a coloro che non sputano nel piatto in cui mangiano. Noi siamo consci dell'importanza di questo Consiglio europeo e al riguardo abbiamo potuto visionare la documentazione fornita in modo ottimale congiuntamente dalla Camera dei deputati e dal Senato Repubblica. E invito E invito tutti, anche chi ci ascolta, a consultare le relative pagine molto fitte e molto bene informate. Al riguardo le dico che non ho proclami da leggere ma solo qualche considerazione da svolgere. La prima è che noi siamo

su «europeisti.org» per primi, a marzo, quando sono stati firmati i relativi trattati e parlato della Conferenza sulla nuova Europa, abbiamo impostato con gli amici del Movimento federalista

una propria architettura *open* *source* che possa far sì che il mercato europeo non sia solo un mercato delle licenze a disposizione degli americani, con tutto il rispetto per i nostri alleati. Abbiamo poi operato nell'ambito del commercio. Siamo contenti che la nuova amministrazione americana possa sbloccare l'operatività del

(CETA) e siamo particolarmente interessati a vedere gli sviluppi dell'azione dell'Unione europea nell'area indocinese con gli accordi con l'ASEAN. Tutto questo dimostra l'importanza, la rilevanza e la centralità dell'Unione europea nel panorama globale. Questo dovrebbe sfidare l'onestà intellettuale di tutti noi e, in particolare, di alcuni colleghi e comprendere quanto rilevante sia per l'Italia giocare in questo campo. Il nostro campo di gioco è quello europeo

potersi muovere nell'ambito di accordi che l'Unione europea prende per conto di 450 milioni di abitanti piuttosto che di 60. Lo sanno bene i nostri amici del Regno Unito che sono usciti e che incontrano una serie di difficoltà non solo logistiche, ma anche nella negoziazione dei trattati internazionali che sono ormai evidenti. Faccio una chiosa sugli amici del Regno Unito. Presidente Draghi, lei ha ricordato che noi siamo co-presidenti della COP26. L'Unione europea ha una sua integrità e una sua coerenza come - per esempio - l'attenzione ai temi ambientali. Gli amici inglesi di recente hanno rinunciato ad alcuni principi tecnici in tema di salvaguardia ambientale pur di concludere un accordo commerciale con l'Australia; un tema molto imbarazzante. confermare ancora una volta l'integrità, la coerenza, l'aspetto precipuo dell'azione dell'Unione europea di cui noi siamo molto fieri, e siamo molto contenti di farne parte. L'Unione Europea è un *soft power*. Abbiamo anche analizzato l'aspetto, e prossimamente, il 3 novembre, faremo un evento su di esso,

ora confermare altri due aspetti. Il primo: nell'integrità dell'azione dell'Unione europea e nell'interesse dell'Italia a farne parte, c'è la coerenza, oltre che con i propri principi democratici e la salvaguardia dell'ambiente, anche con

pubblicò "Lo spirito delle leggi", proprio teorizzando la separazione dei poteri, la Polonia sperimentava, con la Confederazione polacco-lituana, il principio del *liberum veto*, cioè il diritto di veto di ciascuno dei conti che rappresentavano le comunità polacca e lituana, che nel giro di pochi decenni ha portato alla dissoluzione di quella esperienza democratica. Potrebbe essere utile ricordare questo passaggio storico. Noi riteniamo la separazione dei poteri e la lezione di Montesquieu un'acquisizione della nostra civiltà e della nostra cultura su questo non possiamo venir meno. Credo che il Parlamento europeo faccia bene a ricordare alla Commissione il diritto da una parte e il dovere dall'altra di agire per far rispettare la *rule già ricordato che lei sarà il più europeo dei presenti al Consiglio europeo. Lo dico non solo per il fatto che il suo nome è scritto sulle banconote dell'euro che abbiamo in tasca, ma anche perché lei rappresenta una percentuale notevole di italiani residenti in Europa. Si tratta perlomeno di 3 milioni e mezzo di iscritti all'AIRE, ma in realtà il numero potrebbe anche

concludo con un tema meno aulico, ma molto coerente con il collegio e con la *constituency* che rappresento. Noi abbiamo fatto uno sforzo che è stato premiato, l'anno scorso, con l'approvazione di disposizioni di legge per il riconoscimento della ristorazione italiana all'estero, che rappresenta la vetrina del *made in Italy*, nonché la maggiore tutela contro l'*Italian sounding*. Abbiamo visto con piacere che il presidente Macron l'ha invitata in un ristorante francese per un vertice. Noi le chiediamo di rispondere in altrettanti termini, quando e dove lo potrà considerare utile, perché tantissimi ristoranti italiani all'estero, che sono gli ambasciatori del *made in Italy*, sarebbero fieri di ospitare un incontro istituzionale. Noi veniamo da un presenza all'Anuga, che è la maggiore fiera agroalimentare del mondo, in cui abbiamo pubblicamente presentato queste disposizioni di legge; stiamo aspettando da nove mesi il decreto di attuazione. Le chiediamo anche questa attenzione, come ex italiano all'estero e come rappresentante dei tanti italiani in Europa. Per favore andiamo avanti e, nel frattempo, buon lavoro e buon Consiglio europeo.

sul quale condivido molto di quanto da lei esposto nel suo intervento, presidente Draghi. È una questione con cui avremo a che fare ancora per molti mesi, con conseguenze economiche molto preoccupanti sia sul lato dell'inflazione, sia per il pericolo di un rallentamento o addirittura di un'interruzione della ripresa. Questa situazione ha coinvolto tutti gli Stati, anche quelli più nuclearisti, legati comunque alle stesse regole di formazione dei prezzi sui mercati internazionali. Il Governo ha già dato alcune risposte, intervenendo con sussidi sulle bollette. Ma una politica di sussidi non può essere la soluzione strutturale: è doverosa - per carità - ma non risolve il problema nel medio-lungo periodo. Solo con azioni strutturali sul mercato dell'energia in ambito europeo e nazionale il problema potrà essere risolto. La confusione alimentata dai *media* non ha poi aiutato a inquadrare fin da subito le reali cause. Si sono dovuti scomodare von der Leyen e Timmermans per fare chiarezza sull'argomento e ribadire che l'unica alternativa possibile sono le rinnovabili e l'efficienza energetica. *(Applausi)*. Si può non essere d'accordo, ma è la posizione europea, che condividiamo. E lo dimostra la tempesta perfetta in corso: un forte aumento dei prezzi del gas, che si è verificato in questi mesi per la combinazione di situazioni strutturali e congiunturali che potrebbero perdurare. Il sistema energetico nazionale e europeo, fortemente dipendente dal gas, pur disponendo di un sistema di infrastrutture diversificato, non ha potuto sottrarsi alle dinamiche degli aumenti di prezzo. Veniamo alle proposte. Qualcuno suggerisce di ritornare alle produzioni nazionali, e cioè di aumentare le trivellazioni sui suoli e nei mari italiani, per avere gas e petrolio a buon mercato. Ma questi gas e petroli sarebbero estratti da operatori privati e prezzati sempre e comunque sui mercati internazionali, rimanendo quindi legati alle attuali dinamiche di prezzo, che non controlliamo. *(Applausi)*. Dubito fortemente poi che tali operatori privati siano disponibili a effettuare nuovi e costosi investimenti senza avere certezza dei ritorni economici. il settore fossile è fortemente *cost intensive* e gli investimenti abbisognano di diversi anni prima di essere ammortizzati. Inoltre, il quadro politico nazionale, a seguito anche dei nostri *referendum*, si sta predisponendo a un forte giro di vite in senso energetica sostenibile delle aree idonee (PITESAI) che dispone un restringimento delle aree marine trivellabili e il divieto di nuovi pozzi di petrolio in terraferma, con forti limitazioni anche sul gas. Pertanto, nella sua recente comunicazione, la Commissione propone di sostenere imprese e consumatori, in particolare quelli in difficoltà, ma soprattutto di rafforzare la nostra indipendenza energetica tramite la transizione all'energia pulita: il modo migliore, secondo la Commissione, per scongiurare altri *shock* futuri. Per questo tale transizione deve essere accelerata, in linea anche con gli impegni internazionali su clima ed energia.

con totale assolutezza che non ci dovranno essere ulteriori investimenti in fonti fossili. Stop a nuovi investimenti in fonti fossili: lo dice l'Agenzia internazionale dell'energia.

capisce perfettamente. Prima lo facciamo, più risparmiamo e quindi più guadagniamo. Rinnovabili ed efficienza energetica hanno un ruolo chiave: il primo a dirlo fu Nicholas Stern, addirittura nel 2007, quattordici anni fa, ma da allora sono tantissimi gli studi autorevoli che ribaltano la narrativa dei costi maggiori rispetto ai benefici per la transizione e invece dimostrano che prima si fa

Quindi, sostenere le rinnovabili e investire su strumenti come le comunità energetiche e i superbonus al 110 per cento è la chiave per ridurre in modo strutturale i costi energetici e calmierare la crisi in atto. Significa passare a un modello rinnovabile, decentrato, efficiente e molto più resiliente e legato a dinamiche economiche non rischiose. I numeri già adesso lo dimostrano. Recentemente il Gestore dei servizi energetici (GSE) ha calcolato che le oltre 750.000 famiglie e utenze domestiche, che nel nostro Paese hanno già realizzato un impianto fotovoltaico o altro a fonte rinnovabile in autoconsumo, hanno evitato e scansato per un terzo l'aumento del costo dell'energia, perché in parte usano la loro energia autoprodotta. Vantaggi simili ci sono stati anche per le quasi 110.000 imprese, che ugualmente hanno realizzato un impianto a fonte rinnovabile, con cui si autoalimentano. A ciò si aggiungano naturalmente i risultati in termini di risparmio e di riduzione degli approvvigionamenti, conseguiti grazie agli interventi di efficientamento, spinti anche dal superbonus: fatti che dimostrano come questi interventi abbiano ridotto gli aumenti recenti. Quindi, implementare il modello dell'autoconsumo dell'energia rinnovabile sposta i risparmi e, quindi, i guadagni a favore dei cittadini, delle imprese e delle autorità locali. E questo si può fare attraverso la costituzione di comunità energetiche da loro stessi gestite. Crediamo poi sia di fondamentale importanza prorogare l'applicazione del superbonus anche agli immobili unifamiliari *(Applausi)*. Sono strumenti che vanno sostenuti anche per rafforzare la filiera tecnologica e produttiva nazionale e offrire al sistema economico un importante valore aggiunto, scongiurando il rischio di crisi. Presidente, colleghi, quelle che per motivi di tempo sono state solo accennate sono soluzioni reali, concrete e a portata di mano e abbracciano una visione che, se perseguita, porterà un miglioramento strutturale delle condizioni economiche, ambientali e sociali. Come MoVimento 5 Stelle facciamo appello alla sua responsabilità e a quella del Governo, affinché sui tavoli decisionali, europei e non, venga sostenuto e implementato un modello energetico rinnovabile, efficiente, decentrato e spinto verso l'elettrificazione dei consumi. Questo va fatto anche... *(Il microfono Signor Presidente, il Consiglio europeo convocato per il 21 e 22 ottobre tra i temi all'ordine del giorno avrà proprio il recente aumento dei prezzi dell'energia

Sono due mesi che gli italiani sono letteralmente terrorizzati dagli annunci degli aumenti folli dei prezzi dell'energia. Come nel gioco del lotto, si susseguono

soprattutto le famiglie, i lavoratori e le imprese, che sono già stremati da una pandemia cui questa maggioranza non ha saputo rispondere in modo efficace e con prontezza. atto a questo Governo, dopo l'iniziale e anche improvvido annuncio del ministro Cingolani, di aver cercato in qualche modo di trovare una soluzione.

il solito pannicello caldo, ovvero un rinvio. Va preso atto che questo spettro si aggira per l'Europa dall'inizio della stagione invernale. I prezzi dell'energia che determinano quelli di luce e gas pagati dai cittadini sono in forte I rincari sono destinati a salire, soprattutto se si verificassero interruzioni impreviste nelle forniture di gas o forti ondate di freddo, che chiaramente andrebbero a incrementare la domanda e di conseguenza anche i costi.

Questo agire incerto non consente di instaurare alcun tipo di fiducia nelle imprese che dovrebbero comunque investire capitali

immaginare, se in questa fase si trovano a fronteggiare un quadro economico così incerto, cosa potranno fare e come potranno organizzare la loro attività

Signor Presidente, è inutile sbandierare l'adeguamento del mercato energetico europeo alla norma per la tutela del consumatore debole se poi la stangata arriva nei mesi invernali, ma soprattutto senza alcun tipo di

È questo che chiedono i cittadini ed è ciò che Fratelli d'Italia chiede a lei di rappresentare in Europa. Bisogna fare chiarezza, una volta per tutte, sulla linea di politica energetica del nostro Paese e soprattutto sui *target* da raggiungere. Tuttavia, questo non va fatto mese per mese, ma anno per anno, a livello europeo ma anche a livello nazionale, perché non si possono prevedere misure di agevolazione per l'efficientamento energetico come il superbonus 110 e poi non prorogarne la durata o garantire una stabilizzazione di medio-lungo periodo. Non è pensabile attendere ogni anno la legge di bilancio per quanto riguarda le misure come il bonus energetico o lo sconto in fattura, che hanno rappresentato - nel bene e nel male - il vero volano dell'economia reale del nostro Paese, soprattutto per quanto riguarda l'edilizia.

ci ritroviamo qui oggi a svolgere una discussione in vista del prossimo Consiglio europeo che si terrà domani e venerdì, come è noto a tutti. Si tratta di un appuntamento divenuto ormai prassi del Parlamento, che permette a noi parlamentari di conoscere e comprendere meglio i temi all'ordine del giorno, di discuterne insieme e di provare a fornire al Governo atti di indirizzo che lo possano supportare nell'azione politica. In questo senso, il presente dibattito - e parlo anche del mio ruolo istituzionale di Presidente della Commissione affari europei del Senato - ha una valenza politica fondamentale, perché ci permette di entrare nelle dinamiche politiche del Consiglio europeo, di coglierne meglio il funzionamento nelle relazioni tra gli Stati. Con questo spirito ci siamo preparati per la seduta di oggi, con una risoluzione, che voteremo da qui a breve, a cui abbiamo lavorato nei giorni scorsi insieme al sottosegretario Amendola, che ringrazio per la sua disponibilità e sensibilità, e con il contributo di tutti i Gruppi che compongono la maggioranza di Governo: la risoluzione è stata sottoscritta da tutti. È stato un lavoro articolato, che ha permesso di raggiungere una sintesi, che è nel compendio dei vari punti della risoluzione sottoscritta. Naturalmente, ci siamo attenuti ai punti contenuti nell'agenda del Consiglio europeo: la lotta al Covid, il digitale, i fenomeni migratori nella loro dimensione esterna, così come richiesto dal nostro Governo. Abbiamo, poi, discusso anche di altri punti - magari ne stiamo discutendo anche qui oggi - che non sono formalmente all'ordine del giorno, ma che attraversano l'agenda politica di questi giorni. Mi riferisco, signor Presidente, al tema dello Stato di diritto e alla sua declinazione particolare - volendo usare un eufemismo - che viene fatta in Stati come Ungheria e Polonia. Ne abbiamo parlato qualche giorno fa anche con la vice presidente Jurova, alla quale abbiamo manifestato tutte le nostre più vive preoccupazioni. C'è il dialogo sullo Stato di diritto, una procedura informale che abbiamo avviato qualche anno fa proprio sotto la nostra Presidenza dell'Unione; c'è il tema della procedura dell'articolo 7 del Trattato; ci sono le procedure di infrazione. Con questi strumenti penso che l'Unione europea possa garantire il rispetto delle regole da parte di tutti gli Stati che ritengono di porsi al di sopra del diritto europeo, disconoscendo di fatto - come ha fatto di recente la Polonia - il principio della primazia del diritto europeo sugli Stati. Se ne discuterete al Consiglio europeo, signor Presidente, magari anche a margine dei lavori ufficiali, è importante che arrivi da parte dell'Italia, che è e deve essere a fianco delle istituzioni europee, la riaffermazione di uno dei principi fondamentali nella costruzione della Casa europea, che va difeso e confermato ove venga messo in discussione. questo *incipit*, mi riporto ai temi all'ordine del giorno. Signor Presidente, l'Italia sta faticosamente, ma sempre più decisamente, risalendo la china dopo il drammatico periodo della pandemia, con un'azione di Governo vigorosa e incisiva, che il suo Governo, il nostro Governo, presidente Draghi, sta portando avanti in questi mesi e che ha già permesso di recuperare molti posti di lavoro, la fiducia nel futuro e una forte credibilità internazionale. Ora sta a noi, classe dirigente del Paese, renderci meritevoli di questa fiducia, dando seguito alle tante sfide racchiuse nel PNRR. Ci abbiamo lavorato tanto, anche qui in Parlamento, e ora dobbiamo provare a raccoglierne i frutti, visto che le riforme e gli investimenti del Piano permetteranno alla comunità italiana di risollevarsi dopo i durissimi mesi della pandemia. ci dovranno aiutare a riconnetterci alle migliori tradizioni industriali del nostro Paese e a riannodare i fili di un rapporto con le istituzioni europee e con gli altri Stati membri che sia all'altezza della sfida che abbiamo davanti. Nella risoluzione che ci accingiamo a votare, signor Presidente, troverà diversi punti che le voglio evidenziare, con dei *flash*, come punti qualificanti della posizione del Senato. Abbiamo avuto contezza di alcune lacune nella costruzione europea per quanto riguarda il tema della sanità, che è vero essere di competenza nazionale, ma di cui è possibile esercitare meglio a livello europeo alcune competenze. Il vaccino ne è stato l'esempio più evidente. Per questo chiediamo al Governo di sostenere la finalizzazione del pacchetto legislativo relativo all'Unione europea per la salute, per offrire un'assistenza sanitaria di qualità e ridurre le diseguaglianze. Chiediamo anche al Governo di sviluppare il tema del digitale, continuando a perseguire contestualmente gli obiettivi della strategia UE per la sicurezza cibernetica, anche al fine di contribuire allo sviluppo di capacità industriali e di difesa realistiche e credibili nel rispetto delle prerogative nazionali. Come pure chiediamo al Governo di fare dei passi in avanti per arrivare ad una gestione strutturale europea del fenomeno migratorio, superando l'evidente stallo negoziale e politico relativo alla gestione dei flussi. Signor Presidente, abbiamo davanti uno scenario complicato, ma con la sua autorevole autorevole guida l'Italia sta facendo una parte importante, ancora più decisiva in una situazione in cui la Germania sta attraversando un momento di transizione politica e la Francia si avvicina alle elezioni presidenziali del prossimo anno. Abbiamo il dovere di crederci e di giocare la partita con il ruolo che ci compete. *(Applausi)*. presidente Draghi, la pandemia che ha sconvolto il mondo ha inciso significativamente anche sulle politiche dell'Unione europea. Di fronte al dolore e ad un'economia martoriata, abbiamo finalmente visto un'Europa solidale, degna del progetto dei suoi padri fondatori. In questo contesto, l'Italia si è trovata ad essere dapprima semplice beneficiaria delle decisioni storiche prese dall'Unione: mi riferisco al PNRR, grazie alla lungimiranza della cancelliera Merkel e del presidente Macron. Oggi, invece, grazie al suo arrivo a Palazzo Chigi e alla forza di una parte maggioritaria di questo Parlamento, che ha deciso di sostenere il suo Governo andando oltre i meri interessi elettorali, il Paese si trova nella condizione di poter giocare un ruolo trainante e da protagonista nell'Unione. La tornata elettorale tedesca ci consegna, infatti, una Germania più fragile, nella quale pezzi della maggioranza che sembra configurarsi sono promotori di politiche di *austerity*; ipotesi che va assolutamente scongiurata, perché quelle politiche hanno fallito e riattivarle segnerebbe una battuta d'arresto nel processo di crescita e integrazione europea. Nel prossimo Consiglio, quindi, sarà importante continuare a lavorare nel solco della solidarietà, mantenendo al centro dell'azione coordinata degli Stati la lotta al Covid-19 fino a quando non lo avremo sconfitto. L'Italia, anche grazie alla scelta coraggiosa del *green pass*, ha raggiunto risultati soddisfacenti nelle vaccinazioni. L'efficacia delle misure di contenimento del virus ci stanno finalmente facendo uscire dall'emergenza. Apprezziamo la chiarezza e la determinazione del Governo nel voler tutelare la salute pubblica, consci della necessità di non abbassare la guardia. L'attenzione va mantenuta alta, per evitare ciò che sta accadendo in Paesi come il Regno Unito, dove il "liberi tutti" ha fatto riesplodere i contagi, o la Russia, dove la scarsa copertura vaccinale ha fatto registrare nelle ultime ventiquattr'ore oltre mille decessi. La pandemia ci ha insegnato che il virus non ha frontiere. È quindi fondamentale che prosegua l'impegno comune contro questo nemico invisibile, per evitare che una situazione a macchia di leopardo possa far precipitare di nuovo le cose. Ciò passa anche dalla necessità, Presidente, che vi sia un maggiore impegno nella lotta alle *fake news*, che viaggiano veloci sulla Rete e che condizionano il comportamento di molti. Oltre al Covid-19, diversi sono i temi sul tavolo del Consiglio europeo ma, nonostante formalmente all'ordine del giorno non ci sia il tema Polonia, vista la lettera dei dodici Paesi con la quale si chiede di valutare la costruzione di un muro a protezione delle frontiere, per scoraggiare l'arrivo di migranti, ritengo comunque doverosa in questa sede una riflessione su questi due accadimenti. In rappresentanza di un partito, Forza Italia, che ha nell'europeismo uno dei suoi principi principi fondanti, non possiamo che rimanere perplessi di fronte a quanto deciso dal tribunale costituzionale di Varsavia, che ha messo in discussione il carattere sovranazionale dell'Unione. Su questo credo sia urgente un chiarimento, per evitare fughe in avanti di altri Stati membri, che altro non farebbero che minare lo spirito e la costruzione di un'Unione su cui faticosamente, a piccoli passi, stiamo lavorando. La questione posta dal tribunale polacco, presidente Draghi, ci pone, inoltre, di fronte a una questione dirimente: cosa si vuol far decidere all'Europa? Ricorrendo a quale metodo? Le decisioni all'unanimità paralizzano l'azione. Vogliamo provare ad assoggettare altre materie al metodo comunitario? Mi riferisco, per esempio, alle politiche fiscali, per cui l'Italia paga un prezzo molto alto alla mancanza di armonizzazione in materia di imposte dirette, dovuta proprio alla logica dell'unanimità. Credo che la sentenza polacca ponga anche la questione di cosa vogliamo diventi l'Europa dei prossimi anni. Per quanto riguarda, poi, l'iniziativa dei dodici Stati membri volta a un controllo rafforzato delle frontiere via terra, è evidente che, semmai ciò si dovesse verificare, il nostro Paese subirebbe un ulteriore intensificarsi dei flussi migratori via mare, in arrivo sulle coste meridionali attraverso la rotta turca, anche a seguito dell'aggravarsi della crisi crisi afghana. Il populismo cerca di dare risposte semplici a problemi complessi, ma i problemi restano tali, con la lente ideologica di chi vorrebbe, da un lato, innalzare muri e, dall'altro, spalancare le frontiere. Grazie all'iniziativa italiana, il tema migratorio è stato affrontato dal Consiglio europeo di fine giugno come non accadeva dal 2018. Nelle conclusioni di quel Consiglio è stato chiesto alla Commissione di presentare dei piani di cooperazione nei confronti dei Paesi che maggiormente pongono problemi di flussi verso l'Italia; tra questi ci sono l'Afghanistan, la Libia, la Tunisia, la Nigeria, il Marocco. La Commissione è stata, inoltre, invitata a ricorrere ai finanziamenti necessari. Come lei, riteniamo che tutte le rotte del Mediterraneo abbiano pari dignità. È indispensabile, dunque, che, con la riedizione dell'ingente contributo alla Turchia, il prossimo Consiglio europeo dia la spinta decisiva a definire e finanziare la cooperazione anche verso gli altri Paesi d'origine e transito, che devono essere messi nelle condizioni di prevenire le partenze e di avere strumenti efficaci per lo sviluppo. ovviamente - ma questo l'abbiamo detto decine di volte - serve riformare l'accordo di Dublino. Il Consiglio affronterà anche questioni relative alle relazioni esterne e a impegni internazionali. Il ruolo dell'Europa nel mondo non può prescindere da una politica estera estera e di difesa comuni, come chiedono da tempo Forza Italia e il nostro presidente Berlusconi. Se vogliamo un'Unione forte dobbiamo far comprendere agli amici europei che politica estera e di difesa sono strettamente interconnesse. Ma - e questo è il punto essenziale - dobbiamo intendere le politiche europee nel senso proprio del termine, mettendo in comune le scelte e assoggettandole alla regola della maggioranza. Nei prossimi giorni a Bruxelles si discuterà anche del recente aumento dei prezzi dell'energia e delle misure da adottare per ridurre le ripercussioni sulla nostra economia. Signor Presidente, mettiamo in sicurezza famiglie e imprese e sfruttiamo al massimo le opportunità che ci offre la Commissione europea e gli strumenti che ci consente di adottare a livello nazionale; tra questi, proroghe temporanee per il pagamento delle bollette, sostegni al reddito, aiuti alle aziende, sgravi fiscali mirati. Come lei ha ricordato, Presidente, sono già stati fatti dei primi passi, ma proseguiamo su questa strada con coraggio: ridaremo ossigeno agli italiani. Concludo con una riflessione sul Patto di stabilità e crescita, sulla cui revisione siamo tutti d'accordo, penso. Nelle prossime settimane si aprirà il dibattito sul tema e quanto più l'Italia saprà portare avanti le riforme e gli investimenti previsti dal PNRR, rispettando la tempistica che ci siamo prefissi, tanto più potremo chiedere flessibilità e l'esclusione di alcune spese per investimenti, come quelle collegate alle energie rinnovabili e al digitale. Bisognerà convincere gli altri Stati membri e il rispetto degli impegni presi sarà sicuramente il miglior viatico. Alla luce di tutto ciò, Presidente, le auguro un buon lavoro e non solamente in vista del Consiglio europeo, perché da qui ai prossimi mesi ci sarà davvero tanto da fare e noi collaboreremo con lo spirito che fino a oggi abbiamo avuto.

*(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente del Consiglio, colleghe e colleghi, il Consiglio europeo convocato per domani e venerdì andrà ad affrontare delle tematiche importanti: la pandemia, il digitale, il clima, la biodiversità, i prossimi vertici con Asia ed Europa, i prezzi dell'energia, l'immigrazione. Quando questo Parlamento ha approvato il Piano nazionale di ripresa e resilienza lo ha fatto consapevole che quei 235 miliardi di euro sono vincolati a delle riforme che il nostro Paese dovrebbe fare con scadenze fisse. Al fine di poter rispondere alle scadenze degli investimenti previsti, come Lega abbiamo da subito proposto di adeguare la normativa sul codice degli appalti a quella europea e di dar seguito alle indicazioni dell'Unione per una seria riforma della giustizia. Anche per questo, proprio in questi mesi come Lega abbiamo raccolto, grazie ai nostri volontari, centinaia di migliaia di firme in migliaia di piazze italiane su sei quesiti referendari, per essere da sprone al Parlamento ad attuare una seria e concreta riforma della giustizia, che tuteli realmente tutti i cittadini italiani e risponda così ai vincoli imposti da Bruxelles. Noi, con la nostra azione referendaria, vogliamo dare la possibilità agli italiani di esprimersi in una delle forme più alte della democrazia e della partecipazione democratica diretta, in modo tale da evitare che qualcuno, anche di questa maggioranza, possa ridimensionare o addirittura far naufragare una riforma che i cittadini aspettano da anni e che sarà prodromica all'ottenimento delle risorse del PNRR, fondamentali per la ripresa del nostro Paese. Sul tema immigrazione, signor Presidente, i dati parlano chiaro: dall'inizio dell'anno sono sbarcati sulle nostre coste 50.450 clandestini irregolari (dato al 19 il tutto mentre la tanto invocata solidarietà europea non decolla assolutamente, lasciando il nostro Paese completamente solo. Nello stesso periodo del 2020 si sono registrati 26.168 ingressi e nel 2019 9.148.

Noi più volte abbiamo apprezzato le sue parole di richiamo alla responsabilità congiunta dei Paesi dell'Unione europea. Non è accettabile che mentre il nostro Paese lotta quotidianamente nella gestione dei migranti, vi siano Paesi, come la Danimarca, dove i democratici di sinistra fanno approvare a larghissima maggioranza mozioni per evitare persino di avere gli *hotspot* sul suolo danese. Queste sono politiche discriminatorie non solo nei confronti dei migranti, ma anche e soprattutto nei confronti dell'Italia e degli italiani, alla faccia di ogni idea di ricollocamento e gestione condivisa. Questa sarebbe la sinistra europea che si fa chiamare socialdemocratica. *(Applausi)*. Noi, Presidente, dobbiamo trovare un meccanismo strutturato, stabile e permanente di redistribuzione obbligatoria dei migranti, che giungono sul territorio dei Paesi dell'Unione europea; o questo, o continueremo a veder morire persone nel Mediterraneo e ad avere un'Italia lasciata sola dagli altri Stati europei. Un'attenzione particolare va posta alla difesa del nostro agroalimentare. Troppe volte ci siamo sentiti soli a difendere la nostra agricoltura e la nostra pesca. Ancora una volta chiediamo che il Parlamento italiano si presenti unito nel difendere le nostre eccellenze. Ultima, in termine cronologici, è quella del vino Prosecco, una denominazione che rischia di essere bannata dal Prošek croato, che andrebbe a inficiare una delle produzioni italiane di eccellenza. È un *italian sounding* all'interno dell'Unione europea e questo non va assolutamente bene.

Ma lei, signor presidente Draghi, si deve impegnare in prima persona per difendere questa nostra eccellenza che vale 500 milioni di bottiglie e oltre 2,4 miliardi di fatturato al consumo. Con riferimento agli interventi finalizzati all'attuazione delle politiche del *green deal* europeo, in particolare alle misure di contenimento delle emissioni di anidride carbonica, esse devono necessariamente essere perseguite in maniera graduale senza impattare sulle abitudini alimentari e gli stili di vita dei consumatori, ed orientate ad un consumo equilibrato di tutti gli alimenti, secondo il modello della dieta mediterranea, a conferma della centralità del ruolo del *food made in Italy* per l'economia nazionale. Non abbiamo bisogno di lezioni da chi ci vuole imporre la carne sintetica o il cibo universale. Presidente, noi vogliamo che il consumatore possa liberamente scegliere anche in base alla stagionalità alimentare, perché, come lei ben sa, la natura ogni mese ci offre prodotti diversi. Il rispetto della stagionalità si riflette anche e soprattutto nel rispetto dell'ambiente e del pianeta, e ci permette di nutrirci con prodotti di qualità superiore ad un prezzo inferiore, perché i prodotti ci sono e sono freschi. Occorre poi che l'Unione europea riconosca la strategicità delle filiere agroalimentari italiane, dal grano duro alla pasta, all'olio, all'ortofrutta, al florovivaismo, con particolare riferimento alla straordinaria potenzialità del nostro settore zootecnico (latte, carne, uova). Nei riguardi di questo settore è opportuno mettere in campo più azioni volte, da un lato, ad aumentare la redditività delle imprese, degli agricoltori, dei contadini e, dall'altro, a garantire la sostenibilità degli investimenti sia per quanto riguarda *in primis* il benessere animale, sia anche per la salvaguardia dell'ambiente. Le cito questo tema non a caso: proprio ieri il Parlamento europeo ha scritto una pagina piena di ombre sul futuro dell'agricoltura e della zootecnia. Infatti, sta discutendo proprio in queste ore una relazione di iniziativa sul *farm to fork*, la strategia europea che dovrebbe declinare tutti questi obiettivi. Siamo partiti col piede sbagliato: la Commissione europea procede a tappe forzate, senza una valutazione di impatto complessivo, derubricando gli esiti negativi di diversi studi già pubblicati. Sia gli studi del Dipartimento di Stato americano sia quelli della Commissione sottolineano la perdita pesante di produttività delle aziende agricole europee, con il conseguente aumento dei prezzi, il rischio conseguente dell'aumento incontrollato delle importazioni, la possibile spirale negativa del settore zootecnico ancora nel mirino dell'ambientalismo da salotto per colpe che derivano da un approccio ideologico e non scientifico al tema della sostenibilità e del benessere animale. Un ultimo tema riguarda i cambiamenti climatici. Signor Presidente, nel nostro Paese l'agricoltura ha sofferto negli ultimi dieci anni una perdita di 14 miliardi di euro a causa della siccità, dei nubifragi, delle alluvioni e dei cambiamenti climatici in corso. Occorre pensare a una politica di sostenibilità sulle infrastrutture, soprattutto per quanto riguarda l'irrigazione. Il cibo è fatto per il 90 per cento di acqua e questo è un tema che non dobbiamo dimenticare. Sono partiti i primi progetti finanziati, ma occorre fare di più: riuscire a dare una regia corretta alla normativa sugli appalti e una garanzia che i produttori agricoli possano essere sicuri che gli investimenti che mettono in campo vengano realizzati.

parto dalla seconda parte del suo discorso e tornerò poi sulla parte incentrata sull'aspetto sanitario. Lei ha sottolineato l'importanza dell'intervento dello Stato per potenziare o addirittura far nascere i processi di transizione ecologica e digitale, ma a nostro avviso anche altri settori dell'economia necessitano di interventi pubblici per creare ricchezza, posti di lavoro e intere filiere produttive. A questo proposito, speriamo che ci si possa presto che ci si possa presto liberare di un pregiudizio antistorico e antieconomico, secondo cui l'intervento dello Stato è distorsivo del mercato o non efficiente. Al contrario, se portato avanti nella maniera giusta, è motore di progresso e sviluppo, come sta dimostrando la misura da noi fortemente voluta del *super bonus* 110 In proposito, lei ha fatto riferimento all'aumento dei costi di alcune materie prime. Ciò è avvenuto particolarmente nel campo dell'edilizia e probabilmente a causa di un orizzonte limitato temporalmente del *super bonus* 110 Se fosse stato prorogato quando il MoVimento 5 Stelle lo ha chiesto, ciò avrebbe consentito una migliore programmazione e, conseguentemente, nessuno o un limitato incremento dei prezzi rispetto a quello che, purtroppo, invece riscontriamo. Riguardo alla transizione digitale, l'obiettivo è che insieme all'Europa tutta si consolidi la sovranità digitale europea e in questo settore primario dell'economia si creino tanti posti di lavoro. di lavoro. Il digitale è un settore che può svilupparsi e rafforzarsi solo se si investe pesantemente nella formazione di elevate professionalità e specializzazione in un numero molto superiore all'attuale. Questo significa programmare, fin dalla scuola primaria, lo sviluppo delle competenze matematiche e scientifiche integrate nei nostri valori tradizionali umanistici ed etici, con l'obiettivo di precorrere i tempi per l'acquisizione di competenze fondamentali per realizzare la trasformazione digitale nel ruolo di protagonista e non di mera merce. Per questo servono insegnanti preparati e qualificati e occorre investire su di loro. Il tema delle competenze e del capitale umano deve essere al primo posto, anche perché è proprio qui che siamo più deboli, collocandoci all'ultimo posto tra i ventotto Paesi dell'Unione europea, secondo l'indice DESI. Sul tema della *cybersecurity* siamo molto soddisfatti per l'istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Si tratta di una presenza fondamentale per la difesa dei nostri *asset* strategici pubblici e delle nostre aziende private. Abbiamo investito per reclutare nell'Agenzia i migliori professionisti e in qualità sufficiente a svolgere il ruolo loro affidato. Chiediamo, d'altra parte, che anche i cittadini vengano tutelati

Tornando invece alla parte iniziale del suo intervento, il prossimo Consiglio europeo avrà tra i punti all'ordine del giorno la situazione epidemiologica e vaccinale.

percento della popolazione *over* 12 è vaccinata), ma anche una sicura e incontestabile efficacia dei vaccini approvati dall'EMA e dall'Agenzia italiana del farmaco. Non solo, la misura del *green pass* il recente ampliamento dei luoghi nei quali è obbligatorio esibire la certificazione verde (con particolare riferimento a quelli di lavoro) hanno permesso e permetteranno, come speriamo, un costante calo dei contagi, a dimostrazione - occorre ribadirlo ancora dell'efficacia dei vaccini e di un'efficiente e prudente gestione dell'emergenza epidemiologica, che ci vede sempre in prima linea rispetto agli altri Paesi. Ciò emerge anche in considerazione dei dati di altri Paesi, come Romania, Lettonia o Regno Unito, che certamente differiscono dai nostri non solo per l'aumento dei contagi, ma anche per l'allentamento delle restrizioni istituite per arginare la crisi pandemica. L'incremento dei casi in questi Paesi dimostra quanto le misure di limitazione e di controllo dei contagi siano ancora necessarie. Quanto esposto, però, secondo il MoVimento 5 Stelle non può prescindere da alcune modifiche, dal calmierare il prezzo dei tamponi cosiddetti antigenici fino, qualora la situazione epidemiologica continuasse a migliorare, a rimodulare le misure di prevenzione attualmente vigenti. Non solo, non possiamo più rinviare l'adozione dei test sierologici che misurino gli anticorpi neutralizzanti anti-SARS-CoV-2 allo scopo di ottenere il *green pass* o l'esenzione dallo stesso, come del resto stanno già facendo in altri Paesi, come ad esempio l'Austria, dove si ottiene il *green pass* con validità di 90 giorni sottoponendosi a un test sierologico che risulti positivo. Se adottassimo anche noi lo stesso criterio, risolveremmo anche il problema di tutti quei soggetti che si sono vaccinati con vaccini non autorizzati dall'EMA senza bisogno di ulteriori provvedimenti *ad hoc.* Inoltre, riteniamo inevitabili percorsi mirati di *screening* sierologico, anche con lo scopo di verificare le categorie e i soggetti che davvero necessitino della terza dose di vaccino, a parte i soggetti più vulnerabili, per favorire e garantire l'approvvigionamento di dosi ai Paesi in cui la campagna vaccinale stenta a decollare. Per giungere a questo scopo, il MoVimento 5 Stelle ha portato avanti una proposta, trasformata poi in un emendamento al decreto *recovery*, che prevede, in caso di emergenza sanitaria, l'obbligo temporaneo per i possessori di un brevetto su vaccini o medicinali considerati essenziali per la salute a concedere la licenza ad altri soggetti. Lo scopo dell'introduzione di tale licenza obbligatoria è stato ed è senza dubbio garantire un'equa diffusione di vaccini e medicinali tra tutti i Paesi, soprattutto quelli economicamente più svantaggiati. Concludo, pertanto, Presidente, invitandola a portare queste istanze al Consiglio europeo, perché se ci lasciamo guidare dalla scienza e dalla ragionevolezza delle misure, potremo anche arginare le proteste.

I testi sono in distribuzione. Ha facoltà di intervenire il presidente del Consiglio dei ministri, professor Draghi. ministri*. Vorrei ringraziare tutti i senatori per il contributo dato a questa discussione, che certamente informerà il mio intervento in sede di Consiglio europeo.

come si affronta questa sfida all'integrità europea che viene dalle sentenze delle Corti costituzionali nazionali, che rivendicano la primazia nella giurisdizione sulla Corte di giustizia europea. Qui la posizione non può essere che di fermissimo e convinto sostegno alla Commissione nell'azione che sta portando la prima sentenza che sfidò la primazia della Corte di giustizia europea venne dalla Corte costituzionale tedesca, che metteva in discussione l'efficacia della politica monetaria condotta dalla Banca centrale europea. La Banca centrale europea vinse in Corte di giustizia europea, in questo modo naturalmente contribuendo alla formulazione di una politica monetaria la cui strumentazione sarà diversa per sempre da allora in poi.

e per altri aspetti in Ungheria. A questo tipo di posizioni la Commissione europea sta reagendo con fermezza io credo che bisogna semplicemente sostenere quanto la Commissione europea sta facendo seguendo le procedure previste in questi casi. Vedremo come andrà a finire; certamente sono

senza però minare l'Unione europea nella sua politica di solidarietà, responsabilità e universalità della giurisdizione della Corte di giustizia. Si tratta, quindi, di un percorso difficile

Effettivamente, più si va avanti più si scopre che non riusciamo a vincere queste sfide globali, che travalicano il confine nazionale. non saremmo riusciti a vincere la sfida della pandemia, certamente non saremmo riusciti a vincere quella di costruire una ripresa dopo il disastro provocato dalla pandemia. È impossibile vincere la sfida del digitale, della transizione ecologica e a questo devo aggiungere che, visti gli ultimi sviluppi internazionali, non potremo mai vincere sul piano nazionale la sfida della Difesa. È chiaro che gli ultimi sviluppi hanno mostrato come inevitabile, necessaria la costruzione di una Difesa europea, la quale richiede un'enormità di mezzi che certamente un singolo Paese non ha.

ottobre: la stima della Commissione europea di fabbisogno di investimento addizionale privato e pubblico riguardo alla transizione verde e a quella digitale sarà di circa 650 miliardi di euro all'anno fino al 2030; la transizione verde soltanto comporterà investimenti per 520 miliardi per anno; i settori dell'energia e dei trasporti richiederanno una stima d'investimenti di 390 miliardi di euro per anno,

svolgerà necessariamente un ruolo unico e insostituibile, sia per le dimensioni degli interventi, sia per le molte circostanze in cui la solidarietà sarà necessaria, come è stato in passato. passato. Questi sono i fatti che in un certo senso accompagnano le nostre convinzioni ideali, perché non è solo per bisogno che si sta in Europa, ma per realismo e per idealismo.

Come questo possa avvenire non riusciamo a saperlo ora. È un momento, come avete detto, di grande transizione politica nei maggiori Paesi dell'Unione europea, quindi ci vuole certamente una situazione politica con un orizzonte davanti che permetta di riavviare il processo di ricostruzione dei meccanismi di decisione a livello europeo. Il secondo punto affrontato da alcuni di voi, in particolare

Per 6 milioni di piccolissime e piccole imprese e per circa 29 milioni di utenze domestiche sono azzerate le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il quarto trimestre di quest'anno. Per quanto riguarda il gas, per due milioni e mezzo di famiglie che beneficiano del *bonus*, sono stati tendenzialmente azzerati gli effetti del previsto aumento della bolletta nell'ultimo trimestre di quest'anno. Per tutti gli utenti di gas, famiglie e imprese, nello stesso periodo, l'IVA è stata ridotta al 5 per cento e gli oneri di sistema sono stati azzerati. quindi con enorme interesse e grande partecipazione l'iniziativa della Commissione che ha indicato la possibilità di consorziarci in acquisti comuni per avere maggior potere contrattuale, contrattuale, pubblicando altresì una lista di strumenti con l'indicazione di misure di breve periodo di alleggerimento degli oneri e proposte di medio periodo con riferimento allo stoccaggio, all'integrazione del mercato e alle comunità energetiche. È quindi stata avanzata la proposta di considerare acquisti congiunti di gas sostenuta dall'Italia. soffermarmi sulla riduzione dei combustibili fossili. Abbiamo fatto molto bene finora. Nel 2019 in Italia il 18,2 per cento del consumo finale di energia era prodotto con fonti rinnovabili;

dieci anni fa. Abbiamo fatto bene, dobbiamo fare ancora molto, ma è una partita difficile. Le considerazioni dei senatori Arrigoni e Girotto, pur da prospettive diverse,

Ci sono molte ragioni per pensare che una parte di questo aumento sia temporaneo. Il senatore Arrigoni ha citato il mancato utilizzo dell'eolico nel Mar Baltico, la siccità che ha inaridito alcune fonti idroelettriche. Ve ne sono però alcune che probabilmente sono strutturali; mi riferisco, per esempio, alla conversione delle centrali a carbone cinesi in centrali a gas.

che la Cina si fornirà di gas necessariamente europeo perché ad oggi non dispone di grandi produzioni di gas a livello nazionale.

e grandissima parte di questo gas è importata. È anche vero il fatto che, se noi tirassimo oggi più gas, questo sarebbe venduto ai prezzi internazionali, quindi a un prezzo che è più o meno quello mondiale, al netto però dei costi di trasporto e di altri oneri. Questo è un po' il conto che bisogna fare. Credo che attualmente dovremo continuare a percorrere con decisione la strada della transizione verde, affrontare la mitigazione degli oneri che l'aumento del prezzo del gas impone soprattutto ai più fragili e, nello stesso tempo, costruire delle soluzioni strutturali. Non è facile, ma è l'unica strada da percorrere. Di nuovo, una discussione di questo tipo in Europa, che avverrà domani e dopodomani, sarà una prima importantissima occasione per vedere un po' di luce in fondo a questo tunnel.

la senatrice Bonino, attualmente sono stati presentati otto piani di azione dalla Commissione per i Paesi prioritari, che sono Afghanistan, Bosnia-Erzegovina, Iraq, Libia, Marocco, Niger, Nigeria e Tunisia. Possono essere migliorati per quanto concerne le tempistiche e l'identificazione delle risorse finanziarie nel bilancio dell'Unione europea. Come ho detto in un'altra occasione, mi aspetto che la Commissione europea e il Servizio europeo per l'azione esterna assicurino al Consiglio europeo un costante aggiornamento sulla attuazione degli impegni e sulle risorse finanziarie, anche per una questione di trasparenza verso il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali. Sui rimpatri - ripeto quello che ho detto - è inoltre opportuno dare seguito all'impegno dei progressi europei sui rimpatri, troppo spesso e troppo poco attuati. Tali progressi richiedono più Europa; l'azione dell'Unione europea su tale questione è incomparabilmente più vigorosa, più efficace e più penetrante dell'azione svolta da un singolo Paese. Due parole sull'autunno che stiamo vivendo. Questa estate abbiamo continuato a far fronte agli obblighi internazionali di salvataggio in mare e di garanzia di protezione internazionale agli aventi diritto. Abbiamo fatto fronte a sbarchi, registrazioni e prima accoglienza, a dispetto della perdurante emergenza Covid; le cifre attuali indicano sbarchi di fatto doppi rispetto a quelli dello stesso periodo dell'anno scorso (al 19 ottobre sono stati 50.500, a fronte dei 26.000 dell'anno scorso). Circa 87.500 persone sono arrivate nell'Unione europea dal Mediterraneo via terra e via mare; di queste, circa 49.000 sono Infine, nella rotta del Mediterraneo centrale, dall'inizio dell'anno all'11 ottobre, sono morte circa 1.106 persone. persone. Di fronte a questi dati mi trovo a ripetere quel che dissi credo fin dal discorso iniziale di questo Governo: l'approccio del Governo non può che essere equilibrato ed efficace, ma anche umano. Efficace lo deve essere in due sensi: efficace nel proteggere i confini nazionali dall'immigrazione illegale e dai traffici di immigrazione, ma anche efficace nell'accoglienza. *(Applausi)*. È qui il punto, secondo me. Ricordo che proprio in quest'Aula dissi che, per trasformare gli emigrati in fratelli, occorre saperli accogliere

intendiamo investire in ricerca e competenze, nella strategia appena adottata dal Comitato interministeriale per la transizione digitale e prevediamo di potenziare il numero dei dottorati di ricerca da 9.000 a

abbiamo due progetti nel PNRR: ricerca di base e ricerca applicata. A proposito di quanto diceva il senatore Toninelli, sulla puntualità del Governo nell'informare il Parlamento,

la partecipazione delle donne al mercato del lavoro. Il Governo certamente predisporrà la relazione nei tempi previsti e i Ministri sono a disposizione per ogni informazione. Tra l'altro, il 23 settembre è stata data un'informativa nel Consiglio dei ministri sullo stato di attuazione e una cabina di regia presta attenzione speciale ai divari territoriali. Credo di aver terminato e vi ringrazio ancora.

era difficile immaginare che dopo la crisi sanitaria, il mondo sarebbe stato sull'orlo di una crisi energetica. Siamo in una strettoia dalla quale bisogna uscire senza cercare scorciatoie o adagiandosi su quella propaganda, che fa delle politiche di transizione ambientale la causa dell'aumento dei costi. Innanzitutto è necessario che continui, come lei ha appena illustrato, l'intervento statale per scongiurare un aumento dei costi delle bollette, per le famiglie e per le imprese, che intaccherebbe le prospettive di crescita economica. Serve anche un maggior coordinamento europeo, non solo sugli obiettivi, ma anche sulla legislazione, per lo sviluppo delle rinnovabili. per le Autonomie rappresentiamo territori come la Val d'Aosta e la provincia autonoma di Bolzano, che sono tra i principali produttori di energia idroelettrica, un'energia pulita e rinnovabile per definizione. non nascondiamo che siamo preoccupati, ad esempio, per il problema del rinnovo delle concessioni. In particolare, si avverte la mancanza di una normativa europea che omogenizzi le varie discipline soprattutto in merito alla durata delle concessioni. Ciò genera delle disparità e ci pone all'attenzione dei grandi gruppi stranieri, il cui interesse non sempre coincide con quello nazionale. È solo un esempio, ma rende bene l'idea sul tipo di lavoro che andrebbe fatto in un'ottica di rafforzamento e di diversificazione delle energie da fonti pulite. Ciò rimarca l'importanza dell'appuntamento, cui lei ha accennato, della COP26 a Glasgow fra poche settimane. Un altro tema che come autonomisti sentiamo di particolare importanza riguarda il ruolo degli enti locali nella gestione degli aiuti europei. Gli enti locali sono gli unici che in merito ai grandi progetti infrastrutturali hanno sensibilità e conoscenza dei territori tali da poter sviluppare iniziative che incidano direttamente nella vita dei cittadini rispetto alle grandi missioni del Piano. Per questo non bisogna solo fare leva sugli enti di di dimensioni elevate, ma bisogna mettere anche in condizioni i Comuni più piccoli di sviluppare e attuare i progetti per la rigenerazione urbana, esattamente come previsto oggi nelle linee guida di *governance* del PNRR. del PNRR. Voglio dire che su tutti i fronti dobbiamo coniugare dimensione globale e locale perché da sempre questa si è rivelata la strada per rendere concrete le visioni, ma anche per fare in modo che il particolare non fosse del Per questo anche per noi, che da sempre ci riconosciamo nei valori europei, è importante che l'Unione tenga la barra dritta rispetto a quelle situazioni - penso anch'io alla Polonia, che è già stata evocata molto in questo dibattito dibattito - che provano a minare i principi fondativi dell'Unione europea. È un problema se qualcuno pensa di poter rimettere indietro le lancette della storia, della storia, che va, invece, nella direzione esattamente opposta della sempre maggiore integrazione, elemento essenziale per usare le risorse per uscire da questa catastrofica crisi pandemica. Il prossimo banco di prova è la riscrittura delle regole comuni; sarebbe impensabile tornare ai vincoli del patto di stabilità. Il Covid non è una parentesi, ma un cambio di paradigma e un cambio d'epoca, una cesura tra il prima e il dopo.

che oggi è superiore rispetto all'epoca di Maastricht, sia perché, come lei ha ripetutamente spiegato, esiste un debito cattivo e un debito buono. Di sicuro si parla di debito buono quando ci si riferisce a investimenti sulla transizione ecologica, digitale e sulla sanità. Signor Presidente, apprezziamo molto l'attenzione che sta ponendo sulla transizione digitale, che rappresenta un altro cardine importante per lo sviluppo futuro del nostro Paese, soprattutto in territori particolari come quelli alpini. Siamo entrati in una nuova fase del graduale processo di fuoriuscita dalla pandemia: lo siamo dal punto di vista sanitario il suo Governo fa bene - da medico ne sono fermamente convinto - a tenere il punto per raggiungere quanto prima la soglia del 90 per cento I 40.000 casi del Regno Unito sono un monito per tutti perché non ci stancheremo mai di ripetere che più il virus infetta, più aumentano le possibilità di nuove minacciose varianti. La sua esortazione a investire di più su scienza e ricerca rappresenta un punto fondamentale per la crescita della nostra società. Aggiungerei anche di investire molto sull'informazione scientifica e in questo periodo ne abbiamo tanto bisogno. nuova fase anche dal punto di vista economico e noi che rappresentiamo i territori di montagna le possiamo dire quanto è grande l'attesa per la stagione invernale dopo che il turismo è stato mortificato per due anni consecutivi. alle politiche migratorie. Sono originario di un territorio, la Valle d'Aosta, da cui fino a ottanta anni fa molte famiglie dovevano emigrare per poter uscire dalla povertà. Se ci fossero stati muri tra Nazioni - quei muri che tornano oggi a essere invocati - quante nostre famiglie italiane sarebbero rimaste in miseria! Ritengo, quindi, che alzare barriere sia profondamente sbagliato; ma se le si invocano, vuol dire che qualcosa continua a non funzionare nelle politiche europee sulle migrazioni. L'Europa si faccia carico collegialmente del problema, e basta - purtroppo, siamo qui a dircelo da anni - lasciare soli i singoli Stati ad affrontare questo fenomeno epocale delle grandi migrazioni di popoli. In conclusione, al Consiglio di domani, signor Presidente, rappresenti la voglia e l'impegno dell'Italia per un'Europa al servizio di questi obiettivi: un'Europa che si faccia carico della crisi energetica, che non presti il fianco a chi vuole dividerla e che sia protagonista negli anni a venire. Annuncio quindi il voto favorevole alla risoluzione di maggioranza. *(Applausi)*.

è un'Italia che ricomincia a sorridere: i nostri dati economici sono addirittura migliori di quelli della Germania, grazie all'impegno delle italiane e degli italiani, dei lavoratori e degli imprenditori. C'è ottimismo nell'aria, frutto anche della prospettiva che abbiamo creato insieme in Europa, attraverso il Next generation EU. È la voglia europea di ripartire insieme: cosa che non era per niente scontata, anzi, la stessa Europa avrebbe potuto implodere, vittima di un egoistico ripiegamento dei singoli Paesi su se stessi. E invece l'Unione europea ha avuto la capacità di reagire e di mettere in campo misure di grande coraggio: SURE, sblocco del Patto di stabilità, *recovery fund*. Nel mezzo delle difficoltà, l'Europa ha dimostrato tutto il proprio valore, riuscendo a imporre politiche solidali e ad affermare un principio: soltanto uniti possiamo uscire al meglio dalle crisi. Adesso si tratta di ripartire da qui, vedendo se e come le misure adottate durante la pandemia possano trasformarsi in interventi strutturali, capaci di rendere l'Europa ancora più forte. Da qui l'importanza dei prossimi vertici del Consiglio europeo, destinati a segnare il futuro dell'Europa nei decenni a venire, a partire dal Consiglio di domani, che mette al centro del confronto un progressivo ritorno alla normalità, anzitutto dal punto di vista sanitario. Grazie ai successi derivanti dalla campagna vaccinale e dall'introduzione del *green pass*, è motivo di orgoglio il fatto che l'Italia stia facendo scuola a livello internazionale, con le norme introdotte in materia di certificato vaccinale, ad esempio. Alla faccia delle polemiche, infatti, l'obbligo di *green pass* nei luoghi di lavoro sta funzionando e determina un nuovo *boom* delle vaccinazioni, al punto che diversi Paesi esteri guardano con apprezzamento - e forse anche con invidia - alle regole da noi adottate. È positivo che all'ordine del giorno dei lavori di domani ci sia anche la questione dell'impennata dei prezzi dell'energia elettrica. La crescita repentina delle tariffe energetiche rischia di compromettere sia la ripresa economica che la transizione verde; c'è il rischio, infatti, che sorgano proteste che mettano in discussione le misure per la decarbonizzazione, accusate di essere la causa dell'aumento delle bollette. Ecco perché c'è bisogno che l'Europa affronti la questione e dica chiaramente che non è la transizione energetica a determinare l'aumento dei costi, non è la transizione energetica a determinare la perdita di posti di lavoro; semmai il caro prezzi dovrebbe convincerci ancora di più della bontà della conversione energetica. Se avessimo realizzato il *green deal* già anni fa, saremmo meno dipendenti dalle fonti fossili e dal gas naturale, e gli evidenti vantaggi climatici si andrebbero a sommare ai risparmi economici. Intervenendo in ritardo, invece, proprio il conto salato delle bollette rischia di innescare una spirale al ribasso delle ambizioni ambientali anche a livello di economie mondiali, Europa compresa, con danni irreparabili. Riteniamo che per contenere i prezzi sia necessario che l'Europa si doti in via preventiva di un sistema di stoccaggio comune europeo, così da non dover dipendere da possibili ricatti da parte dei Paesi fornitori di energia. Ecco che è importante che l'Europa definisca delle linee guida che consentano agli Stati di reagire prontamente. È necessario che il peso della transizione energetica non gravi sui più fragili. Ha ragione, presidente Draghi. Lei lo diceva nel corso del suo intervento: è una partita complessa, che non può essere rimandata e deve essere equa, così che possa essere condivisa e perseguita da tutti gli attori, anche i più recalcitranti. Contemporaneamente, serve un confronto internazionale costruttivo, che eviti che ci siano passi indietro nella lotta ai cambiamenti climatici e che consenta di pervenire a degli impegni concreti per la COP26 in programma a Glasgow a novembre; un appuntamento importante, dove è auspicabile che si arrivi con una posizione negoziale comune sugli obiettivi di riduzione delle emissioni, su cui possano convergere anche Paesi come Polonia, Bulgaria e Romania, ancora fortemente dipendenti dal carbone. Altro aspetto importante all'ordine del giorno è la digitalizzazione. La salvaguardia della ripartenza economica, sociale, commerciale, ma anche culturale, passa anche per la buona riuscita della transizione digitale. A questo scopo è strategico avviare una politica di messa in sicurezza dei dati attraverso la realizzazione di un *cloud* europeo, cioè una sorta di archivio telematico dove poter conservare e tutelare tutti i nostri dati. Allo stesso tempo, va favorita l'innovazione aziendale, operando affinché si riportino in Italia ed in Europa diverse produzioni strategiche, a partire ad esempio dalla produzione di semiconduttori. Insomma, signora Presidente, nonostante tutte le difficoltà e nonostante tutto, la pandemia ha ricompattato l'Europa. L'Europa ha dimostrato di saper reagire ed ha intrapreso una nuova strada.

presidente Draghi, signori del Governo, colleghi, abbiamo ascoltato le sue comunicazioni, presidente

tutti e sei i punti dell'ordine del giorno che discuterete domani; ma contiene anche, la nostra risoluzione, alcuni suggerimenti rispetto a quello che lei, signor Presidente, nelle comunicazioni invece non ha detto. Quello che colpisce è che la sua comunicazione, anche suggestiva in taluni passaggi, che poi dirò, è costruita giornalisticamente, ovvero con enunciazioni di titoli, ma manca sempre il come e il quindi. Il metodo di enunciazione dei titoli va bene, forse, per un Consiglio dei ministri, che deve dire sempre di sì, ma non va bene per un Parlamento. Per esempio, lei ha dedicato alla questione vaccini pochi minuti, i primi cinque del suo intervento. Ha giustamente sottolineato il successo della campagna vaccinale italiana, che ha definito più spedita della media europea. Fratelli d'Italia ha sempre sostenuto i successi della campagna vaccinale e non è un caso che tali successi siano iniziati dopo la sostituzione dell'*ex* commissario Arcuri e della sua mala gestione. Mi consenta solo un inciso: le tornerà utile in questi giorni rivedere quel *dossier* che le consegnammo, come delegazione di Fratelli d'Italia, durante un incontro. Tale *dossier* puntualmente quelle che, già allora, a noi sembravano evidenti opacità, per non dire di più, nella gestione commissariale dell'emergenza epidemiologica. Torniamo ad oggi. Concordiamo sull'esigenza, lo cito testualmente, di evitare quello che lei ha elegantemente definito protezionismo sanitario, che però ha avuto il significato, molto più pressante e meno elegante, di limitazioni delle libertà personali, di costi umani, esistenziali ed economici elevatissimi. Ci chiedevamo, presidente Draghi,

con l'estensione dell'obbligo di *green pass* ai luoghi di lavoro, con le conseguenze drammatiche che sono sotto gli occhi di tutti e che non sfuggiranno neanche a Bruxelles. E se è condivisibile - e lo è - l'impegno europeo, detto Covax, nei confronti dei Paesi a basso reddito, non si dimentichi, Presidente, che il Covax serve anche qui, con la stessa logica, perché sono tante e in aumento le sacche di emarginazione sociale ed economica, anche di quelle persone che liberamente manifestano scegliendo di non vaccinarsi. Infatti, in una Repubblica fondata sul lavoro (articolo 1), creare il precedente, come si sta facendo, che per lavorare serva un lasciapassare del Governo è inaccettabile e contraddice anche il principio di non essere discriminati sul posto di lavoro, così come vuole la Costituzione e come richiesto anche dall'Unione europea, che domani lei incontrerà in questo Consiglio. Presidente, in piazza manifestano pacificamente persone che hanno dubbi e che dovrebbero essere convinte e accompagnate. Non possiamo liquidare chiunque abbia dubbi sul *green pass* e sulla sicurezza dei vaccini come un criminale; lasciamo stare gli agitatori, ma nella stragrande maggioranza sono persone che manifestano pacificamente e dovrebbero farlo liberamente. Non vorremmo che con ciò si distraesse l'attenzione da quanto, invece, non è stato fatto, per esempio, per potenziare i mezzi pubblici o nelle scuole per evitare le classi pollaio. Sono pochi, Presidente, i minuti a un tema gigantesco come quello dell'immigrazione, rispetto al quale lei ha sostenuto - ed è vero - che i Paesi europei hanno preso atto dei rischi connessi ai flussi migratori irregolari e ha aggiunto che bisogna difendere le frontiere, comprese quelle marittime. Giusto, Presidente: peccato non aver sentito nulla su come farlo, visto l'aumento, ormai fuori controllo, degli sbarchi dei migranti, irritarvi) presidio navale, che impedirebbe a monte le partenze. Neppure ha detto nulla su come fermare gli arrivi in Europa dalla rotta balcanica e ha omesso di dire, come ha puntualizzato il collega Ruspandini, che c'è stata una lettera appello da parte di dodici Paesi europei, che hanno chiesto finanziamenti destinati alla difesa dei confini esterni, richiesta che l'Italia dovrebbe sottoscrivere. È bello sentirle dire che l'Unione europea deve fare di più; Presidente, lei non c'era, ma noi lo diciamo da anni. Ci accontenteremmo che l'Unione europea, invece di fare di più, iniziasse magari a fare qualcosa, visto che non ha mai fatto niente, lasciando l'Italia sola - sola! gestire l'emergenza migratoria. Gli accordi di Malta - ormai si sa - erano fasulli, perché non c'è stata alcuna assunzione di responsabilità concreta da parte dei Paesi dell'Unione europea. Questo lei potrà dirlo domani. Faccio soltanto un breve passaggio sulla parte suggestiva alla quale, invece, lei, Presidente, ha dedicato ampio spazio, che è compresa anche nella nostra risoluzione, che entra puntualmente nel merito, ovvero il tema della transizione digitale ed ecologica. Noi condividiamo - non abbiamo difficoltà ad ammetterlo, perché siamo un'opposizione intellettualmente onesta - gli impegni per recuperare il *gap* e le disparità che ci sono rispetto alla media europea. Vanno bene anche gli obiettivi sull'intelligenza artificiale e le buone intenzioni sul quadro normativo chiaro per la sicurezza

che parte di questi investimenti di cui lei ha parlato porti allo sviluppo di megafabbriche in Italia. Penso, ad esempio, a quella per la produzione di batterie elettriche a Termoli o a Torino, ovunque, altrove, comunque in Italia, per lo sviluppo industriale italiano. Questo avremmo voluto sentirle dire, Presidente. *(Applausi)*. E sempre a sottolineare quello che le sue parole non dicono, come ha anche evidenziato il collega Nastri, lei ci ha spiegato come fronteggiare il caro bollette, ma non ci ha spiegato esattamente come fronteggiare il caro energia, considerato che il prezzo del gas naturale resterà sopra i 200 euro/megawattora fino ad aprile. Ritorno al digitale: noi nella nostra risoluzione chiediamo di di rafforzare la *leadership* digitale dell'Unione europea e di garantire l'autonomia strategica con scelte tecnologiche autonome. Chiediamo, altresì, per favorire la transizione

tecnologica, cioè la possibilità di un *mix* autentico tra diverse fonti energetiche con lo sviluppo di un'apposita filiera industriale europea che riduca la dipendenza tecnologica. Questo c'è nella nostra risoluzione: un'autonomia dell'Europa nella produzione di fonti energetiche rinnovabili, garantendone al contempo la competitività nell'economia globale. Signor Presidente, noi vorremmo che la nostra risoluzione venisse approvata, perché i pericolosi sovranisti di Fratelli d'Italia hanno fornito

per esprimere il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico sulla risoluzione di maggioranza, ma anche per esprimere piena fiducia a lei, Presidente, nel momento in cui si recherà al Consiglio europeo. Sa di avere

il viatico migliore per presentarsi in Europa. La credibilità del Paese Italia serve anche a combattere le battaglie principali. Mi soffermerò su ciò che sta funzionando e ciò che non sta funzionando, in modo tale da fare anche qualche critica costruttiva che può essere utile

tranquillizzare i Paesi che da soli non ce la fanno, ma è un tema simbolico. Se l'Europa vuole essere faro della democrazia, se vuole essere conseguente rispetto alla capacità di esprimere valori liberali e di tutelare diritti fondamentali, lo deve manifestare non solo all'interno dei suoi confini, ma anche all'esterno, soprattutto nei Paesi che sono in ritardo di sviluppo e che incontrano difficoltà. In questa prospettiva, il tema dell'investimento nella ricerca e nella scienza deve trovare compiutezza nel progetto dell'Unione europea della salute; ne parleremo anche all'interno della Conferenza sul futuro dell'Europa per accompagnare lo sforzo che state facendo come Governo. L'altro grande tema è quello della politica industriale europea.

serve l'intervento dello Stato, inteso in senso largo, inteso come sovranità europea. È l'Europa che deve investire su un'idea di sviluppo, su una politica industriale europea, e deve saper accompagnare la fase di transizione ecologica e digitale, tutelando certo anche l'occupazione ed evitando quel derby cui spesso anche all'interno del nostro partito, tra partito del lavoro e partito dell'impresa. Si vince se si investe su un'idea di sviluppo sostenibile che tiene insieme imprenditori e lavoratori. Io vengo da una terra del Nord, dove spesso imprenditori e lavoratori, anche senza l'intermediazione del sindacato, trovano loro stessi la via per Da questo punto di vista dovremo prendere spunto. Penso che vada bene il lavoro che si sta facendo per riprendere e accompagnare un'idea multilaterale: il lavoro sul G20 e COP26. Vengo però a quello che non funziona, signor Presidente.

venite all'interno di quest'area di pace, benessere e prosperità; noi vi daremo una mano a colmare i ritardi di sviluppo e voi dovrete rispettare non solo le regole di un mercato comune, ma

al suo fianco ha i Gruppi parlamentari, i principali partiti e la società civile italiana. Non possiamo permetterci di diventare una fortezza europea che chiude i suoi confini con la logica delle piccole patrie, proprio nel momento in cui rischiamo di non essere più egemoni come Europa, l'attenzione si sposta sull'Indo-Pacifico e USA e Cina costruiscono nuove reti di relazioni internazionali. Se l'Europa non è forte e non parla con una voce sola, rischiamo di non contare negli scenari internazionali,

la dimostrazione anche simbolica che mettiamo in campo, il principio di solidarietà e, insieme, l'equa ripartizione delle responsabilità, che già è scritta dentro i Trattati e oggi dobbiamo e oggi dobbiamo trovare il coraggio di fare un passo in più. Lei lo ha detto nel suo intervento. Occorrono quindi non solo il contrasto e la prevenzione dei flussi irregolari; sfatiamo questo tabù e cominciamo a ragionare di immigrazione regolare, non solo per i corridoi umanitari, come ha detto, per chi scappa da guerre e persecuzioni politiche, ma anche legandola a un ragionamento di demografia, di *welfare* e di invecchiamento della popolazione. Perdiamo popolazione e, in vista del 2030, rischiamo di avere 4 milioni di persone in meno. non serve neanche più a colmare il saldo tra nati e morti: negli ultimi anni, abbiamo perso popolazione. Se non ragioniamo anche in termini di quote da Paese maturo, di cosa ha bisogno il nostro settore produttivo e di come dev'essere di come dev'essere aiutata la curva della demografia, rischiamo di perdere una partita fondamentale. Mi soffermo infine sull'attuazione dei piani. È giusto essere severi: abbiamo messo 6 miliardi sulla rotta balcanica ed è inaccettabile che si mettano solo 500 milioni sul *trust fund* per l'Africa. *(Applausi)*. Se non investiamo in quel Continente, rischiamo di perdere la partita. A me ha impressionato il colloquio avuto

e di analisi condivisa delle priorità. Fa bene a insistere sulla rotta meridionale, a fianco all'attenzione che ci dev'essere sul versante dei Balcani.

perché in Germania ci sarà una nuova *leadership*, che avrà bisogno di affermarsi, e in Francia penseranno alle elezioni. Sull'Italia ci sono molte aspettative e possiamo sfruttare anche quell'occasione per far passare messaggi importanti. Oggi non si vince da soli, ma insieme, come Europa unita.

In particolare, su questa proposta di risoluzione abbiamo posto nella maggioranza alcune questioni che riteniamo prioritarie per quanto riguarda

Adesso siamo arrivati al punto che si vuole ristabilire una sorta di sovranità e supremazia della normativa interna dei Paesi membri rispetto a quella europea.

delle delocalizzazioni). È veramente paradossale che oggi si metta in discussione, dalle basi, l'idea stessa dell'Europa. Questo è il punto. Pensiamo anche alle risorse. Abbiamo fatto tutti un grande sforzo con il PNRR e non ci stancheremo mai di dire qual è stato il grande investimento

Lo dico perché abbiamo fatto un grande lavoro sulle vaccinazioni e l'Europa sta lavorando su questo, ma dobbiamo capire una volta per tutte che il problema della della messa in sicurezza anche dei cittadini dei Paesi poveri è enorme e dobbiamo affrontarlo di petto. l'Europa dopo la pandemia - e non solo per quella - ha fatto la scelta del *green deal*, si è data obiettivi molto chiari e precisi al 2030 e al 2050 per la neutralità climatica e, alla luce di questi e anche delle assunzioni

decisioni molto forti in questo senso, come la lotta ai cambiamenti climatici e l'investimento sulla transizione energetica e sulle fonti rinnovabili. La capacità del nostro Paese e dell'Europa di affrancarci in modo molto rapido dalla dipendenza dai fossili è la chiave su cui dobbiamo lavorare. È chiaro che vi sono questioni complesse (nella sua replica ha giustamente

per agire nel contrasto al riscaldamento globale dobbiamo avere ben chiara l'emergenza in cui ci troviamo, perché anche la crisi energetica è una questione che stiamo toccando con mano, ma potremmo avere problemi molto più gravi d'impatto sulla vita delle persone.

che il nostro Paese, insieme all'Europa - perché questo è lo sforzo europeo - possiamo trascinare, creare nuova occupazione e sostenere anche chi ha bisogno di essere sostenuto, perché è nell'interesse collettivo. Altrimenti

indispensabile per fare un punto sull'efficacia delle misure adottate sia a livello comunitario sia dai singoli Stati membri. Questo Consiglio europeo, signor Presidente del Consiglio, è un passaggio nel quale l'Italia ha la possibilità di svolgere un ruolo di primo piano, come pilastro della stabilità in Europa. A tal proposito, i dati epidemiologici, l'andamento dei contagi, delle ospedalizzazioni e dei ricoveri in terapia intensiva e la ripartenza dei settori che hanno subito le maggiori ripercussioni nella fase più acuta della pandemia, ma anche la ripresa degli scambi e della libera circolazione dei cittadini in Europa dimostrano inequivocabilmente che la strada fin qui seguita ha pagato. Siamo passati - e lo abbiamo avvertito fortemente - dall'inseguire gli effetti della pandemia a gestirla, anticipandone, e quindi evitandone, le ripercussioni più drastiche. È indubbio che con il cambio di Governo, l'arrivo del generale Figliuolo e la riscrittura del piano vaccinale si sia avviata una campagna d'immunizzazione che ha avuto un grande successo.

con la dedizione degli operatori sanitari e l'incessante impegno delle Forze dell'ordine, così come con la solidarietà e la responsabilità che i cittadini hanno dimostrato davanti a eventi devastanti come questa pandemia, abbiamo certamente capito che sono il senso di appartenenza e il senso di comunità a fare la differenza. Se vediamo la luce in fondo al *tunnel,* lo dobbiamo a queste scelte coraggiose e talvolta impopolari che ci stanno inevitabilmente salvando la vita.

Le minacce nei confronti di chi responsabilmente promuove il vaccino, le violenze e le devastazioni nelle nostre città perpetrate al grido di "libertà" non sono soltanto un oltraggio alla maggioranza degli italiani, ma rappresentano una ferita alla democrazia. Questo è un grave errore, perché in un momento in cui la politica (come tutto il Paese ha fatto) è unita contro un nemico comune, non si può sfruttare l'occasione del dissenso di una minoranza violenta per fare propaganda Questi atteggiamenti non fanno il bene del Paese, perché hanno tradito quello spirito di reale unità che ha portato alla nascita di questo Governo e che avrebbe dovuto essere di esempio per tutti i cittadini. Sono orgogliosa del mio partito, Forza Italia, che ha saggiamente preteso che la politica trovasse risposte adeguate alle criticità sollevate da scienziati e tecnici. Sono orgogliosa che il nostro atteggiamento e le nostre ricette abbiano fatto sì che l'Italia si avviasse fuori dall'emergenza. Sia chiaro: questo non significa che la pandemia è superata, tutt'altro; il lavoro non è finito, dobbiamo portare l'Italia fuori dalla crisi. L'Italia è stato il primo Paese a vedersi approvato il PNRR, il più grande documento d'investimento che si è visto dal dopoguerra ad oggi, con cui potremo cambiare il volto del nostro Paese e portarlo nel futuro. Siamo stati i primi a ottenere 24,9 miliardi come anticipo dall'Unione europea in segno di fiducia per il lavoro che stiamo portando avanti e i primi a effettuare riforme come quella della giustizia e della pubblica amministrazione; adesso, con la prossima legge di bilancio, si passa dalla politica della domanda, fatta di sussidi, fondamentali nella pandemia, alla politica dell'offerta, per aumentare la crescita e ridurre le tasse per famiglie e imprese, attraverso il taglio del cuneo fiscale. di dire, non da economista, ma da madre di famiglia, che sa far di conto, che servono almeno 10 miliardi, quindi più di un terzo dell'intera manovra e lo possiamo fare anche grazie all'allentamento delle maglie del patto di stabilità europeo, una scelta giusta, tanto più perché è in atto una pandemia, con tutte le sue conseguenze sanitarie, economiche e sociali, che rende necessaria una politica sinergica e realmente comune tra i vari Stati dell'Unione, anche sul fronte dell'immigrazione. Il Mediterraneo bagna i confini europei, prima ancora di quelli italiani; non si può prescindere dall'ovvia necessità che la gestione del contenimento dei flussi migratori diventi una priorità politica di tutta l'Europa e smetta di essere un problema esclusivo dell'Italia. L'Europa è chiamata a farsi carico di una questione che sta investendo il nostro Stato, geograficamente esposto in maniera particolare, ma questo fenomeno riguarda l'intera Unione. Ciò ha che fare sia con il ricollocamento dei migranti, sia con le politiche da attuare in ambito internazionale, anche con i Paesi da cui hanno origine i flussi migratori. Sulla scorta di quanto fatto dall'Italia con i governi Berlusconi, bisogna stabilire un'interlocuzione forte e fattiva a livello europeo con gli Stati di origine o di transito per bloccare i viaggi della speranza, troppo spesso incentivati o favoriti, che, quando va bene, mandano in *tilt* il nostro sistema di accoglienza, e, quando va male, aumentano le già spropositate dimensioni del cimitero subacqueo che occupa i fondali del Mediterraneo. È arrivato il momento che l'Europa attui una politica estera e di difesa realmente comuni. All'emergenza Covid quest'estate si è aggiunta anche la crisi afgana, sfociata in una nuova emergenza, anche migratoria, che incombe su tutto il nostro Continente. Allo stesso modo, bisogna rispondere alla necessaria realizzazione delle infrastrutture digitali necessarie a proiettarci realmente verso il futuro. Il *gap* digitale divide non solo il nostro Paese, ma l'intero mondo in due. In Italia lo abbiamo visto con tutta evidenza con la chiusura delle scuole, con lo *smart* *working*, con la connessione che non arrivava ovunque, il *digital* *divide* fortemente marcato fra le aree del Paese, la didattica a distanza la didattica a distanza che ha creato studenti di serie a e di serie b. Durante il *lockdown* e, più in generale, nel corso delle limitazioni che hanno comportato anche lo *stop* del lavoro in presenza, non per tutti e non ovunque è stato possibile lavorare da casa. Dalla funzionalità e dall'accessibilità della rete dipendono ormai lo sviluppo e la crescita della società. Se forniremo ai cittadini la banda larga, collegheremo i nostri figli all'istruzione, i nostri anziani alla telemedicina e alle più moderne forme di cura effettuabili anche da remoto, nonché le famiglie e le persone tra loro, chi offre lavoro con chi lo cerca, e proietteremo i giovani verso il futuro. L'impegno dell'Italia al prossimo Consiglio europeo dev'essere improntato a questi punti, che costituiscono una condizione indispensabile per rialzarci e rialzare l'intera Europa dalle macerie lasciate dal Covid. L'Italia può essere protagonista di questo cambiamento: abbiamo tutte le carte in regola perché ciò avvenga, la possibilità di contribuire a disegnare un'Europa realmente solidale al proprio interno e l'opportunità di uscire da questa crisi più forti di prima. È indubbio che tutto questo è possibile grazie alla sua autorevolezza, signor Presidente, ad un Governo forte e stabile, ad un'ampia maggioranza che lo sostiene e, mi permetta di dirlo da questi banchi, anche grazie a un Parlamento che si è messo in sintonia con il Paese. È questo il mandato che con la risoluzione di maggioranza voteremo convintamente e che affidiamo a lei, signor presidente Draghi, in vista del prossimo Consiglio europeo, nella consapevolezza che è indispensabile spianare la strada verso un nuovo modo di intendere e rafforzare le politiche comunitarie,

democrazia. A queste ritualità parlamentari non ci vogliamo però disabituare, quindi oggi voteremo una proposta di risoluzione che ha avuto il favore del Governo e che è stata scritta dalle forze di maggioranza.

dal sottosegretario Amendola. Indubbiamente, trovare una sintesi sui temi all'ordine del giorno del Consiglio europeo non è stata cosa complicata.

per quanto riguarda la politica estera. Se non si parte da lì, è difficile poi riuscire a trovare una ragione di tutto il resto. Lei ha fatto un'affermazione che può essere sottoscritta (difficilmente non può esserlo): non si sta in Europa solamente per interessi, ma anche per ideali.

Tornando alle questioni, le sono state sottoposte attenzioni e sensibilità da parte di tutti i Gruppi. Abbiamo accennato - e lo abbiamo fatto in maniera compiuta - alle grave difficoltà relativa alla crisi energetica. Non perdiamo di vista questo aspetto, che qualche analisi mette in evidenza. Ne cito testualmente una, che ho trovato molto interessante: attenzione, perché la frenata cinese ci deve impensierire. La Cina non è solamente un concorrente da tenere distante, in quanto invasivo rispetto alle nostre economie, ma è la locomotiva che ha trainato l'economia mondiale e che adesso rischia di metterla in crisi, anche per la sua incapacità di gestire il suo grande *boom*. Alla Cina si aggiunge la possibilità di una crisi energetica globale strisciante e permanente, che distrugge la domanda nell'industria e toglie potere d'acquisto alle famiglie. Attenzione: se la risposta dall'altra parte dovessero essere restrizioni fiscali e monetarie premature, in presenza di un livello di indebitamento che non ha precedenti, rischiano di soffocare la nascente ripresa delle famiglie. Da qua ovviamente la riflessione va sull'azione che deve fare il Governo,

che non basta trasferire quote di finanziamento dal livello periferico a quello centrale, ma che serve anche una politica fiscale comune; qui continuiamo a essere in arretrato, con concorrenze, anche al suo interno, che certamente la dicono lunga rispetto a un'Unione europea che continua a essere molto accennata, ma non completata.

Se di fronte alle incapacità dell'Unione europea di affrontare i problemi non ci poniamo la domanda di come superare queste situazioni, stiamo nascondendo il problema sotto il tappeto, pensando che si risolva da solo.

Quando poi il ricatto aumenta, non c'è più la capacità di sostenere quel pagamento e si resta prigionieri dello stesso meccanismo che si è innescato. Dobbiamo portare la stabilità in quei Paesi dove oggi invece si genera il problema della migrazione e dove lo stesso viene indirizzato, con origine politica, come sappiamo. Mi consenta di essere un attimo

tanto superficiali da pensare che basti mettere i soldi in un sistema di accoglienza per creare integrazione, perché sappiamo che non è così. C'è integrazione, se c'è il lavoro.

Ieri c'è stato un dibattito qui, in Aula. Fra pochi giorni ci sarà il G20 in Italia, concluderemo la nostra Presidenza abbiamo bisogno di avere certezza che nel Governo tutti siano responsabili, come lei sta dimostrando a livello europeo. Quindi anche la gestione della sicurezza interna dev'essere messa a fuoco, altrimenti rischiamo di fare brutte figure a livello europeo e a livello generale. presidente Draghi, non spendo altre parole, anche perché sarebbero solo ripetitive rispetto ai temi che sono già stati affrontati. Siamo sempre convinti che la nostra azione in Europa debba essere innanzitutto di orgoglio, certamente attiva, non passiva e non remissiva.

saluta con soddisfazione le parole del presidente Draghi sulla transizione ecologica. Ce n'è voluto di tempo, ma adesso

Anche questo è un piccolo obiettivo che abbiamo raggiunto negli ultimi mesi: cercare di far capire alla gente che dietro alla transizione ecologica ci sono aziende più veloci e più moderne, moderne, suoli da bonificare, energie da trasformare, abitazioni che devono essere implementate energeticamente e davvero un nuovo modello di economia,

che tutte le crescite sono possibili, ma solo a patto che siano sostenibili. *(Applausi)*. Questo è il primo concetto che dobbiamo portare in Europa. lei andrà a Bruxelles e si troverà davanti uno dei temi più scottanti del momento, che è quello dell'energia.

perché, se solo avessimo iniziato la nostra transizione ecologica dieci anni fa, non avremmo sofferto l'aumento del prezzo delle bollette e dell'energia.

ha fatto piacere averla ascoltata nel passaggio in cui ha detto che l'aumento del costo dell'energia è un problema legato alla dipendenza energetica dell'Unione europea

è soddisfatto attraverso l'importazione di petrolio e gas naturale fuori dai confini dell'Europa. È una quota che addirittura sale al 75 per cento per il nostro Paese. andiamo a Bruxelles con il problema del caro bollette, su cui il Governo doverosamente ha messo mano con interventi pubblici di mitigazione dei costi, ma si combatte solo in un modo:

La strada è solo una: investire nella ricerca di nuovi fonti rinnovabili, promuovere la decentralizzazione della produzione energetica rinnovabile e stimolare l'autoconsumo collettivo, che è rappresentato dalle nostre comunità energetiche. Creiamo comunità energetiche. La misura del MoVimento 5 Stelle è un invito; approfittiamo anche di questo palco che ci dà il Parlamento per rivolgerci ai cittadini: unitevi insieme; create comunità energetiche; siate voi produttori di energia per poterla vendere. L'energia non fa perdere soldi, ma li fa guadagnare. Non avete bisogno del sindaco o del Comune per poterlo fare. Ci sono interi paesi che si sono resi autonomi da un punto di vista energetico e la gente non lo sa. Le persone non sanno che ci sono comunità che ormai non pagano più un euro di energia, perché se la fanno da soli. Dobbiamo promuovere: questa è la strada che ci può portare davvero verso una democrazia energetica.

Leggo sul giornale oggi che il superbonus è prorogato al 2023, ma restano escluse le ville e le villette.

a tutto quel segmento di fasce deboli che, anche da un punto di vista produttivo, dev'essere preso in considerazione. *(Applausi)*. Facciamo attenzione a non tagliare questa misura in modo tale che non vada a esclusivo detrimento dei dei tornitori, degli elettricisti, degli idraulici, dei piccoli imprenditori edili, di quel settore dell'edilizia che solo adesso stava vedendo la luce, dopo quindici anni di crisi. Abbiamo apprezzato che pian piano il superbonus abbia quasi smesso di essere una misura del MoVimento 5 Stelle, perché è diventato un po' l'emblema del riscatto e della ripresa economica italiana. *(Applausi)*. Siamo contenti, perché i temi non sono nostri; sono vie di sviluppo che offriamo ai cittadini. Lei deve offrire ai cittadini forme di sviluppo che possano naturalmente portare verso una forma di transizione ecologica che rispetti effettivamente sia il pianeta che le persone. Da questo punto di vista, ragioniamo qui in Parlamento, vediamo come poter migliorare il superbonus 110 per cento, senza frustrare senza frustrare le aspettative e i diritti di tutte quelle categorie che ho citato. Passo alla digitalizzazione che, come sa, è il secondo tema che ci sta più a cuore: la transizione digitale viene immediatamente dopo la transizione ecologica. Non esiste la ringraziamo, e guardi che non stiamo parlando solo di garantire la competitività dell'Europa nel campo dell'innovazione digitale. No, qui è in ballo la sovranità tecnologica dell'Europa; quindi, mi raccomando, l'Italia da tempo è capofila di un nuovo corso economico e sociale. Siamo punto di riferimento per l'Europa intera e vogliamo vedere in lei il punto di riferimento perché possa effettivamente portare questo Paese pian piano, finalmente, verso un futuro di prosperità e di occupazione per i nostri giovani.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

mozioni su iniziative volte a contrastare ogni forma di violenza e di totalitarismo. Ha facoltà di parlare il senatore Parrini per illustrare la mozione n. 422. Presidente, procedo a illustrare la mozione n. 422, che abbiamo depositato come Partito Democratico dopo i fatti del 9 ottobre. Noi partiamo innanzitutto dalla considerazione che ci troviamo di fronte ad avvenimenti molto gravi che non dobbiamo assolutamente circondare di sottovalutazioni. Abbiamo visto la devastazione ad opera di un movimento dichiaratamente fascista contro un sindacato: è un fatto inaccettabile, com'è inaccettabile ogni atto di violenza politica illegale. è un atto che è reso ancor più inaccettabile dalla circostanza che eventi del genere richiamano pagine tra le più buie della storia del nostro Paese - un movimento fascista che assalta un sindacato

a cui va la nostra solidarietà - che riunisce milioni di lavoratori. *(Applausi)*. La CGIL rappresenta un pilastro della nostra democrazia e una forza di coesione sociale nel nostro Paese. Sono stati fatti di eccezionale gravità, dobbiamo dircelo: ci sono stati quasi 40 feriti tra Forze dell'ordine, giornalisti, comuni cittadini. Questo episodio di violenza è stato - anche questo va detto - l'ultimo di una serie, ma più esecrabile di tutti gli altri che lo hanno preceduto.

fascista e antidemocratico della propaganda e dell'attività di questo movimento. E vogliamo dire con grande forza in Parlamento che non sono molto comprensibili per i cittadini normali le discussioni su quale sia stata la matrice delle violenze del 9 ottobre. delle violenze del 9 ottobre è chiaramente fascista, per le parole dette, per i propositi enunciati, per i fatti messi in campo e per il nemico scelto. Quindi, nella nostra mozione diciamo anche che è altamente condannabile qualsiasi ambiguità sul punto crediamo che nessuno debba avere alcuna difficoltà a riconoscere la matrice fascista di quella serie di avvenimenti che abbiamo ricordato. Come sappiamo, nella storia del nostro Paese la violenza politica illegale di diversa origine, purtroppo, si è affermata come fatto di grande rilevanza pubblica in più momenti e con particolare gravità. Sappiamo che ci sono precedenti nei quali è stata applicata la cosiddetta legge Scelba, che fu fatta nel 1952 per dare attuazione alla XII disposizione transitoria e finale della Costituzione. Sappiamo che questi precedenti riguardano Ordine Nuovo nel 1973, dopo una sentenza di primo grado; Avanguardia Nazionale nel 1976, anche in questo caso dopo una sentenza di primo grado; Fronte Nazionale nel 2000, sciolto con un decreto del ministro Bianco dopo una sentenza di terzo grado. Conosciamo questi precedenti, sappiamo qual è la storia del nostro Paese e vediamo che, a nostro avviso con grande chiarezza, i fatti del 9 ottobre determinano l'entrata in scena di quegli elementi di fatto che fanno scattare l'applicabilità della legge Scelba appena menzionata. La legge Scelba, con le integrazioni apportate dalla legge Mancino, attribuisce, di fronte a fenomeni come quelli del 9 ottobre, competenze precise alla magistratura e al Governo, verso le quali noi abbiamo il massimo rispetto. Ferme restando queste competenze, riteniamo che il Parlamento abbia, di fronte a fatti come questi questi e alla luce della loro eccezionale gravità, non soltanto il diritto, ma anche il dovere di levare la propria voce e di esprimere una posizione chiara. La nostra posizione, che esprimiamo in maniera ferma e composta ma con grande chiarezza, è che nei modi previsti dalla legge si debba arrivare allo scioglimento di Forza Nuova. *(Applausi)*. Nel dire questo, il Parlamento non fa niente di meno che il proprio dovere, non invade alcuna competenza, assolve ad un obbligo morale e politico: crediamo che questo debba essere ben chiaro. Da alcune parti - e mi avvio a concludere ci è stato chiesto di condannare tutte le forze eversive. Voglio dirlo con forza: stupisce che si possa dubitare della nostra opinione in merito. Io rappresento un partito che si chiama Partito Democratico non per un capriccio semantico o aggettivale *(Applausi)*, ma per una ragione profonda. Chi siede su questi banchi conosce molto bene non soltanto la XII disposizione transitoria e finale, ma anche l'articolo 18 della nostra Costituzione, che dice che non ci si può riunire come singoli in associazione per fini vietati dalla legge, così come conosce l'articolo 270 del codice penale e - lasciatemi dire - conosce anche l'articolo 49 della nostra Costituzione, che dice che i partiti sono determinanti

Non possiamo giocare a buttare la palla in tribuna o in calcio d'angolo. Il Parlamento si riunisce oggi, 20 ottobre, a undici giorni da fatti che hanno una connotazione precisa e che ho ricordato, e nelle supreme Assemblee popolari siamo chiamati ad esprimere un giudizio su quei fatti, non a parlare di altro per sminuirne la gravità. Credo che in in questa Assemblea siamo anche chiamati ad essere memori che abbiamo una Costituzione che ha una precisa origine, che deriva da precise lotte e che non configura la possibilità di scioglimento genericamente per forze che vanno contro la democrazia e l'ordine costituito, ma prefigura la possibilità di scioglimento esclusivamente per forze di cui sia accertata la volontà di ricostituire un partito che adotta i metodi del disciolto partito fascista. *(Applausi)*. Nella nostra Costituzione, come al solito, si trovano molte risposte alle domande dell'oggi.

e delle attività di questi gruppi neofascisti, alcuni dei quali si sono segnalati in modo molto chiaro, tant'è - arrivo così al punto - che non soltanto, come abbiamo visto, il 9 ottobre è Forza Nuova che guida l'assalto alla CGIL, ma proprio su Forza Nuova vi sono stati già pronunciamenti della magistratura, vi sono state già sentenze nel merito, proprio sul carattere fascista e di riorganizzazione del partito fascista.

che sono spesso, come alcune sentenze della magistratura ci dicono, costellate da atti veri e propri di aggressione e di violenza. Su questo dobbiamo essere molto chiari,

(comma primo) della Costituzione, si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione o un movimento - o comunque un gruppo di persone perseguano "finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando

che sgombra il campo e che dice con chiarezza e solennemente qual era la matrice dell'assalto fascista, che respinge e invita anche le forze qui presenti a respingere tutti gli atteggiamenti ambigui sul punto, perché questo riguarda il il rispetto dei valori costituzionali.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, la richiesta di scioglimento di un movimento politico è una misura estrema, che occorre sempre valutare con grandissima attenzione. Si tratta di una decisione politica prima ancora che di un meccanismo di ordine pubblico, quindi non può germinare dall'emozione di un momento: deve essere ponderata e soprattutto fondata su quei principi e quei valori che inverano la Costituzione, evitando di farne strumento di lotta politica e di utilizzarla come fosse una clava contro l'avversario politico. però, signor Presidente, non è in discussione la libertà delle idee. Apprezzi il fascismo? Molti di noi avrebbero e hanno buoni argomenti per dimostrare che si trattò di un regime totalitario che si servì dello squadrismo armato per andare al potere. I morti ammazzati furono più di 3.000, un paio di migliaia i circoli e le sedi sindacali e operaie distrutte, le leghe bracciantili devastate. Un calvario che durò perlomeno quattro anni. Alcune centinaia furono i sindaci bastonati, esiliati, commissariati con la complicità dello Stato liberale. Il punto, dunque, non è oggi e qui la libertà delle idee; il punto è la ricostituzione di una forza politica che si richiama e che è di stampo fascista, che utilizza e applica la lotta armata come metodo di iniziativa politica.

è accaduto, è un fatto; le minacce di ripercorrere questa strada in un futuro sono un altro fatto e non un'opinione. Mi domando anch'io perché non si sia intervenuti con decisione per scongiurare l'attacco alla CGIL visto che non era decisamente ignoto, ma questa evidenza non cambia naturalmente lo stato delle cose, tanto meno anzi ne riduce la gravità. C'è dell'altro e c'è di più: la coerenza mai profanata dai protagonisti. Forza Nuova non nega l'ispirazione che la muove e molti dei suoi dirigenti hanno processi in corso per violenza, non per opinioni inneggianti al Ventennio: atti concreti e non gesti simbolici. Questo è il punto di confine e questo è il discrimine. Se questo è il discrimine, quanto meglio avessimo ascoltato giorni fa un coro unanime di voci di condanna, non solo dei fatti accaduti sabato 9 ottobre, ma del fascismo senza bisogno di altri aggettivi. Era sufficiente una parola: basta con quel passato. Non tutti l'hanno detta. C'è chi ha preferito girarci intorno piroettando tra le pagine del Devoto-Oli. La cosa giusta da fare sabato scorso era aderire alla manifestazione indetta unitariamente dai sindacati, tutti i partiti, senza eccezione alcuna, magari qualcuno tappandosi il naso, magari mettendosi sulla scia dell'articolo pubblicato molti anni fa dal quotidiano «l'Unità» in omaggio a Gobetti, malgrado i difetti insiti nella sua origine culturale, fu un sincero amico della classe operaia. C'è dell'altro: il clima in cui questi eventi maturano, la somma tra un forte cambiamento che si innesta su una grave crisi socio-economica. Le istituzioni sono le prime ad essere messa nel mirino; non solo le istituzioni degli eletti, ma quelle che hanno articolazioni territoriali e rappresentano un mondo, come il sindacato. annoverate anche le istituzioni parlamentari: ricordo il Senato solo pochissimi anni fa, una manciata di anni fa, trattato - si scrisse - come fosse la latrina della Nazione, una scatoletta di tonno da aprire, urla inneggianti all'uomo solo al comando, peggio che se fossimo su un *set* cinematografico. Non dimentico nemmeno i *flirt* con il complottismo no vax, secondo la tesi pericolosa che la libertà è un privilegio individuale da non condividere mai con nessuno. Per queste ragioni il Gruppo Italia Viva-PSI, nel rispetto della Costituzione, citata dall'amico senatore Parrini e dall'amica senatrice De Petris; nel rispetto della legge, citata da chi mi ha preceduto, rispetto delle sentenze della Corte costituzionale, tutte di una chiarezza inequivocabile, chiede al Senato di impegnare il Governo ad adottare provvedimenti di sua competenza per procedere allo scioglimento di Forza Nuova. A tal fine questo Gruppo confluisce nella mozione unitaria che condivide questa prospettiva. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nella giornata del 9 ottobre, in pieno centro a Roma, si è svolta una manifestazione contro l'estensione dell'obbligo del *green pass* alla generalità dei lavoratori, che è sfociata purtroppo in una serie di episodi di inusata violenza e vandalismo, che conosciamo tutti. Sono i motivi per i quali noi oggi siamo qui qui e siamo chiamati a un'assunzione di responsabilità. Quanto è accaduto nella sede nazionale della CGIL è un episodio che fa male a tutti noi parlamentari rappresentanti delle istituzioni, ma soprattutto cittadini. È stato compiuto infatti un atto violento contro la democrazia e contro la Costituzione italiana Dobbiamo capire bene il solco sul quale ci muoviamo, che è costituito da due strade: una è quella costituzionale, l'altra è quella normativa delle nostre leggi che sono in vigore da troppo tempo e non sono state nemmeno applicate. Pensiamo alla legge 20 giugno 1952,

ma attenzione a non assumersi finalmente oggi la responsabilità verso un atto che ha delimitato il superamento di un limite forse già superato tempo fa, per il quale fin troppo si aspetta un intervento delle istituzioni e della politica italiana.

Se guardiamo però poi le norme transitorie e in particolare la XII norma di attuazione transitoria della nostra Costituzione, noi rientriamo in quel perimetro. Noi oggi non facciamo altro che applicare quel perimetro costituzionale attraverso la richiesta della valutazione dell'applicazione della legge Scelba del 1952. essere da monito in quanto rappresentanti dei cittadini italiani. Attenzione, colleghi: si prende una posizione una posizione contraria a quello che è stato fino ad oggi, soffiando sul vento di alcuni movimenti sovversivi ed eversivi perché facevano comodo al proprio partito e alla propria compagine politica. Bisogna avere coraggio oggi. Ecco il coraggio e la responsabilità dei rappresentanti delle istituzioni. *(Applausi)*. Si può essere di un partito di sinistra o di destra, ma destra non vuol dire essere per forza fascisti. Se fossi un rappresentante di destra, sarei antifascista, chiaramente antifascista perché, essendo un rappresentante di una compagine politica, prima ancora viene il rispetto della nostra Carta costituzionale. È questo che chiediamo: semplicemente l'applicazione della Costituzione attraverso l'applicazione della legge Scelba. Per questo motivo il MoVimento 5 Stelle aderisce all'impegno chiesto dalle altre compagini che mi hanno preceduto, chiedendo di valutare gli elementi per lo scioglimento di Forza Nuova e di altre forze simili, eversive e fasciste.

c'è anche la condanna dei totalitarismi e di ogni forma di violenza. Fratelli d'Italia è un partito che non deve fare i conti con la storia, distinto e distante da ogni esperienza politica che voglia affermare il metodo della violenza nella lotta

2009, di condanna di tutti i totalitarismi e di ogni forma di violenza perpetrata dai regimi comunisti nell'Europa centrale e orientale, debba trovare anche in quest'Aula

la violenza e il totalitarismo non vanno bene, da qualunque parte provengano. Noi riteniamo che fare i conti con la storia e con con l'attualità del mondo rappresenti una necessità per tutte le forze politiche, per dire tutti insieme, in questa occasione, che che ci si riconosce nella democrazia, che non ci sono persone che rilasciano patenti e che non si possono assolutamente strumentalizzare vicende che ricevono una condanna unanime. Dobbiamo necessariamente dire che il mondo, se vive un pericolo, lo vive da parte dei regimi totalitari comunisti, come i rapporti affermano in oltre 34 Nazioni. E dobbiamo necessariamente insieme condannare anche chi ha rapporti con quei regimi che non coltivano il valore assoluto della libertà. vogliamo giungere a questa definizione e aspiriamo all'affermazione della condanna di ogni violenza. Voglio ricordare anche i 215 milioni di cristiani che sono che sono perseguitati in tutto il mondo da regimi islamici, che proprio nelle terre di origine della cristianità tendono a cancellare questa identità. Non dobbiamo assolutamente cedere alla vergogna della nostra identità. Noi chiediamo, con la nostra mozione, una serie di impegni al Governo in questa direzione. Ma, proprio perché aspiriamo, aneliamo e speriamo che ci sia lo stesso atteggiamento da parte di tutte le forze politiche,

con uno spirito estremamente positivo. E questo perché - forse a nessuno interessa - io vivo e sono stato sindaco in un Comune decorato dalla medaglia d'oro al valor militare per la strage di Sant'Anna di Stazzema, in cui sono morte 560 persone, oltre ad essere uno dei primi iscritti all'anagrafe antifascista del Comune di Stazzema e del Parco nazionale della pace. La mia tradizione socialista mi ha portato quindi sempre ad avere chiari il mio punto di vista e la mia posizione. Non serve che io testimoni il fatto che sono antifascista. Io sono italiano, repubblicano e ho voluto testimoniare con la mia sottoscrizione e la mia adesione un principio e un valore importante che hanno caratterizzato la Repubblica dal 1948 in poi. in poi. Ora, siccome uno dei principi costituzionali e repubblicani è la libertà, all'interno di regole precise, peraltro previste e sanzionate da norme che prevedono che qualsiasi pazzo scatenato, sia pure con targhe diverse, debba essere in qualche modo fermato, sanzionato, arrestato, condannato e debba scontare tutto ciò che è giusto che sconti,

ornato dai più grandi artisti di Pietrasanta dell'epoca, e di Vittorio Emanuele. Rimasi basito perché non mi sono mai trincerato e impaurito di fronte alle immagini, andando senza dubbio alla sostanza.

stava occupando indebitamente una casa cantoniera dell'ANAS in località Montignoso, qualcuno esperto di pubblica sicurezza e di *intelligence* mi disse: «Senta, senatore, siamo tutti d'accordo: almeno sappiamo dove sono e li teniamo tutti d'occhio». Francamente non accolsi di buon grado questo tipo di impostazione, ma, con l'aumento dei capelli bianchi in questi ultimi tre anni e mezzo, mi sono accorto che probabilmente quel concetto non era Oggi prendere una "roba" del genere e cancellarla non vuol dire che coloro che ci sono dentro improvvisamente svaniscono; forse scompaiono dai radar, ma non è quello che vogliamo noi. Noi dobbiamo vedere dove sono, tenerli d'occhio e possibilmente impedirgli ogni azione di movimento, perché si tratta probabilmente di delinquenti, maledetti, mascalzoni che vanno portati in galera. Questo bisogna fare. Dico probabilmente perché poi c'è la giustizia, ci sono i tribunali e, quindi, bisogna vedere se arrivano al giudizio o meno, visto che per me sono tutti innocenti fino al terzo grado di giudizio.

che non posso dire qual era, LA7, condotto da Enrico Mentana, notoriamente di sinistra, diceva a vari giornalisti, quasi tutti di estrazione

Chiudo come ho iniziato. Se io, che sono antifascista, iscritto all'anagrafe antifascista, socialista di famiglia, di tradizione e di cultura, repubblicano, fedele alla Costituzione, non la penso come voi sono fascista? No: voi siete fascisti che mi volete trascinare in un buco che non è il mio. *(Applausi)*. È per questo motivo che Forza Italia ha presentato il documento contenuto

Noi convintamente sediamo in questo Parlamento. Siamo leali e fedeli alla Repubblica e alla Costituzione. Ma siamo leali e fedeli alla libertà che deve essere organizzata e seguita con senso di responsabilità e alla giustizia, che viene amministrata - come diciamo noi spesso - non sempre come vorremmo. è sicuramente a loro che lasciamo questo tipo di mestiere e non ci dobbiamo sostituire alla giustizia come Parlamento. In caso contrario, lo stesso Parlamento ricorderebbe molto quello del ventennio.

Presidente, l'Italia sta ricominciando a vivere, dopo mesi interminabili. Portiamo addosso il lutto di oltre 132.000 nostri concittadini che sono caduti per la pandemia, che non è sconfitta e ancora fronteggiamo in parti d'Europa, come dicono i dati allarmanti in Russia, nel Regno Unito di Gran Bretagna e in molte parti del mondo, in particolare i Paesi più poveri, dove mancano i vaccini,

l'Italia, a dimostrazione di come la salute e la sanità gratuita e universale siano il principale bene comune, il cardine di una democrazia e di uno Stato di diritto. Presidente, l'Italia sta ricominciando a vivere e a lavorare e, in particolare, le nostre imprese manifatturiere, che più hanno sofferto negli ultimi mesi. Quando l'Italia prova a ripartire, a costo di sacrifici enormi, c'è chi in modo canagliesco, in maniera organizzata e premeditata, cerca di strumentalizzare le difficoltà e la rabbia per attaccare la democrazia in un momento critico. È quanto cercano di fare da mesi, dall'inizio della pandemia, le organizzazioni di stampo fascista che ancora operano nel nostro Paese. Sigle diverse, ma tutte legate da un filo nero, dal tentativo di aizzare il ribellismo contro

Il pomeriggio di sabato 9 ottobre l'assalto alla sede della CGIL, il principale sindacato italiano, emblema di tutto il mondo del lavoro, è stato a tutti gli effetti un atto eversivo, violento e pianificato; un'azione di squadrismo condotta e apertamente annunciata da esponenti di un'organizzazione fascista, Forza Nuova. L'attacco contro le organizzazioni dei lavoratori è un atto che volutamente ed esplicitamente richiama lo squadrismo fascista che un secolo fa si faceva largo devastando le camere del lavoro, operaie e i luoghi di incontro dei braccianti. Guai a banalizzare o a sottovalutare quello che sta avvenendo. Ha un grande valore, allora - per la reazione unitaria di tutto il Paese che testimonia - la visita immediata del presidente Draghi nella sede della CGIL, perché, di fronte a un attacco eversivo, che è un attacco alla democrazia, a ogni cittadino, a ognuno di noi, abbiamo il dovere di reagire, di dire "mai più fascismi", come migliaia e migliaia di persone hanno scandito a Piazza San Giovanni solo pochi giorni fa, riaffermando l'appartenenza non a una parte politica, ma l'appartenenza ai valori della nostra Costituzione, della nostra Repubblica. Perché la Costituzione nasce dalla Resistenza ed è antifascista, laddove il fascismo è discriminazione, sopruso, negazione dei diritti di libertà e di dignità della persona. L'articolo 3 della nostra Costituzione che afferma i principi universali di uguaglianza e di non discriminazione; che afferma il diritto di ognuno di poter realizzare il proprio progetto di vita, qualunque sia la condizione sociale di partenza, partenza, rappresenta il riscatto del nostro Paese, di tutti noi, dopo l'abominio, dopo l'orrore assoluto delle leggi razziali e razziste volute dal fascismo.

Spetta a ciascuno di noi impegnarsi per impedire che il fascismo possa tornare: ha detto il presidente Mattarella nel gennaio 2018. perché il veleno del fascismo è un pericolo sempre attuale per le nostre democrazie. Oggi si manifesta nelle forme subdole dei discorsi discriminatori e di istigazione che sono enormemente cresciuti durante la pandemia, in particolare in rete, e molto spesso amplificati da false informazioni, da algoritmi per nulla trasparenti, l'antidoto più forte è la memoria, è la testimonianza civile della memoria. Per questo non saremo mai abbastanza grati al presidente Mattarella per aver nominato Liliana Segre senatrice a vita. Gli insulti a Liliana Segre di qualche isolato odiatore sono un'ignominia per tutti noi; l'affetto che ovunque invece le viene tributato, in particolare dalle nuove generazioni, è la speranza vitale che abbiamo. Presidente, tra le norme contenute nella nostra Costituzione, ci sono gli strumenti per difendere la nostra democrazia da atti violenti ed eversivi, come quello dirompente del 9 ottobre, o da altri innumerevoli, meno eclatanti, ma altrettanto pericolosi, come le continue minacce e intimidazioni ai giornalisti che indagano sulla rete del neofascismo. Ci sono strumenti che vanno utilizzati, e per questo chiediamo lo scioglimento, a norma di legge e sulla base del dettato costituzionale, di Forza Nuova e delle altre organizzazioni fasciste. con una mozione, Presidente, che fino all'ultimo abbiamo chiesto a tutte le forze politiche, di ogni colore, di sostenere. Ma così non è stato, e questo è un rammarico grande, ed è anche un problema per la nostra democrazia. Perché l'Italia ha bisogno sia una destra europeista, capace di dirsi "antifascista", nel solco della Costituzione. Ma così ancora non è, e lo dimostrano, ancora una volta, le parole ambigue di Giorgia Meloni e di Matteo Salvini. A chi ancora avesse difficoltà a riconoscere quale sia la matrice dell'attacco squadrista del 9 ottobre, diciamo di andare a vedere le foto, le svastiche tatuate sul braccio degli assalitori.

una notte intera medici e infermieri al pronto soccorso del Policlinico Umberto I non ha nulla a che fare con i lavoratori, con i cittadini, con le famiglie che, tra mille difficoltà, danno il massimo per portare l'Italia fuori dal *tunnel* della pandemia. È a loro, ai loro bisogni, alle loro ansie e alle loro aspettative che noi e la nostra democrazia dovremo dare risposte. *(Applausi)*. Signor Presidente, membri del Governo, colleghi senatori, io spero e sinceramente mi auguro di non mancare di rispetto ad alcuno nel sostenere che stiamo perdendo di vista il senso della realtà. Come spesso capita nel nostro complicato Paese, il combinato disposto tra calcoli politici di parte, tic ideologici in buona fede e la naturale emotività del dibattito pubblico ci sta portando a perdere di vista la realtà. La realtà, colleghi, è che non non siamo all'alba di un ritorno in auge del fascismo. Il paragone tra l'Italia di oggi e l'Italia del 1921 è ridicolo, oltre a essere offensivo oltre a essere offensivo per la memoria di chi il fascismo, quello vero, lo ha veramente avversato. *(Applausi)*. La realtà, colleghi, è che stiamo parlando di una forza più simile a un movimento da stadio, frequentato da criminali più o meno comuni, inclini allo spaccio e alla delazione, che alle ultime elezioni cui si è presentata, le europee di due anni fa, non molto tempo fa, ha preso lo 0,15 per cento è il vero seguito di Forza Nuova. *(Applausi)*. La realtà, colleghi, è quella perfettamente rappresentata dal Capo dello Stato quando ha detto che l'aggressione alla CGIL è un fatto che turba, ma non preoccupa. *(Applausi)*. Queste sono state le parole del Capo dello Stato: giusto turbarsi; giusto punire con il massimo della pena e tutte le aggravanti di legge possibili chi ha commesso quei fatti; assurdo preoccuparsi. E sarebbe opportuno che i rappresentanti del partito di cui il Capo dello Stato è espressione aderissero al senso, oltre che alla lettera, di quelle parole. Il senso è quello di evitare che, drammatizzando, le cose peggiorino anziché migliorare. Naturalmente, sarebbe opportuno che tutti quanti abbassassimo i toni. Io ho trovato a dir poco sconveniente l'evocazione della strategia della tensione. È evidente che ci sono state delle gravi sottovalutazioni da parte dei responsabili della pubblica sicurezza lo scorso 9 ottobre. È evidente che sono stati commessi degli errori gravi. È naturale che responsabile politico di quegli errori e di quelle sottovalutazioni sia il Ministro dell'interno. È legittimo che chi sta all'opposizione ne chieda la testa, se ritiene opportuno chiederne la testa. È sconsiderato evocare la strategia della tensione. È sconsiderato, perché non si delegittima la persona, il Ministro dell'interno in quanto tale, ma si delegittima la funzione che la persona ricopre. Si delegittima quello che Cossiga riteneva fosse il Ministero più delicato, sensibile e potente della Repubblica: il Ministero dell'interno. Si crea un clima per cui si diffonde nell'opinione pubblica una sensazione di sfiducia e di sospetto, non nei confronti dell'attuale Ministro dell'interno, ma nei confronti delle istituzioni tutte. E questo, chiunque abbia senso della realtà e dello Stato, non lo fa. Evita di farlo; semplicemente evita di farlo, colleghi. *(Applausi)*. Poi, naturalmente, stiamo assistendo a una rappresentazione un po' di comodo, che tace una parte della verità. Ora, cos'è che fa orrore del fascismo a occhi antifascisti e democratici? La violenza e la prevaricazione. Vi racconto tre episodi, avvenuti in quella che è stata recentemente definita la città più progressista d'Italia. Si tratta di Bologna, ma episodi del genere sono avvenuti, avvengono e temo che avverranno in tutte le città italiane. Il protagonista di questi episodi è il Collettivo Universitario Autonomo, acronimo CUA. durante una riunione del rettorato. Irrompe un manipolo del CUA di 30 persone, che mette a soqquadro i locali e appende un cartello al collo del rettore, un cartello ovviamente denigratorio. Il povero rettore di allora, Ivano Dionigi, un illustre latinista, persona più che mite,

di pascolo di giovani non iscritti all'università, vengono impiantati dei tornelli all'ingresso, e possono accedere solo gli iscritti all'università, un modo per garantire il diritto allo studio. Sia mai! Al grido «Riprendiamoci la nostra università!» il manipolo consueto del CUA irrompe, divelle i tornelli, mette a soqquadro i locali e impedisce agli studenti di fruire di quella biblioteca per lungo tempo. Terzo episodio: Angelo Panebianco, capofila alla scienza politica italiana, uomo di solida cultura liberale, quindi un nemico del popolo, tiene la sua lezione a Scienze politiche; la lezione viene interrotta, Panebianco viene aggredito, minacciato, ridotto al silenzio. Ora vi posso dire, con cognizione di causa, non solo che non ci fu alcuna mobilitazione, alcuna chiamata alla difesa della democrazia, alcun appello editoriale dei grandi giornali nazionali, anche impossibile per il giornale della città trovare un solo professore universitario, collega di Angelo Panebianco, disposto a dare un'intervista non in solidarietà di Panebianco, ma in difesa di quei sacri principi che tutti quanti noi ci onoriamo di rappresentare. Perché qualcuno era connivente ideologicamente con i violenti del CUA e la maggior parte aveva paura: aveva semplicemente paura, colleghi. Allora, esiste il fascismo nero, come esiste quello che Amendola definiva il "fascismo rosso". Se mi avessero detto che avrei rimpianto il vecchio PC, non ci avrei creduto, ma è così: i fascisti rossi esistono e il vecchio PC li riconosceva e li condannava al pari dei fascisti neri. Entrambi, quando commettono reati, vanno puniti con il massimo della pena e con tutte le aggravanti possibili, ma né l'uno, né l'altro rappresentano una minaccia per la democrazia, con tutta evidenza, come ha detto il Capo dello Stato. Stato. Colleghi, credo che bisognerebbe essere un po' più realisti, un po' meno ideologici, un po' meno emotivi. Credo che sarebbe opportuno fissare dei principi: violenza e prevaricazione vanno sempre - sempre! - condannati; i responsabili di atti criminali di violenza politica vanno puniti, con tutti gli strumenti che la legge consente. Ma starei attento a sciogliere un partito politico, men che meno a scioglierlo per spinta del Parlamento (tra l'altro viviamo in un quasi stato di eccezione). È una decisione molto, molto scivolosa. Per quanto orrore ci possa fare il partito politico in questione, andiamoci piano. Peraltro, la norma dello scioglimento evidentemente si riferiva a un altro mondo, quando i partiti erano il luogo della mobilitazione, del consenso e della propaganda. Tutto questo non è più in capo ai partiti, che non esistono neanche più - diciamoci la verità esistono i *social* e, quindi, sciogliere per decreto un partito politico non solo non inibisce la sua capacità di propaganda e di mobilitazione, ma indiscutibilmente l'aumenta, e fa del disciolto un punto di riferimento per un mondo confuso, complesso, variegato. Li metteremmo a capo dell'universo no vax e questo non credo che sia nell'interesse di nessuno, davvero di nessuno; oltre ad essere vero - come diceva il collega Mallegni - che scomparirebbero e quindi si renderebbe più difficile

*(PD)*. Signor Presidente, colleghi, se il 9 ottobre non ci fosse stato l'assalto squadrista, di stampo fascista, alla sede nazionale della CGIL dopo poche ore, al pronto soccorso del Policlinico Umberto I, oggi non saremmo qui a discutere sulla richiesta di scioglimento di Forza Nuova. Abbiamo assistito ad atti gravissimi di violenza, caratterizzati da un'inquietante carica eversiva. Abbiamo sentito ieri le parole da parte della Ministra dell'interno: «inquietante carica eversiva», di evidente matrice fascista. Mi sembra che l'abbiamo letto ovunque, lo abbiamo ascoltato ovunque. Strano che ci si interroghi sulla matrice, e Quello del 9 ottobre è stato un vero e proprio attacco alla nostra democrazia, ma soprattutto alla nostra Costituzione. La nostra Costituzione è garante della nostra democrazia. È proprio la Costituzione che detta le regole del dibattito democratico. Si partecipa certamente e liberamente al dibattito democratico se si resta nelle sue regole, ed è sempre solo il rispetto della Costituzione che detta le regole del dibattito. È stata già evocata dagli interventi prima di me la XII disposizione transitoria della Costituzione, pone proprio il limite esterno, molto chiaro, e il confine del dibattito democratico. Il confine esterno posto dalla nostra Costituzione è proprio il divieto di ricostituzione del disciolto partito fascista. Quando ci sono evidenze che ciò può accadere, si può e si deve agire a difesa della nostra democrazia. Si può agire con una sentenza della magistratura o con un decreto del Governo. Ma l'esigenza è sempre la stessa: cambia il modo per perseguirla, ma l'esigenza è sempre quella di protezione della nostra democrazia.

o chiusura di alcune sedi, ma l'articolo 3 della legge Scelba parla di necessità e urgenza. Per arrivare a questo si deve si deve indagare e farlo davvero, non banalizzare e non parlare di folclore. Le indagini ben fatte e approfondite, anche con l'aiuto della legge Scelba, hanno già dato i risultati su questo stesso tema. Nel 1973 è stato sciolto Ordine Nuovo, nel 1976 è stata sciolta Avanguardia Nazionale, nel 2000 è stato sciolto il Fronte Nazionale. Gli strumenti normativi ci sono chiediamo che si proceda a tutela della legalità democratica e repubblicana. Ho detto che i fatti di cui stiamo discutendo non vanno banalizzati, né sminuiti. Quindi è proprio questi fatti che dobbiamo analizzare nel contesto attuale, un contesto che anche nell'Unione europea vede crescere intolleranza ed estremismo. A proposito di intolleranza, vorrei ricordare a quest'Aula che 12 esponenti di Forza Nuova sono stati condannati dal tribunale di Forlì dopo aver inscenato un finto funerale davanti al comune di Rimini, proprio mentre il sindaco, *illo tempore*, celebrava la prima unione civile. L'intolleranza contro qualunque persona venga, a loro parere, ritenuta diversa è un segno specifico dei fascisti. Questo va detto con chiarezza. Non vorrei dover ricordare a quest'Aula l'assalto fascista di Forza Nuova fatto contro la mia stessa persona a Gaeta qualche tempo fa, proprio a ridosso dell'approvazione della legge sulle unioni civili. E ben lo sa il sottosegretario Scalfarotto, che con me combatté per ottenere quella legge. Il neofascismo attuale ammicca proprio a questo: a tutto ciò che è eversivo, a tutto ciò che è ribellismo, occhieggia all'irrazionalità, al sospetto, al complotto contro la scienza, contro la cultura dominante. la cultura dominante. Alla base della saldatura tra questo neofascismo e il ribellismo c'è la rabbia sociale, frutto della frustrazione individuale causata dalle situazioni economiche soggettive in tempi di emergenza pandemica e non solo. È a questa rabbia sociale che si rivolge la cultura sovranista e nazionalista, usando in modo strumentale il disagio sociale. È anche su questo disagio che noi Parlamento dobbiamo intervenire per evitare che le istituzioni nelle quali tutti sediamo - le istituzioni siamo anche noi - siano viste come nemiche. Dobbiamo essere invece luoghi di ascolto e di elaborazione di risposte, perché solo combattendo le disuguaglianze e le solitudini saranno sconfitti tutti gli estremismi.

il senatore Cangini ci richiamava al senso della realtà; io però vorrei che il senso della realtà non offuscasse il senso della storia. Sono passati undici giorni da fatti gravissimi non che hanno minacciato, ma che minacciano la democrazia costituzionale e l'ordine costituito repubblicano; fatti gravissimi messi in atto da forze di dichiarata ispirazione fascista. Non è uno spauracchio fascista, senatore Mallegni, ma è una dichiarata ispirazione fascista. Basta consultare, sfogliare, nemmeno leggere, la loro pubblicistica per farsene un'idea. Oggi il Parlamento si assume la responsabilità costituzionale, prima ancora che politica, di denunciare quei fatti e di proclamare che è la Costituzione il riferimento che come parlamentari ci deve orientare sempre. Non c'è nessuna pretesa fuori luogo, come qualcuno vorrebbe far credere, ma solo la nostra responsabilità parlamentare proclamata con chiarezza e senza infingimenti. Vorrei ricordare in quest'Aula il pensiero di due eminenti filosofi politici tedeschi che hanno studiato il totalitarismo e hanno in qualche modo dedicato la loro vita, non solo intellettuale ma anche personale, per combattere il totalitarismo. Mi riferisco ad Hannah Arendt, la quale diceva che una volta che una forma di governo si è affermata essa può sempre ritornare, al di là delle temporanee sconfitte storiche. La seconda riflessione che vi invito ad approfondire è quella di un altro filosofo, Norbert Elias, il quale a proposito della Germania di Hitler scriveva che il totalitarismo non è stato una conseguenza necessaria, ma solo una conseguenza possibile, e che il fatto che la possibilità si sia realizzata deve farci riflettere sulla fragilità del processo di civilizzazione e sulla necessità di non abbassare mai la guardia nel difenderla. oggi il nostro compito è esattamente questo: non abbassare la guardia per difendere la civiltà nazionale ispirata alla e dalla Costituzione.

stiamo discutendo di un fatto specifico, vale a dire di persone individuate che si riconoscono in una formazione politica individuata e che hanno dato l'assalto a una sede sindacale Non vedo come si possa affermare che sciogliere, come la legge prevede, questo tipo di formazioni, siccome

di una pulsione ancora inneggiante al fascismo, al neofascismo e al neonazismo? Sinceramente non riesco a seguire questo ragionamento e credo che porti a

Vorrei leggere alcune storie: don Giovanni Minzoni, cappellano nella Grande guerra, medaglia d'argento, sacerdote ad Argenta, da sempre vicino ai braccianti agricoli, sostenitore del sindacalismo cattolico fonda circoli per l'acculturamento delle classi più umili, si oppone alle violenze fasciste di Italo Balbo, ucciso a manganellate nei pressi della canonica il 23 agosto 1923. Tina Anselmi si schierò con l'antifascismo quando vide giovani partigiani portati all'impiccagione. Staffetta delle Brigate partigiane, Cesare Battisti entrò nella Democrazia Cristiana nel 1944 e ne divenne dirigente. Piero Calamandrei, giurista, docente e rettore dell'Università di Firenze, collaborò con Salvemini, fu fondatore e partecipò a Giustizia e Libertà e poi al Partito d'Azione e si oppose alla legge truffa. Dante Livio Bianco fu anch'egli un grande liberale. Ernesto Rossi nel Primo dopoguerra polemizzò con i socialisti per le loro posizioni sui reduci; collaborò al Popolo d'Italia, aderì all'Unione Nazionale di Giovanni Amendola, fu tra i fondatori di Giustizia e Libertà e fece parte del Governo Pardi per poi essere, più tardi, uno dei fondatori del Partito Radicale. Laura Bianchini, bresciana, durante l'occupazione nazista entra nella Resistenza con le Fiamme Verdi, coordina la stampa clandestina diretta alle formazioni cattoliche e, dopo la liberazione, è membro della Costituente e poi deputata eletta nella Democrazia Cristiana. Sono molti altri i nomi che potrei fare, ma il punto è uno solo. La discriminante antifascista fonda l'unità della Resistenza e il patto politico e istituzionale sul quale si fonda la Costituzione; fonda l'unità repubblicana nelle diverse culture politiche animatrici dei grandi partiti di massa e non solo (anche del partito liberale e repubblicano); fonda la democrazia repubblicana post-bellica e la connotazione unitaria e plurale è indissolubilmente legata alla caratteristica democratica, repubblicana e antifascista. Quindi, quando parliamo di antifascismo non ci riferiamo a un momento storico e non possiamo accettare l'idea che sia un qualcosa di superato, è la cifra fondante e unificante della nostra Costituzione e del nostro impianto democratico e liberale. Come ha detto Carlo Smuraglia, l'antifascismo di oggi non è la nostalgia dell'antifascismo di allora, la connotazione che ci rende cittadini democratici. Antifascista è la nostra Costituzione, con un complesso di norme a tutela di democrazia, libertà, unità, dimensione sociale ed equilibrio tra i poteri dello Stato, rispetto, tutela e dialogo con le minoranze, ruolo del Parlamento, dialettica politica come confronto libero e nel rispetto di tutti. Per questo, richiamarsi al fascismo oggi e attaccare la sede di un importante sindacato non è un fenomeno folkloristico, ma è un attacco anche simbolico ed è quindi dirimente

e nel chiedere lo scioglimento di Forza Nuova. Questa è l'unità repubblicana, nel pluralismo e nel riconoscimento pieno dei valori della nostra Costituzione. Questo è l'alto compito cui siamo richiamati ed è lo spirito repubblicano. Non vi è spazio per distinzioni, benaltrismi, strade alternative o vie di mezzo.

Forza Nuova. È vero che lo scioglimento di organizzazioni fasciste spetta al Governo o alla magistratura, ma come parlamentari non possiamo non dare indicazioni al Governo affinché intervenga in questo senso. senso. Noi ovviamente diamo indicazioni, poi il Governo troverà la maniera migliore per dare attuazione alla XII disposizione transitoria della Costituzione e per dare attuazione alla legge Scelba del 1952. Sono state ricordate da vari senatori le diverse sentenze che hanno sciolto altri movimenti neofascisti: nel 1973 Ordine Nuovo, nel 1976 Avanguardia Nazionale e nel 2000 Fronte Nazionale. Parlamento lasciar correre l'attacco alla CGIL che tanto ricorda gli attacchi alle camere del lavoro? No, non può, ma non solo per l'attacco alla CGIL, bensì perché ci sono delle rivendicazioni neofasciste da parte di Forza Nuova,

questo non eliminerà le pulsioni di ricostituzione del partito fascista nel nostro Paese, ma noi abbiamo il dovere, come rappresentanti di un Parlamento che è nato da una Costituzione antifascista, di tenere alte le antenne, di guardare lontano e di prevenire qualunque

queste pulsioni e che non sono delinquenti qualunque - sono stati anche europarlamentari, avevano un Daspo e sono note nel Lazio, a Roma, come persone che da sempre portano avanti queste idee - raggiungessero - raggiungessero la sede della CGIL dopo averlo annunciato? Questo non è solo responsabilità del Ministro, mi dispiace, ma a Roma abbiamo il prefetto Piantedosi, che è stato capo Gabinetto del ministro Salvini, che ho avuto modo di vedere come fosse forte con i deboli quando quest'estate abbiamo fatto un presidio alla discarica di Albano e ha dato il Daspo a un ragazzo di diciotto anni che non può più passare per il territorio di Albano solo per essersi messo per strada a bloccare un camion che portava dell'immondizia non a norma. Eppure è stato forte, il prefetto, in quell'occasione, sapeva benissimo il prefetto, in quell'occasione, sapeva benissimo fare il forte con i deboli, ma non è stato in grado di fare il forte con i potenti e pericolosi, invocando l'ordine pubblico. Su questo ho presentato un'interrogazione, perché è troppo semplice dare la colpa al Ministro quando abbiamo un prefetto.

perché qui abbiamo una senatrice a vita che ha subito tale folklore e veramente, avendo sentito i suoi discorsi, dovremmo essere in grado di capire cos'è fascismo e cos'è antifascismo.

e l'antifascismo e solo all'interno della democrazia si collocano Destra e Sinistra, che hanno il dovere di essere antifasciste e di avere gli anticorpi contro qualunque tipo di fascismo si presenti, con qualunque bandiera esso sia portato avanti.

solidarietà è una debolezza; la solidarietà del dopoguerra è stata un errore, perché ci hanno invaso; la solidarietà nei confronti degli altri, da praticare vaccinandosi, è una debolezza, perché ognuno deve preservare la propria identità, il proprio egoismo. È questo il nuovo fascismo che ci troviamo di fronte. Mi aspetto che questo Parlamento sappia rispondere con forza a questi rigurgiti che non sono per niente innocenti, perché hanno una forza economica e una forza internazionale che come Parlamento non possiamo ignorare. Pertanto, a nome di Sinistra Italiana, ma a nome di qualunque persona democratica, anche se fosse di Destra (non lo sono, ma rispetto una Destra antifascista), voterò a favore della mozione per lo scioglimento di Forza Nuova e di tutte le organizzazioni che inneggiano a queste follie

maturata in famiglia in anni, come potete facilmente immaginare, molto vicini al dopoguerra, in cui lo *slogan* era molto semplice: né fascisti né comunisti. Eravamo molto chiaramente determinati a cogliere, a sapere, a sperimentare che c'era davvero una violenza di Destra e una violenza di Sinistra. Anche negli anni successivi, per esempio con i movimenti studenteschi che si sono avuti attorno alla fine degli anni Sessanta, era evidente che esisteva una violenza di Destra e una violenza di Sinistra. Oggi si vuole collocare la violenza di Destra fuori dall'arco costituzionale, ma è quanto è accaduto finché non è apparsa sullo scenario politico la figura di Berlusconi, che fece quella singolare operazione di sintesi politica di riunire l'intera area del Centro, con un Centro forte, significativo, culturalmente capace di rielaborare teorie e concetti, ma anche

all'interno dell'arco democratico, ma era una violenza possibile, la sperimentavamo: chiunque abbia una certa età l'ha vissuta e noi, che da sempre insieme a tanti amici rappresentavamo il famoso Centro, eravamo lì a difenderci dalla Destra e dalla Sinistra, dall'esperienza di una violenza fisica e dall'esperienza di una violenza intellettuale. Prima il collega Cangini ha

della violenza che appare facilmente sulla stampa. Basta prendere i titoli dei giornali di pochi giorni fa: c'è questa paura che ti porta dire - e vorrei far riecheggiare le parole di una famosa trasmissione di Gigi Proietti

le risorse di chi vorrebbe testimoniare una posizione politica diversa. È indubbio che il nostro no alla violenza vada scritto a caratteri cubitali dovunque e comunque, perché è lo stigma proprio della nostra posizione politica. Un centro è per definizione non violento, è per definizione inclusivo e dialogante, è per definizione aperto ad accogliere e ad ascoltare, ancorché non a condividere, le ragioni dell'altro. Ora io credo, colleghi, che noi siamo in questo momento davanti a questa sfida:

da professionisti, con competenze, con una loro propria capacità di governo, ma comunque guardavano verso un centro. centro. Noi oggi abbiamo davanti questa sfida. Davanti alla ricostruzione dei fatti possiamo accentuarne l'interpretazione che stressa che stressa la dimensione della violenza del singolo, facendola assurgere al rango di violenza di un gruppo non solo di facinorosi, ma addirittura di una parte del Paese, oppure la saggezza, che è quella che assume la violenza come condanna di una responsabilità personale, precisa e concreta per la per la quale non ci possono essere scusanti e che in un certo senso va a cercare anche le complicità. Non è possibile infatti che tutto sia accaduto per uno solo, esattamente come la ricostruzione degli eventi, a cominciare dall'impropria presenza di quel soggetto su quel palco, aveva dietro una serie di connivenze. Andare a cogliere le connivenze e andare a ricaratterizzarle sotto il profilo della responsabilità personale, professionale e politica, è un'azione concreta e positiva che dice alla gente che sta fuori «Guarda» - lo dico anche secondo i famosi versetti - «davanti a te c'è il bene e c'è il male,

detto, far credere che qualunque soggetto che in questo momento ha timore, ansia o preoccupazione davanti alla vaccinazione sia *ipso facto* uno di un raggruppamento eversivo e violento è veramente eccessivo. Posso avere le mie perplessità nei confronti del vaccino. Io ovviamente non le ho, ho già scritto, detto e fatto tutto quello che potevo fare

fatto, nei confronti di chiunque non si vuole vaccinare, chiunque in qualche modo non crede nella scienza. Io sono profondamente convinta che abbiamo bisogno di più educazione scientifica,

Però non possiamo innescare questo corto circuito, preoccupantissimo in chi l'ha fatto, perché allora la violenza del singolo diventa l'ignoranza del soggetto e l'ignoranza del soggetto diventa la demonizzazione della scienza. Troppo, signori! Noi abbiamo bisogno di pace. Se vogliamo che quest'ultima fase della nostra legislatura sia costruttiva

Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi, all'inizio di questo mio intervento voglio esprimere, a nome mio e a nome di tutto il Gruppo Lega per Salvini Premier,

un tale Capitani, presidente dell'associazione "Primum non nocere", l'ha definita come una persona vergognosa che dovrebbe sparire. Da parte nostra c'è tutta la solidarietà nei confronti della senatrice Liliana Segre. Sottolineo che l'autore di questo gesto vigliacco si è da sempre definito antifascista. Voglio al contempo ricordare ciò che è accaduto a Milano alcuni giorni fa, allorquando degli anarchici di matrice rossa hanno cercato di assalire la sede del "Corriere della Sera", la sede della Regione e per ultimo la CGIL milanese. Anche a costoro va la nostra solidarietà, rimarcando che questi facinorosi, che non sono riusciti nel loro intento solo grazie alle Forze dell'ordine, sono anarchici dichiaratamente di matrice rossa. l'occasione per esprimere vicinanza e rispetto nei confronti di tutte le Forze dell'ordine, per il lavoro che stanno facendo soprattutto in questi giorni difficili; sia alle Forze dell'ordine in quel di Trieste, laddove sono state costrette a eseguire purtroppo disposizioni scellerate, sia alle Forze dell'ordine in quel di Genova, dove, non essendoci queste disposizioni, hanno potuto finanche portare la colazione a manifestanti democratici e pacifici. Cosa voglio dire con questo, care colleghe e cari colleghi? Voglio fare una gara per stabilire chi è più violento e chi è meno violento? Assolutamente no. Voglio soltanto ribadire in quest'Aula un dato banale, oggettivo, incontestabile, secondo il quale la violenza e l'intolleranza hanno qualsiasi colore politico e secondo il quale gli stupidi, i delinquenti e i facinorosi li troviamo ovunque. Per cui andare a fare delle divisioni che sono fuori dal nostro tempo e che non hanno una connessione sociale e culturale rispetto all'epoca in cui viviamo è un grave errore politico. Il pericolo fascista è una farsa ed è realistico come un'astronave in un buco nero. Le condizioni storiche, sociali e culturali di quel caratteristico fenomeno totalitario non hanno alcun remoto riscontro nella realtà attuale di nessun Paese. Questo non l'ha dichiarato un burbero nostalgico di qualche decennio fa, ma l'ha dichiarato pochi giorni fa Massimo Cacciari, il vostro Massimo Cacciari, che evidentemente vi sta dicendo che ignorate completamente il contesto nel quale viviamo. Veniamo alle mozioni. ritengo che le mozioni che chiedono lo scioglimento di Forza Nuova e di altri movimenti che vengono definiti estremisti siano politicamente controverse e scivolose - come è stato non ha nessuna competenza e perché mancano i presupposti per addivenire allo scioglimento di questo piuttosto che di quell'altro movimento politico. è giusto rimarcare che l'unico motivo per il quale un movimento può essere sciolto è il tentativo di ricostituire il disciolto Partito fascista. Né l'apologia, né tantomeno le manifestazioni fasciste, né altri sentimenti dei quali ho sentito parlare nei precedenti interventi possono essere causa dello scioglimento di un movimento politico, perché a garanzia di questi movimenti c'è il pluralismo riconosciuto e garantito dalla nostra Costituzione. Dopodiché, venendo ai presupposti e alle competenze, per poter sciogliere un movimento politico per ricostituzione del disciolto partito fascista ci possono essere due condizioni:

oppure la necessità e l'urgenza per cui si procede immediatamente allo scioglimento. È chiaro a tutti che in questo contesto non ricorre né l'uno, né tantomeno l'altro presupposto, per cui avete piazzato oggi qui una bandierina politica nel momento nel quale quest'Aula avrebbe potuto occuparsi di cose ben più urgenti che interessano gli italiani *(Applausi)*, soprattutto in un momento difficile come quello Sorge forte e fondato il dubbio che sta circolando nella società italiana: non è che con il passare delle elezioni stia svanendo anche il pericolo fascista? Se infatti così fosse, il vostro comportamento, l'utilizzare il pericolo fascista strumentalmente, magari anche per fini elettorali, sarebbe una grave, gravissima mancanza di rispetto nei confronti di tutti gli italiani. Se dovessimo Se dovessimo sciogliere Forza Nuova, risolveremmo il problema della violenza e dell'intolleranza? No. È già stato detto prima benissimo: se si dovesse sciogliere un movimento politico estremista, daremmo un'opportunità in più a questi stupidi delinquenti di operare nell'anonimato; daremmo un'opportunità in più a questi stupidi delinquenti di perseguire il loro fine delinquenziale, che significa anche disturbare sacrosante sacrosante manifestazioni democratiche, al di là della condivisione o meno di questi principi. L'invito che rivolgo è evitare di di guardare a fantasmi del passato che non ritorneranno più, ma di concentrarci invece su quello che è lo stato attuale e il rischio attuale, che può essere espressione di chiunque, da destra a sinistra, cercando di reprimere chi non osserva le regole democratiche e agisce con violenza e intolleranza. La sfida attuale rispetto a questo tema è adottare un provvedimento che sia al passo con i tempi e che scongiuri il degenerare, tanto della violenza, quanto dell'intolleranza. La via è soltanto una, quella dell'unità.

per il contesto nel quale si è svolta, ovvero durante il silenzio elettorale, in una città nella quale - la capitale d'Italia - si stava per scegliere il sindaco; avete reso di parte e quindi più debole una manifestazione che poteva e doveva essere la manifestazione di tutti gli italiani,

Che tristezza, poi, proprio nel momento in cui si parla di libertà e di democrazia, aver visto la bandiera del regime sovietico piantata in Piazza San Giovanni quel regime che ricorda la sofferenza dei gulag e la drammatica divisione del muro di Berlino. Bisogna essere uniti per isolare i delinquenti,

La via per arrivare all'unità è una e magari per voi, cari colleghi di sinistra, è anche dolorosa: dovete fare un grande bagno di umiltà, dovete dismettere la vantata superiorità morale, che in realtà non avete mai avuto. Bisogna superare questo vezzo e l'esempio che sia ancora attuale è dato dalla gravissima affermazione del vice segretario del Partito Democratico Provenzano, che si è pronunciato pochi giorni fa. Nessuno - nemmeno il vice segretario del Partito Democratico - deve permettersi di sentenziare che una forza politica

L'Italia ha pagato un caro prezzo su questo conflitto tra buoni e cattivi. Bisogna superare la legge Scelba, così come modificata dalla legge Mancino e soprattutto bisogna superare questo conflitto. Tante sono state le vittime negli anni di piombo e anche dopo, a destra e a sinistra, giovani e giovanissimi. Voglio concludere questo intervento con una frase che mette fine a una rappresentazione teatrale che descrive la drammatica vicenda di Sergio Ramelli, ma che può riguardare qualsiasi ragazzo di qualsiasi parte politica. E quando siete felici e godete della libertà che i coraggiosi vi hanno regalato, abbiate una carezza per loro che sono passati come passa una carezza nel vento. Mai più intolleranza, mai più violenza! Bisogna essere giusti, maturi e responsabili. *(Applausi)*.

mozioni nn. 422, 423, 424 e 425 sono ritirate e trasformate nell'ordine del giorno G1.

Presidente, volevo scusarmi per avere disturbato l'ordine dei lavori e per non essere potuto intervenire

Sei talmente lontana che è difficile che ti possa contagiare. PRESIDENTE. Per cortesia, abbiamo tenuto un comportamento corretto e regolare su tutto il dibattito, anche se la materia è estremamente delicata.

di stampa che esiste non ero a giocare, ma ho accompagnato Giorgia Meloni al vertice con Silvio Berlusconi e Matteo Salvini. (*Commenti*). Non è una spiegazione e sto chiedendo scusa. Potete avere la bontà di ascoltare due minuti o avete una fretta terribile? Il Presidente ha deciso.

l'esclusione della possibilità di intervenire prima che chiudesse la discussione generale. Capisco che c'è un ordine degli interventi e mi sono scusato, ma si tratta di una prassi tante volte superata per volere della Presidenza e della cortesia dei colleghi. Mi duole che in questo caso su un tema su cui sono l'unico dell'opposizione a intervenire si sia ritenuto di registrare l'impossibilità di intervento in maniera così rigida. Presidente, avrei detto che il Gruppo Fratelli d'Italia è compatto nelle sue motivazioni; non è come certa sinistra che in Europa contro tutti i totalitarismi ha votato in maniera

Il presidente Ettore Licheri». Quindi, l'iniziale richiesta si intende ritirata.

se non fosse tragico, sarebbe comico. «Democrazia e libertà!» urlano in piazza i neofascisti; proprio loro, i nostalgici di un regime che ha privato della libertà di parola e ucciso chi lo denunciava. Cosa avrebbe fatto il loro Mussolini con i no mask, no vax, no pass, con quelli per i quali l'unica legge è la trasgressione alla legge? È un grande lusso gridare alla dittatura in una democrazia; soprattutto è una vera e propria truffa evocare un'ideologia della sottomissione dei singoli per parlare di libertà calpestate. Per dire cosa sono stati Hitler e Mussolini e cos'è stata la dittatura, basterebbe rileggere gli scritti dei sospettati di omosessualità e dei dissidenti politici; basterebbe chiederlo alla comunità ebraica, ma anche i sudtirolesi possono raccontarlo: quel regime disprezzava tutto il diverso e i diversi, voleva costringerci a diventare italiani a tutti gli effetti, ha vietato la nostra lingua e le nostre tradizioni e cambiato i nomi delle nostre città e perfino i nostri cognomi. Anche dopo la fine del regime, il Sudtirolo è stato un campo di battaglia per i neofascisti, che hanno fatto di tutto per far saltare l'impegno per la convivenza pacifica tra le due culture, tanto che, a distanza di anni, ancora troppi italiani scambiano quelli del fascismo con i simboli della cultura italiana. Per questo siamo particolarmente sensibili al risveglio di un'ideologia che ha avvelenato i pozzi del nostro vivere civile anche dopo la sua caduta. È per questo che, a inizio legislatura, abbiamo depositato una proposta per l'estensione della legge Mancino a tutte le forme di propaganda fascista. problema, infatti, è che l'Italia non ha mai fatto davvero i conti con la propria storia. C'è troppa tolleranza nei confronti di quelli che elogiano il duce e gli anni del regime; troppa condiscendenza verso il saluto romano e certi modi di dire del ventennio; troppa indulgenza verso la simbologia fascista, sbandierata per la vendita di bottiglie di vino, portachiavi e calendari. Non si tratta, come sostiene qualcuno, di folklore: è propaganda politica, volta a legittimare, soprattutto agli occhi delle giovani generazioni, il ventennio fascista. Per non dire, poi, delle ambiguità e delle capriole linguistiche di alcuni partiti della destra, fino ad arrivare a definire «non chiara» la matrice dello squadrismo del 9 ottobre. Tutto questo ovviamente rappresenta un terreno ottimale per organizzazioni come Forza Nuova, Forza Nuova, nazifascista, xenofoba, razzista, violenta e antisemita, com'è stato stabilito anche da due pronunciamenti della Cassazione, Cassazione, che ha collezionato una quantità di condanne per episodi di violenza, intimidazioni e minacce e che, allo stesso tempo, si batte per una concezione tradizionalista della famiglia, contro l'aborto e l'emancipazione femminile. Con la pandemia per gli squadristi si è aperto un nuovo fronte politico: mettersi alla guida di quell'area magmatica che nega la scienza e vede nel Covid una punizione di Dio e un complotto mondiale per la dittatura sanitaria, il tutto provocando un clima di crescente tensione fino all'assalto alla CGIL, che troppo ricorda le aggressioni alle Camere del lavoro di cento anni fa con cui ebbe inizio il regime. È stata superata la soglia di tolleranza: la politica deve agire. In Germania la legge proibisce ogni forma di elogio del nazismo, dai simboli al saluto nazista. L'unico partito che strizza l'occhio alle organizzazioni neonaziste è l'Alternative für Deutschland (AFD), che in Parlamento è completamente isolato. Nessun'altra forza politica collabora con una che non prende chiaramente le distanze dal nazismo non di rado è accaduto che un politico si sia dovuto dimettere per una frase ambigua. È il momento di fare altrettanto in Italia. Quanto avvenuto il 9 ottobre a Roma rientra chiaramente tra le fattispecie previste dalla legge Scelba, ovvero la denigrazione della democrazia e delle sue istituzioni e la violenza come metodo di lotta politica. Forza Nuova non può essere trattata come un reducismo fuori tempo massimo; ci vuole tolleranza zero per le violenze, le intimidazioni, i messaggi xenofobi e razzisti. Per questo vanno applicate quelle leggi che sono lì per ricordarci che l'Italia si fonda sull'antifascismo, su un'idea di convivenza e di tolleranza che ha permesso di lenire le ferite di tutto il Paese e anche del Sudtirolo. Per tutte queste ragioni, annuncio il voto favorevole del Gruppo per le Autonomie alle mozioni che chiedono lo scioglimento di Forza Nuova. rappresentanti del Governo, vorrei fare una breve premessa, prima di entrare del merito del contenuto della mozione di centrosinistra. Occorre tenere distinti i due piani su cui oggi ci stiamo muovendo. Ho sentito parlare sia ieri, in occasione dell'informativa della ministra Lamorgese, sia nei scorsi giorni, di libertà fondamentali, in particolare di libertà di manifestazione del pensiero. Voglio sgombrare il campo da qualsiasi tipo di equivoco: da un lato, ci sono le libertà fondamentali, che sono tutelate dalla nostra Costituzione; dall'altro, i comportamenti e gli atti del 9 ottobre, che sono da qualificare, per le modalità con le quali sono stati portati avanti, come una chiara espressione di squadrismo neofascista. Lo ripeto: squadrismo neofascista. Questi ultimi non solo devono essere oggetto dell'attenzione della magistratura, che accerterà - come già sta facendo - le eventuali responsabilità penali, ma debbono essere condannati senza esitazione, *in primis* da noi, qui siamo tutti rappresentanti dello Stato. Ci saremmo dunque aspettati l'appoggio trasversale di tutte le forze politiche, comprese quelle del centrodestra, che hanno invece presentato una mozione per condannare, in maniera del tutto generica, ogni movimento eversivo dell'ordine democratico. bene che la condanna coinvolga tutti i partiti o i movimenti che si pongono in contrasto con i valori democratici del nostro ordinamento, ma abbiamo gli strumenti sufficienti per espellere dal perimetro costituzionale un movimento che certamente è di ispirazione neofascista. In via preliminare, basti guardare a chi rappresenta questo movimento: i *leader* di Forza Nuova a livello nazionale, Fiore e Morsello, sono stati condannati in passato per associazione sovversiva e banda armata; lo stesso Giuliano Castellino, rappresentante romano di questo movimento, come sappiamo, è già stato condannato per un'aggressione nei confronti di due giornalisti ed era già stato raggiunto da un provvedimento di Daspo. Anche a non voler considerare i singoli casi, non si può tacere di fronte a metodi di violenza, brutalità, odio e terrore che vengono adoperati in maniera costante da tale movimento. Questi fatti ci hanno riportato alla memoria momenti bui e drammatici che abbiamo vissuto durante il ventennio fascista. La modalità squadrista che veniva adoperata allora per la devastazione e le violenze perpetrate nelle Case del popolo, nelle sedi della stampa e in quelle sindacali - solo per fare alcuni esempi - è stata riproposta il 9 ottobre scorso. La scelta di colpire la sede della CGIL non è casuale: è un attacco al lavoro, che è valore fondante della nostra Repubblica, e dunque è un attacco alla stessa democrazia. Le frasi intimidatorie e brutali che sono state pronunciate nei confronti del presidente Landini ne sono solo la conferma. Come se ciò non bastasse, da quello che si è appreso dalle testate giornalistiche, i vertici di Forza Nuova, attraverso i loro canali *social*, hanno dimostrato di non essere in alcun modo intenzionati a porre fine a simili episodi di violenza, che, al contrario, saranno destinati a ripetersi, se non interveniamo, nelle prossime settimane. È evidente allora che non si tratta di un episodio isolato, ma di un modo di procedere stabile e organizzato, così com'era premeditato l'attacco alla CGIL nella sua sede romana. Di fronte a ciò, è del tutto legittimo domandarsi se lo scioglimento di un movimento politico, sebbene estremista, debba passare dal Parlamento e dal Governo. Noi di Italia Viva-PSI crediamo di sì e in questo non rinveniamo alcun atto di leggerezza. Quello che chiediamo oggi è che il Governo predisponga, con gli strumenti che riterrà idonei e che sono previsti dalla legge, lo scioglimento di una forza politica che chiaramente si pone in senso contrario a ciò che è sancito dalla nostra Costituzione. Si tratterebbe ovviamente di un intervento invasivo, ne siamo ben consci: sciogliere un movimento politico, anche il più antidemocratico, è sempre una sorta di trauma per la democrazia; lo è ancora di più se un simile atto è frutto di un provvedimento del Governo.

che prevede in maniera netta il divieto di riorganizzazione sotto qualsiasi forma del disciolto Partito Nazionale Fascista. L'importanza di un simile precetto si coglie dal fatto che quello previsto dalla XII disposizione è l'unico limite di natura ideologica per quanto concerne la costituzione di un movimento politico dentro un progetto di democrazia aperta. Si tratta di una norma di carattere eccezionale, che muove dall'esigenza di consentire che forze neofasciste, che contemplino tra i loro obiettivi specifiche finalità antidemocratiche proprie di quell'esperienza storica che si avvalgano del metodo della violenza fascista, possano essere disciolte. Sappiamo che la cosiddetta legge Scelba prevede due modalità per procedere allo scioglimento: una segue l'*iter* giudiziario, attraverso una sentenza della magistratura, e l'altra segue la decisione del Governo, attraverso l'adozione di un decreto-legge, in casi straordinari di necessità e urgenza. Sappiamo che quello della magistratura è sicuramente un percorso più lungo; qui siamo invece di fronte a un vero attentato alla Costituzione, che va sventato immediatamente. Si tratta chiaramente anche di una decisione politica. In questo senso, lo strumento del decreto-legge non ammette incertezze sul punto. La gravità dei fatti del 9 ottobre, però, richiama proprio la nostra attenzione. Certo, la magistratura sta muovendo i primi passi per l'accertamento delle responsabilità penali dei singoli autori, attraverso l'adozione di provvedimenti puntuali, ma i tempi per arrivare a una sentenza saranno ovviamente più lunghi. Al contrario, la matrice nera degli attacchi di ottobre richiede un'azione celere e puntuale. Per questo motivo, chiediamo al Governo, con la mozione in esame, di valutare gli strumenti di cui dispone per procedere immediatamente allo scioglimento di Forza Nuova, così come di ogni movimento politico che si ponga in contrasto con i principi ispiratori di uno Stato democratico. Ci rendiamo conto che per avallare questa direzione è indispensabile abbracciare *in toto* i valori della nostra Costituzione e, al contempo, ripudiare tutte quelle forze e quei movimenti politici che strizzano l'occhio ai fascismi. Ciò risulta difficile da immaginare per certe forze politiche che attualmente siedono in quest'Aula, ma che fino a qualche anno fa magari sedevano anche in ristoranti, ritratti in foto, con vertici importanti di CasaPound. modo, lasciamo stare queste polemiche e andiamo avanti in una direzione ben precisa, che è quella di difendere la democrazia e i principi della Costituzione. Certo, è importante che ci sia una mozione come quella del centrodestra, che faccia un passo avanti nella direzione di ripudiare ogni forma di movimento eversivo dell'ordine democratico, ma non è sufficiente.

chiedendo con noi lo scioglimento di Forza Nuova e dando così seguito a quanto prevede il dettato costituzionale. Spero che questo invito non rimanga vano e disatteso. Noi ci crediamo ancora e lavoreremo affinché anche in questo Parlamento, purtroppo non oggi, si possa avviare una fase diversa, con

le trasmissioni televisive, sembrava che la nostra democrazia stesse per cadere sotto i colpi dell'emergenza eversiva e fascista; dopodiché, al momento di discutere di questi problemi, su vostra iniziativa, noi ci siamo e voi siete assenti, lo sottolineo. *(Applausi)*. Il secondo motivo di sorpresa e anche di amarezza deriva dal fatto che questa discussione sui fatti di Roma, ma anche di Trieste e di altre piazze d'Italia, deriva da una gestione sbagliata dell'emergenza pandemica. Questi problemi si dovevano e si potevano evitare con un po' di buon senso e pragmatismo, come abbiamo suggerito

e la curva sud. La conseguenza sono state purtroppo le proteste di piazza, con gli esiti che abbiamo anche conosciuto, perché quella gente cercava semplicemente di far valere le proprie ragioni, giuste o sbagliate che siano.

è che il Parlamento non può sciogliere alcuna forza politica. Questo dev'essere chiaro e lo ribadiamo ancora una volta. *(Applausi)*. Tale compito spetta al Governo o alla magistratura. L'idea che aveva qualcuno di poter cancellare l'avversario politico per via parlamentare, questa sì, tradisce una concezione leninista e giacobina della politica *(Applausi)*: è l'idea

Se la magistratura o il Governo hanno le prove sufficienti per chiudere quell'associazione, lo facciano subito. La domanda invece è un'altra: perché non l'ha fatto prima, visto che erano così pericolosi? Perché ha consentito a queste persone di andare in piazza, arringare la folla e guidare l'assalto alla sede della CGIL? Vorrei essere ancora più chiaro, se serve. Per quello che mi riguarda - ma so di parlare anche a nome dei colleghi del Gruppo - facendo parte della destra politica da quando ero al liceo, ho sempre ritenuto che queste formazioni estremiste, gruppi e gruppuscoli fossero e siano tutt'oggi, per molti aspetti, il nostro nemico più pericoloso. Ho e abbiamo sempre combattuto l'idea di una destra macchiettistica e caricaturale

volte? Detto questo, però, vorrei essere altrettanto chiaro nel dire che non accettiamo che le patenti di democrazia le rilasci la sinistra italiana, perché davvero non ne ha alcun titolo, non le può dare e non le può togliere, perché potrei fare un elenco lunghissimo di situazioni storiche, non degli anni Trenta o Quaranta, ma successive alla fine della guerra, in cui il Partito Comunista e la sinistra politica o quella radicale si sono posti sempre costantemente contro gli interessi nazionali, europei e atlantici. *(Applausi)*. Lo hanno sempre fatto e adesso vorrebbero spiegare a noi cos'è la tutela dell'interesse nazionale, dopo aver difeso i carri armati dell'Ungheria, Praga e l'Afghanistan e dopo aver usato parole di grande ambiguità durante gli anni del terrorismo. Tutto questo, naturalmente, non lo dimentichiamo. lo dimentichiamo. Oggi è il 20 ottobre 2021: ma davvero il Senato della Repubblica italiana pensa che questo sia l'argomento di cui dobbiamo discutere? Davvero dobbiamo ancora rinfacciarci il nostro passato? Davvero non è servito a nulla quanto ha detto un grande esponente della sinistra, l'onorevole Violante, Presidente della Camera, quando ha invitato una volta per tutte gli italiani alla pacificazione nazionale?

quindi cancellate tutte le pagine che abbiamo scritto insieme per cercare di superare la guerra civile strisciante, gli anni di piombo e la rivalità anche armata tra le fazioni. d'Italia, in questo Parlamento, siamo l'unica forza di opposizione: facendo l'opposizione, colleghi, siamo importanti per la democrazia quanto voi che fate la maggioranza. Facendo l'opposizione in questo Senato, facciamo in modo che il Parlamento rimanga tale, perché un Parlamento senza opposizione è un'altra cosa: sono 1.000 figuranti che schiacciano un bottone su ordine di qualcun altro e questo non vogliamo che sia il Parlamento.

anni fa. Abbiamo sempre creduto che l'opposizione sia una scelta, in questo caso di coerenza e di responsabilità, ma non un obbligo, né un destino. Siamo nati per diventare ed essere Destra di Governo e chi governa guarda il futuro, non il passato. Questo è sempre stato chiaro per noi,

che lavorano bene, sono preparati e competenti e servono le loro comunità con onore e responsabilità, rispettando le leggi e la Costituzione bravi come quelli di Sinistra, ma spesso anche di più. *(Applausi)*. È questo che mi dà fastidio, perché noi vogliamo il confronto sulla base delle idee e delle proposte, invece voi vorreste una Destra chiusa negli stereotipi che avete creato!

e, siccome non esiste, la cercate disperatamente, rovistando nella spazzatura e guardando dal buco della serratura.

perché la stagione dell'odio è finalmente alle nostre spalle e non deve più tornare. Mi chiedo però se ciò valga anche per voi nei nostri confronti, perché questo è il discrimine tra chi è democratico veramente e chi lo è soltanto a parole. Vogliamo occuparci dell'Italia, non dei problemi del fascismo e del comunismo, che fortunatamente non esistono più; vogliamo occuparci del futuro dell'Italia, di una democrazia parlamentare a cui apparteniamo non per caso, non per vostra concessione, ma per nostra volontà, sostenuta da milioni di elettori.

Ciò che importa veramente è che questo è ciò che siamo e che pensiamo e vale per l'oggi, ma soprattutto per il domani. È iscritta a parlare la senatrice Gallone. Ne ha facoltà. prima di sedere tra i banchi di questo Parlamento, stavo in classe, facevo l'insegnante di italiano e storia nelle scuole superiori. superiori. Quando mi capitava di prendere una terza classe, quindi all'inizio di un triennio, non era raro che gli studenti mi chiedessero perché fosse necessario studiare la storia, spesso vista solo come un susseguirsi di date, magari difficili da memorizzare. Io invece cercavo di raccontare loro l'importanza e il valore della storia per sapere chi siamo

il sindacato, che è la casa della libertà dei lavoratori. È stato un segnale brutto e forte che chi ha voluto scegliere quello come luogo simbolico per andare a manifestare la propria rabbia, ha utilizzato cavalcando la protesta e la paura di chi magari era in piazza a manifestare pacificamente e si è trovato poi spinto da chi invece, ben organizzato, aveva un altro disegno in testa. Un disegno che ha un nome

Di fronte a tutto questo si procede attraverso quello che la storia ci ha insegnato, né più, né meno, senza cercare di fare distinguo. Dovremmo essere tutti d'accordo sappiamo che la nostra Costituzione, che in questa sede noi tutti difendiamo e che dovrebbe essere la stella polare di tutti noi che abbiamo un ruolo forte ed importante in quanto eletti, parla chiaro: non si può ricostituire il partito fascista. Sulla base di questo il Parlamento aveva un'unica possibilità:

perché ledono il nostro ordinamento costituzionale, perché sono state compiute delle mosse e delle azioni che hanno un significato forte e violento e la Costituzione dice chiaramente

mi sarei aspettata che ci fosse l'accordo di tutti, perché quando si dice che vogliamo semplicemente che venga messo in atto il dettato costituzionale, e quindi vogliamo semplicemente difendere la nostra Costituzione, non diciamo certo che ce l'abbiamo con i partiti di destra. Dovremmo fare un po' di chiarezza e avere un po' di onestà intellettuale tra di noi.

che gli danno la Costituzione e una legge dello Stato per sciogliere un partito che è fascista e si dichiara lui stesso fascista, come abbiamo sentito anche oggi dalle belle illustrazioni fatte

la difendiamo noi quanto la difendete voi. E allora perché continuare a raccontare una storia che non è quella che noi abbiamo scritto con le parole chiare della nostra mozione? Le regole fondamentali del nostro vivere comune dovrebbero essere chiare e inequivocabili; l'antifascismo è una matrice che ci contraddistingue tutti;

di undici giorni dai fatti, siamo qui per chiedere una cosa che è sacrosanta e che dovrebbe essere chiesta da tutti, che non è, ripeto, lo scioglimento ad opera del Parlamento di un partito. Non ci saremmo mai sognati di chiederlo. Noi chiediamo, e questa è una forza propria del Parlamento, di fare in modo che la Costituzione venga rispettata. E allora dove è la notizia? Forse qualcuno non vuole difendere la Costituzione? Forse qualcuno non vede nei gesti del 9 ottobre un attentato alla nostra vita democratica, un attentato a quelli che sono i simboli del nostro vivere comune, un attentato all'accordo che dovrebbe esserci nella condivisione di un piano valoriale che dovrebbe mettere al primo posto la nostra stella polare, che è la Costituzione antifascista nata per quei motivi? Rimango perplessa. Prima il collega Ciriani parlava dell'amarezza nell'affrontare questo dibattito. Io rimango invece perplessa; ho una perplessità di fondo, perché temo che ci sia stata una sorta di strumentalizzazione, piuttosto che invece quello che doveva essere lo spirito giusto di condivisione collettiva e della difesa di una memoria comune,

come se quella parola facesse fatica a uscire. Io ritengo invece che tutti noi, in questa sede, dovremmo essere concordi nel consegnare al Governo con forza una spinta che viene proprio dal Parlamento, per andare in quella direzione, per dire al Governo di usare gli strumenti che sono nelle sue mani. Rispetto a questo non dovrebbero esserci distinzioni: siamo tutti dalla stessa parte.

costruito insieme questa mozione; una grande alleanza a difesa della nostra Costituzione, a difesa dei valori antifascisti e a difesa di una libertà che è patrimonio di tutti, nessuno escluso.

che non stiamo proponendo nulla di ideologico, ma stiamo proponendo di applicare la Costituzione. Colleghe e colleghi, è già stato detto, ma voglio ribadire che io non ho mai pensato lo dico con grande sincerità - che la Resistenza, la Costituzione e la Repubblica (perché è un processo storico quello che ha fatto nascere la Costituzione) fossero una cosa della sinistra. Non sono della sinistra, ma sono del popolo italiano. A questo hanno collaborato tantissime componenti, fin dall'inizio. dall'inizio. È stato il grande capolavoro dei Padri della Costituzione, che ideologicamente erano su posizioni opposte, con scontri pesantissimi; tuttavia, in nome appunto dell'esperienza della Resistenza e della necessità di uscire dal Ventennio fascista, hanno costruito la casa di tutti, tutti, questa, dove siete seduti voi e dove siamo seduti noi. La casa di tutti. Quindi non è un'iniziativa di parte chiedere l'applicazione della Costituzione. Secondo punto:

perfino nei filmati, con i capi di Forza Nuova che guidavano la ribellione, l'assedio e la distruzione delle opere d'arte e degli strumenti di comunicazione. Non dico che siamo nel 1920, ci mancherebbe, ma bisogna fare attenzione: tutto ciò che va in quella direzione per me - e lo dico da sincero democratico

i problemi, i conflitti, i rancori che ci sono stanno mettendo a dura prova la comunità, che è un valore fondamentale, e la stessa efficacia della democrazia. È vero o no? Colleghi e colleghe,

Di fronte a questa situazione in cui c'è un attacco alla scienza, in cui si contrappone la libertà individuale alla comunità,

e non penso affatto che tutte quelle persone siano nemmeno miei avversari. Penso che dobbiamo lavorare tutti senza messaggi ambigui, senza cavalcare l'onda, aiutando a capire lo sforzo che è indispensabile fare per garantire la sicurezza della comunità e la ripresa economica.

perché, se le vostre idee sono diverse dalle mie, lo riconosco e lo accetto come un fatto di democrazia, ma insieme dovremmo dire che queste strumentalizzazioni sono pericolose e inaccettabili. Non capisco la reticenza, non capisco perché sia difficile dire che Forza Nuova è una forza fascista, non capisco perché, visto che voi siete lontani da quella forza.

Da questo punto di vista non ho dubbi: c'è il codice penale. La mia solidarietà va a tutte le persone, uomini e donne, che sono minacciate

piena solidarietà alla senatrice Segre e vorrei anche dire che sono stato dalla parte in cui era, per esempio, Guido Rossa, comunista operaio assassinato dalle brigate rosse.

impegno costituzionale che chiediamo al Governo e sono convinto che sia utile per il Paese, non perché risolveremo il problema, ma perché diamo un'indicazione: diciamo che quella roba lì in questo Paese non può esistere.

i nostri approcci di posizione. Per riprendere le ultime parole del collega Errani, come facevo prima con la mia collega Gallone, è giusto: non vogliamo questa roba qui, ma non vogliamo neanche quella roba là perché la violenza, amici - questo è un dato che dobbiamo tenere tutti presente - è questa roba qui, cioè l'attacco neofascista sfascista del 9 ottobre, e nessuno ha mai avuto alcun dubbio né alcuna reticenza per riconoscerlo come tale, per quanto ci riguarda. È l'attacco - ricordiamocelo - anche a un pronto soccorso dove venivano curate le persone; è un atteggiamento assolutamente eversivo e violento in una piazza della città di Roma, è questa roba qui, amici, ma è anche quella roba là: sono le piazze di Milano, le piazze di Trieste come le piazze di Bologna.

con il vostro approccio di posizione, che ha bisogno di parole chiave: fascismo, antifascismo, scioglimento di Forza Nuova, a cui legittimamente in questi giorni avete detto di non poter rinunciare. Il vostro è un approccio particolare, di sintesi, legato al 9 ottobre; il nostro è un approccio generale, legato a ogni forma di violenza, intolleranza, mancanza di inclusività, totalitarismo comunque configurato. *(Applausi)*. Ho ascoltato con molta attenzione e con profondo rispetto, e devo dire che c'è stato anche molto rispetto nel nostro modo di confrontarci in questi giorni. Non indichiamoci con il dito; ho trovato abbastanza mortificante alcune indicazioni con il dito da parte vostra: «Dovete». Ma cosa dobbiamo fare? Non accettiamo lezioni di democrazia da nessuno, amici, né tantomeno ci permettiamo di darne a voi. Sono, purtroppo, atteggiamenti di matrice politica più che di matrice tecnica. Possibilmente, non dateci neanche lezioni di diritto costituzionale, altrimenti vi dobbiamo rendere la cortesia. Sono approcci politici. Lo diceva un grande scrittore che sicuramente non è nel *pantheon* del centrodestra, anche se noi lo ammiriamo moltissimo. Era lui che probabilmente non avrebbe desiderato essere inserito nel nostro *pantheon.* Sto parlando di Umberto Eco. Ve lo ricordate il fascismo eterno di Umberto Eco? Il fascismo col *timer,* l'antifascismo col *timer*, che veniva fuori ogni volta che c'era bisogno di animare la piazza, possibilmente, normalmente, in occasione di competizioni elettorali. Amici, è legittimo, ma non dateci lezioni di morale e neanche lezioni di stile, perché non siete in grado di farlo su questi presupposti. *(Applausi)*. Noi vi chiediamo di dare un senso al nostro confronto e al nostro dibattito, riconoscendo che

Non è meno simbolicamente oscena quando i Black Bloc, gli anarco-insurrezionalisti, i no TAV, i centri sociali si scagliano contro le vetrine dei commercianti e rubano i loro prodotti? *(Applausi)*. Perché anche per loro è una suggestione molto poco evocativa! O magari quando i proprietari di automobili ritrovano la propria vettura, che magari hanno pagato facendo sacrifici a titolo personale e familiare; distrutta perché qualcuno sta affermando un principio. Come lo vogliamo chiamare questo principio: fascista, antifascista, fascista nero, fascista rosso, fascista verde fascista giallo? È violenza! Punto! Certamente, anche le monetine davanti all'hotel *Raphaël* erano violenza. Hai ragione, Stefania. Se posso permettermi una piccola notazione personale, visto che si parlava di Bologna, a un partito politico è una violenza fortemente evocativa. Il fatto che la sede di Forza Italia a Bologna sia stata distrutta due giorni prima dell'inaugurazione, con le vetrine sfasciate dalle sassate, è ugualmente fortemente evocativo. *(Applausi)*. Non ho visto, però, mozioni. Non so se si trattasse di fascisti o di antifascisti, se si applicasse la XII disposizione, la legge Scelba, la legge Mancino o l'articolo 210 del codice penale. Non ho visto tutta questa solidarietà, amici, ma probabilmente mi sono distratta.

delle considerazioni fatte, appunto, dai colleghi che mi hanno preceduto, per le quali li ringrazio. Quello che è emerso, come diceva il collega Cangini insieme al collega Mallegni, è che l'Italia è sicuramente una democrazia matura, una democrazia evoluta. L'Italia è un Paese libero e che si è sviluppato dal 1943. Perché qui stiamo ancora parlando di 1919 e di 1943, quando si andava in giro con la carrozza a cavalli. *(Applausi)*. Ma oggi abbiamo Internet, YouTube, Instagram e Tik Tok*.* Che senso hanno i partiti politici quando, come ricordava giustamente il collega Cangini, la politica, e non sempre la bella politica, si fa in quelle sedi e in quelle piazze virtuali? Amici, l'Italia ha sviluppato tanti, fortissimi e potentissimi anticorpi per contrastare tutto questo. È abbastanza triste e sa di bancarella dei *remainder*. Un po' come le famose domande che Marzullo fa a mezzanotte e mezza: sei antifascista? Se io sono antifascista e tu non sei d'accordo con me, sei automaticamente fascista? No, amici, no. La penso diversamente da te e, semplicemente, non accetto di essere etichettata in un certo modo, perché libertà significa non dare e non avere etichette. E se non si vogliono ricevere etichette, non le si devono dare, Perdonatemi, ma io ho visto troppe dita, soprattutto negli ultimi interventi, rivolte verso di noi. Io non credo che ci siano qui dentro maestri e discepoli di libertà. Noi siamo l'organo maggiormente rappresentativo. All'interno dell'organigramma costituzionale siamo i più vicini al popolo, e quindi siamo coloro che hanno una responsabilità maggiore

che sosteneva che potesse avere derive troppo autoritarie e convinse gente come Nenni, Dossetti e Moro ad ammorbidirla. Noi riteniamo che tutto questo possa indurre effetti paradossali. Non possiamo parlare dello scioglimento di un partito politico senza pensare che questo potrebbe produrre un effetto vagale di clandestinità, di menti deboli o di pensieri ancora più deboli, che magari trasformano in martiri-eroi i cattivi maestri. Mi scuso per avere preso più tempo del previsto, ma è un tema che ci sta profondamente a cuore e su cui vorremmo fosse fatta la massima chiarezza. Devo dire che il Governo e anche l'altra parte dell'Emiciclo ci hanno aiutato a trattarlo in maniera molto civile. La libertà è di tutti. La violenza non ha colore. Gli atti più terribili sono stati compiuti, purtroppo, con la mano tesa, ma anche col pugno alzato. *(Applausi)*. Quindi, colleghi, evitiamo la violenza comunque configurata. Questa è la nostra missione.

Signor Presidente, dopo i brillanti interventi sia del collega Ciriani che della collega Anna Maria Bernini, non farò a nome della Lega considerazioni di carattere politico, perché non sarei

semplicemente perché, pur condividendo ed essendo favorevoli allo spirito contenuto nella XII disposizione transitoria e finale che vieta la ricostituzione, sotto ogni forma, del disciolto partito fascista, pur condividendo lo spirito della legge Scelba del 1952, non riteniamo giusto e corretto che il Parlamento - e nella fattispecie una maggioranza parlamentare - promuova, peraltro con un atto di indirizzo al Governo, lo scioglimento di un movimento o di un'associazione politica senza un previo accertamento giurisdizionale, senza una sentenza che

Se non c'è una sentenza, il Parlamento non ha alcun diritto di fare pressioni politiche sul Governo. Questo deve essere chiaro. Invece, voteremo a favore della nostra mozione, presentata dal centrodestra, perché nel dispositivo si impegna il Governo a condannare qualsiasi realtà che vuole sovvertire l'ordine costituzionale. anche gli anarchici che andavano a distruggere i lavori dell'Alta velocità, o impedivano che i lavori potessero essere realizzati. Tutti quei gruppi, come diceva bene la collega Bernini, che hanno sfasciato le vetrine - ricordo - a Corso Buenos Aires, incendiando pure le auto. Tutti coloro che hanno assaltato le sedi della Lega per anni e sono rimasti impuniti. Ci hanno pure buttato le bombe nelle nostre sedi e nessuno ha fatto niente. Così come vanno condannati anche "i fascisti dell'antifascismo", come li chiamava Pasolini. *(Applausi)*. Voteremo a favore della nostra mozione, perché noi, a differenza vostra, chiediamo che a seguito dei fatti del 9 ottobre il Governo dia seguito a degli accertamenti e a delle sentenze, che la magistratura dovrà fare, verificando gli atti violenti che sono stati commessi. Noi non sottovalutiamo quello che è successo nelle piazze da parte di questi facinorosi e di questi criminali; assolutamente, guai a sottovalutarlo (ha fatto bene a ricordarlo il ma anche questo Parlamento stia attento a non sottovalutare le migliaia di persone che civilmente sono scese nelle piazze per esprimere la loro legittima opinione Difenderemo sempre il diritto di manifestare. Poi ognuno la pensi come vuole, ma prima di tutto il diritto di manifestare. *(Applausi)*.

Signor Presidente, colleghe e colleghi, oggi discutiamo atti mirati ad adottare provvedimenti per procedere allo scioglimento di Forza Nuova e di tutti i movimenti politici di chiara ispirazione neofascista, perché riteniamo che questa forma di estremismo costituisca oggi un serio attacco alla coesione sociale della nostra organizzazione democratica. A chi puntualizza che Forza Nuova e altre organizzazioni politiche di estrema destra (penso a CasaPound) non siano nate oggi, rispondiamo che questo è vero, ma non possiamo negare che la linea della tolleranza, dell'inclusione e del contenimento adottata finora non sia più praticabile, alla luce dei recenti avvenimenti. Ho letto le mozioni presentate dalle forze politiche di destra, in cui si chiede un'equiparazione tra le forme di violenza neofascista e i fatti del G8, risalenti addirittura a venti anni fa e persino al radicalismo islamico. Vorrei ricordare ai colleghi che la nostra Costituzione è antifascista e prevede il divieto di ricostituzione del disciolto partito fascista: è di questo che stiamo parlando. Inoltre, sebbene l'estremismo islamico rappresenti certamente una criticità da affrontare, esso è afferente alla sfera religiosa e non a quella politica di cui stiamo discutendo oggi. Chiunque osservi con un minimo di attenzione o di onestà intellettuale la realtà socio-politica, deve riconoscere il continuo crescendo di propaganda e intolleranza di stampo neofascista, di ostentazione di linguaggio, simboli e iconografie che fanno riferimento inequivocabile al ventennio. All'apologia astratta, che pure si osserva da anni, si aggiunge un incrementale uso della violenza quale metodo di lotta politica, e questo - come sappiamo - è un chiaro segnale di una potenziale riorganizzazione del disciolto Partito Nazionale Il malessere sociale viene strumentalizzato in modo sempre più frequente da queste formazioni, che propongono soluzioni e modalità di protesta squadriste incompatibili con i valori repubblicani e democratici, valori protetti dalle nostre Forze dell'ordine, alle quali voglio esprimere un sentito ringraziamento e tutta la solidarietà del MoVimento 5 Stelle *(Applausi)* per il loro impegno nell'arginare le derive più violente di questi criminali.

pare piuttosto un tentativo disperato di spostare l'attenzione dalla questione di cui dobbiamo discutere oggi. Nessuno più del MoVimento 5 Stelle sa quanto ogni forma di estremismo ideologico sia contrario all'interesse dei cittadini, ma è sbagliato e dannoso mescolare in un unico ragionamento il crescente rigurgito neofascista con eventuali forme di violenza e intolleranza riconducibili a formazioni di estrema sinistra, perché oggettivamente al momento non c'è alcun livello di allarme. C'è un motivo in particolare per il quale siamo in quest'Aula a discutere le mozioni per lo scioglimento di Forza Nuova e degli altri gruppi: nella manifestazione del 9 ottobre, i ben noti rappresentanti di questa formazione politica hanno promosso un'inaccettabile aggressione alla sede della CGIL che ricorda in modo inquietante gli assalti alle camere del lavoro del biennio del 1921-1922. Diciamolo chiaramente: tale vile atto è un attacco diretto alla democrazia *(Applausi),* e altrettanto inaccettabile è stata l'aggressione al pronto soccorso del Policlinico Umberto I. In questa sede voglio esprimere la vicinanza del mio Gruppo al personale sanitario che è stato brutalmente attaccato. Il giorno successivo a questi inquietanti fatti, con il presidente Licheri e il collega Santillo siamo stati alla CGIL e abbiamo portato la solidarietà della nostra forza politica al segretario Landini. Non so quanti di voi hanno visitato quella sede, vi posso garantire che tali atti di squadrismo, condotti con il pretesto della dittatura sanitaria, sono stati davvero devastanti. Vorrei sottolineare che mi sembra quantomeno ipocrita sentir parlare di dittatura da chi spesso manifesta addirittura nostalgia della dittatura stessa, di quella vera, quella che ha portato alla morte e all'oppressione di milioni di persone. Data la matrice che, anche se non è chiaro a tutti, è fascista *(Applausi)*, la violenza di questi gruppi deve essere affrontata con maggiore rigore, perché è importante sì scioglierli, ma è altresì indispensabile agire subito con determinazione, nel momento esatto in cui tali manifestazioni prendono piede. In estrema sintesi, serve tolleranza zero. Viviamo mesi di complessità senza precedenti, con una pandemia che ha stravolto le vite di tutti noi e ha creato enormi difficoltà economiche e sociali. Sono state prese decisioni importanti, necessarie a contrastare l'emergenza sanitaria che hanno pesantemente inciso sulle libertà e sulla quotidianità di ogni cittadino. Ancora in questi giorni, il Governo ha adottato nuove misure di estrema delicatezza. Tutto ciò ha generato un legittimo moto di protesta che è sfociato in manifestazioni pubbliche. A mio avviso, è però fondamentale distinguere e proteggere chi pubblicamente palesa il proprio dissenso pacificamente, come previsto e garantito dalla nostra Carta costituzionale, da chi invece, infiltrandosi in tali manifestazioni, le strumentalizza con l'intento di sovvertire le strutture democratiche. È gravissimo che questo malessere venga sfruttato da formazioni politiche che non puntano certo a difendere le libertà costituzionali ma, al contrario, a diffondere ideologie liberticide, violente e intolleranti. Sono proprio la gravità delle loro azioni e la particolare delicatezza della fase storica a imporci una diversa postura verso le formazioni politiche che richiamano a metodi, simboli e idee del fascismo. La condanna di ogni forma di intolleranza e manipolazione del disagio devono unire in un solo fronte democratico tutte le forze politiche, così come unitarie dovrebbero essere le azioni conseguenti. Purtroppo, invece, così non è. Dalla Lega e da Fratelli d'Italia abbiamo assistito a un atteggiamento ambiguo che non ci aiuta a difendere i valori repubblicani che si basano sull'antifascismo, perché la nostra Costituzione è antifascista. La realtà, cari colleghi, è che si ha tanta timidezza a dissociarsi chiaramente perché quei mondi rappresentano un bacino elettorale e di finanziamenti poco cristallini. Giorgia Meloni ha addirittura lasciato in sospeso il dubbio su quale fosse la matrice dei fatti accaduti il 9 ottobre scorso. Si tratta francamente di un'uscita surreale e desolante, esattamente come gli assurdi contrattacchi all'inchiesta di Fanpage, che ha svelato un impressionante sottobosco di nostalgici del fascismo e addirittura del nazismo, con consuetudini, simboli e ostentazioni di camerati orgogliosamente militanti e mimetizzati nelle fila di Fratelli d'Italia. *(Applausi)*. Ma c'è dell'altro. Periodicamente dalle Regioni, dai Comuni e persino da un Municipio di Roma saltano fuori altri esponenti del partito di Giorgia Meloni che tradiscono in pubblico un'irrefrenabile nostalgia nera che rappresenta un brutto passo indietro rispetto al percorso di moderazione che la destra italiana aveva compiuto alcuni anni fa. Concludo dicendo che la custodia della memoria della storia del nostro Paese e la condivisione dei valori che hanno fondato la Costituzione sono i pilastri su cui ogni forza politica deve costruire i messaggi e le proposte che sottopone ai cittadini. Mentre attraversiamo una fase storica drammatica, non possiamo consentire che qualcuno si permetta di fomentare la disperazione per rinforzare nella società il germe dell'odio. Per questo motivo, preannuncio il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle all'ordine del giorno

Tutti i reparti dell'ospedale di San Francesco soffrono la grave carenza di personale, in particolare di medici. Si tratta dei reparti di ortopedia e di chirurgia, che non stanno più accettando ricoveri, di radiologia, stanno per essere trasferiti altri due medici, di ginecologia e oncologia trasferito di recente in un altro piano. Tutti questi reparti rischiano la paralisi. Non si tratta di un allarme preventivo per il futuro, perché già oggi i pazienti nuoresi sono costretti a recarsi in altri poli sanitari, a Sassari, a Cagliari, o peggio a rivolgersi alla sanità privata, con conseguenti ingenti costi per le famiglie. La medicina territoriale è quasi inesistente; nei paesi mancano i medici di base e i pediatri. E non si pensi che tutto ciò sia dovuto alla pandemia e alla conseguente riorganizzazione emergenziale degli ospedali: sono criticità evidenti da tempo, che avevamo sollevato già prima dell'arrivo del Covid. Siamo di fronte alla compromissione quotidiana del diritto alla salute dei cittadini e la Regione Sardegna deve assumersi la responsabilità di questi disservizi e l'onere di risolverli in fretta.

si fermi e cerchi di risolvere la situazione, perché l'intento sembra proprio quello di voler smantellare l'ospedale di Nuoro e quello di Sorgono, a favore di altri poli sanitari come Sassari e Cagliari. Se è così, lo si dica chiaramente, si dica chiaramente quali sono le intenzioni politiche, perché in questo caso i cittadini nuoresi non lo permetteranno. *(Applausi)*. Signor Presidente, mi rivolgo a lei con riferimento a quello che è successo la settimana scorsa nella trasmissione «Non è l'arena», condotta da Massimo Giletti, intitolata: «Toscana e veleni». Abbiamo visto, purtroppo, come in una zona ben precisa viene versata dell'acqua visibilmente non perfettamente pulita. Abbiamo visto poi il famoso *keu* distribuito, secondo l'inchiesta, in dieci zone della Toscana.

responsabilità politiche hanno un nome ben preciso: la Regione Toscana - perché poi in televisione dicono che è colpa di tutti i politici - è sempre stata governata dalla sinistra e la responsabilità

per sistemare questa situazione, perché i cittadini sono fortemente preoccupati per la loro salute. Parlano tanto di ambiente, ma mi sembra che in Toscana dell'ambiente gliene importi

Nel Documento programmatico di bilancio approvato dal Consiglio dei ministri si prevede, infatti, la proroga del superbonus al 2023 per i soli condomini: una doccia fredda per migliaia di cittadini che vivono in unità abitative unifamiliari indipendenti e che erano in attesa di beneficiare di queste misure per migliorare la propria abitazione. Oggi ho apprezzato molto che il presidente Draghi in sede di replica abbia richiamato gli interventi di numerosi colleghi che si era scrupolosamente appuntato; purtroppo, però, ha dimenticato proprio di fare riferimento al superbonus, nonostante ne avessero parlato praticamente tutti. Non mi sono demoralizzato: ho preso carta e penna e gli ho scritto immediatamente un foglietto che gli ho consegnato in Aula, pregandolo di rivedere questa ipotesi poco lungimirante. Non intendo citare alcun numero. Ormai le potenzialità e gli effetti positivi di queste misure sono più che evidenti. intervenire soltanto sui condomini significa depotenziare sensibilmente la loro efficacia. Aggiungo che si devono prorogare tutti gli altri *bonus* edilizi come quello sulle facciate: non si consuma suolo, si efficientano gli edifici e i pagamenti sono tutti tracciati. Come si fa a lasciare nel dubbio intere filiere? Sto parlando di una misura che ha ricevuto sempre tante belle parole in quest'Aula da parte di diversi colleghi appartenenti a tutte le forze politiche,

non vi voglio tediare con alcun numero, ma vi porto nel mondo reale dove accade quanto segue. Stamani Vittorio, un amico di Torino ingegnere elettronico, mi ha mandato un messaggio esprimendo tutta la sua delusione per la notizia. tenore: tante promesse, tanti proclami tre giorni prima delle elezioni poi niente; stamattina ha chiamato il direttore dei lavori e il termotecnico per bloccare;

avete detto che questo era uno dei motivi validi per essere entrati e rimanere al Governo: difendere il superbonus che con voi dentro sarebbe stato intoccabile. Che cosa è accaduto? Concludo citando Francesco Serra di Bologna: ci sono centinaia di migliaia di aziende e professionisti che hanno lavorato per dodici-diciotto mesi a fare progetti e preventivi, da rifare ogni tre settimane perché i prezzi aumentano continuamente, con la promessa di essere pagati quando apre il cantiere, perché prima ovviamente non si può o si perde l'agevolazione su queste spese. Adesso salterà gran parte dei progetti e che si fa? Tantissima gente dovrà sborsare 5.000 o 10.000 euro ai professionisti per progetti che butterà via perché la proroga non è arrivata. messaggi come questi ne ho senza soluzione di continuità. Non possiamo diventare il Parlamento dove si bloccano o depotenziano le misure efficaci. In conclusione, mi auguro che il Governo ci ripensi. Signor Presidente, in questi giorni si è molto parlato delle indagini riguardanti il commissario per l'emergenza Covid Domenico Arcuri e constato che le numerose interrogazioni che sono state presentate su vari aspetti della sua gestione non hanno mai avuto risposta. La magistratura deve fare il suo lavoro, lo farà e lo sta facendo, ma il Parlamento non può essere ignorato. andava avanti addirittura per DPCM, poi per decreti-legge; il ruolo del Parlamento è già abbastanza sacrificato, e il ruolo ispettivo non va dimenticato.

del 16 settembre del 2020, sulla questione dei famosi banchi a rotelle, sul loro costo, sul perché sono stati comprati in una certa condizione e non in altre; finestra"), riguardante il caso di un bambino che ha subito delle rappresaglie per non aver partecipato a una celebrazione dell'ideologia *gender* a scuola, in un prestigioso istituto pubblico. Richiamo poi

dell'acquisizione delle quote dei Benetton in Aspi a un prezzo che farà spendere agli italiani 8 miliardi in più di quello che sarebbe possibile: un bel regalo per i Benetton, responsabili della gestione che ha portato al crollo del ponte Morandi con 43 vittime. Sono numerose le